se il Parlamento, in particolare il Senato, rispondesse all'assunto di essere il pilastro della Repubblica parlamentare, credo che tutti potrebbero serenamente firmare la mozione che noi abbiamo presentato. È una mozione molto serena, che prende in esame alcuni fatti che si sono verificati ed esprime dei giudizi che sono propri di un Parlamento, di una Repubblica parlamentare fatta di parlamentari indipendenti e che hanno una certa consistenza e deontologia. Purtroppo non è così, e quindi anche questa discussione, che avrebbe dovuto prendere in esame certi comportamenti indubbiamente sorprendenti, invece, come al solito, ad una battaglia tra maggioranza e opposizione, ad un compatto spirito di contrarietà nei confronti della nostra mozione, da quella parte, e ad un compatto sostegno da questa, continuando ancora una volta a rendere assolutamente insignificante la funzione che questo Parlamento dovrebbe svolgere.

di un illustre Vice ministro nello svolgimento delle proprie funzioni. Che cosa ha fatto di disdicevole il vice ministro Visco?

perché ha cercato di inserirsi, in competenze del comandante della Guardia di finanza, senza che questo gli toccasse.

altro mio ministro fu l'onorevole Formica, ma nessuno mai ha assunto un atteggiamento del tipo di quello adottato dal vice ministro Visco, il quale ha violato le norme. Non solo, ma ha anche cercato di convincere il comandante e ufficiali della Guardia di finanza che gli muovevano delle osservazioni sul suo desiderio di cambiare immediatamente quattro uomini della Guardia a Milano,

ad un certo punto, ha usato toni arroganti, è passato anche alle minacce, dicendo al generale: «Guardi che se lei non ottempererà, succederà quello che succederà».

stavano esaminando, studiando, indagando su certe porcherie del mondo finanziario. Il generale Speciale ha preso atto, ha anche preso in considerazione la richiesta del suo Vice Ministro, ha variato il piano e ha iniziato le procedure, resistendo all'imposizione del Vice ministro di agire immediatamente contro legge.

con buona pace di qualsiasi politico), né questioni di carattere funzionale (la magistratura di Milano chiedeva di continuare a disporre dei quattro ufficiali ai quali un mese prima aveva fatto

A questo punto, visto il polverone che aveva alzato il vice ministro Visco, ci si sarebbe aspettati che esplodesse, che procedesse contro il generale Speciale; invece si è immediatamente afflosciato e non è successo nulla:

e l'atteggiamento fermo del generale Speciale hanno bloccato la mancanza di rispetto delle norme e delle leggi fatta dal vice ministro Visco, e tutto sarebbe finito. e tutto sarebbe finito. Nel frattempo, il Presidente del Consiglio - non so chi consigli il Presidente del Consiglio e anche il ministro Padoa-Schioppa, al quale mi legano motivi di stima e di affetto reciproco e di affetto reciproco - viene in Parlamento a rispondere ad un'interrogazione che si riferiva al ventilato trasferimento e afferma: ma no, il trasferimento avverrà, è tutto normale, è un normale trasferimento, tra l'altro, dicendo anche una panzana - che gli fanno dire - perché poi il trasferimento non avviene, quindi siamo addirittura al ridicolo nei confronti del Presidente del Consiglio. Dopodiché, il quotidiano «il Giornale» pubblica la deposizione di Speciale, esplode di nuovo il caso e questa volta diventa di dominio pubblico. Il vice ministro Visco immediatamente afferma che sono tutte bugie, salvo poi, due giorni dopo, rassegnare le deleghe, non per un atto di deontologia e di correttezza, ma perché ha paura che, dopo le affermazioni di Di Pietro e di altri, qui vada a finire che venga approvata la nostra mozione. Anche qui - mi rivolgo specialmente a lei, signor Ministro - se il Vice ministro avesse rassegnato le dimissioni, finiva quasi quasi per fare una bella figura, perché tutti avrebbero detto: beh, vedi, dignitosamente ha data le dimissioni; invece no, decidete che lui dà le dimissioni, ma sferra il calcio del mulo, il colpo di coda, pretendendo che lei mandi via il generale Speciale. Abbiate pazienza, il fatto era accaduto un anno fa: se il generale Speciale - adesso qui purtroppo non conosciamo la motivazione per cui parliamo per ipotesi,

Perché di grande errore si tratta. Non parlatemi poi di promozione del comandante della Guardia di finanza a magistrato della Corte dei conti, perché - con tutto il rispetto per la magistratura contabile - c'è un abisso tra il prestigio, la valenza,

l'onorevole Vincenzo Visco, si sa, non è certo uno dei beniamini del popolo del centro-destra e di chi nelle istituzioni lo rappresenta.

che fa della spremitura del comune cittadino - che non sia riconducibile alla categoria, ormai specie protetta, del lavoratore dipendente a reddito basso - prima ancora che un prassi comune, una sorta di dovere morale. I demeriti politici delle successive torchiature di cui l'onorevole Visco si è fatto vassallo per ben due legislature sono in questi giorni sotto gli occhi di milioni di cittadini alle prese con le dichiarazioni dei redditi. Oggi dobbiamo però ringraziare l'onorevole Visco, con i suoi modi caratteriali, o per meglio dire forse un po' inurbani e prepotenti, se è riuscito a strappare quel velo, ormai consunto, che assegnava - comunque e a prescindere - alla Sinistra una sorta di superiorità morale nel rapporto con i Corpi indipendenti dello Stato. Che esagerazione quelle lettere e quelle parole. Ma meglio, molto meglio questa esagerazione che gli atti successivi, così melliflui, così cerchiobottisti, così sottilmente ipocriti che arrivano da altri Palazzi. Meglio la sua prepotenza che i tentativi delle belle penne italiane di intorpidire le acque, di fare dell'onorevole Visco l'Orlando in campo nella lotta. Leggo su «la Repubblica»: «... contro una varietà modernizzata della loggia P2, di cui il generale Speciale sarebbe punta di diamante». Bella lezione di superiorità morale! Un servitore dello Stato denuncia indebite e interessatissime pressioni da parte di un Ministro (sia pure in formato *mignon*), e il risultato qual è? che a pagare è il servitore dello Stato e che solo le sopracciglia alzate di chi, nella maggioranza, cerca di mantenere un residuo di dignità, inducono sua eccellenza l'onorevole Visco a farsi da parte. Cerchio e botte. per chi, servitore di questo Paese, ha un residuo di senso dello Stato. Se il generale Speciale avesse mentito, sia colpito col massimo rigore, ma se avesse detto la verità - come credo sia sull'onorevole Visco a cadere la scure della censura, innanzitutto politica, ma non solo politica. Lo dobbiamo, tutti, alle migliaia di servitori dello Stato, che ancora oggi, verrebbe da dire, con romantica dabbenaggine, credono a parole quali autonomia e indipendenza. Lo dobbiamo al COCER della Guardia di finanza. Lo dobbiamo a cittadini che vogliono trasparenza e serietà e il cui nervosismo di fronte a una casta presentata come impunibile e intoccabile sta montando in rabbia. Si parla tanto di costi della politica. Ma il costo delle immoralità politiche è più alto di qualunque indennità. *(Applausi parlare di "Religione civile", di concorso di tutte le forze democratiche a creare un clima di rispetto, se si calpestano le elementari fondamenta dello Stato moderno. Inutile richiamarsi al 2 giugno e alla Costituzione, se «Il Re tentenna» di questa coalizione ha perso ogni residuale barlume di lucidità per comprendere che nel caso Visco-Speciale non sono in gioco due carriere e due storie personali, ma la capacità e la volontà di distinguere il bene dal male, il vero dal falso, senza cui non c'è possibilità di operare, in maniera magari non condivisibile, ma perlomeno giusta e corretta.

sospiro fatto in apertura di intervento dal generale Ramponi quando ha detto: ah, se fossimo un Senato nel quale si prende un problema che ci tormenta e ci divide e si potesse discuterne, come se si fosse davvero tra persone politicamente responsabili, come di un problema vero, per quello che è, per quello che ci appare, per quanto ci preoccupa e ci tormenta! Non è il caso. Perché non lo è, purtroppo? Perché una cornice mediatica immensamente più forte di noi sta intorno ad un argomento come questo e ci impone di affrontarlo, di discuterne, di parlarne finché questa cornice mediatica vorrà, perché questa è la condizione dell'Italia in questo momento. Nulla è cambiato, da questo punto di vista, tra un'elezione e l'altra, tra un periodo e l'altro. Chi ha visto la trasmissione «Porta a Porta» di ieri sera sa che ci sono servitori dello Stato e servitori. Il servitore di ieri sera, nella veste o meglio nel travestimento di moderatore, incalzava, come un accusatore implacabile, i protagonisti Violante e Russo Spena

dell'unico potere per il quale siamo qui in questo momento a svolgere l'odierno dibattito. L'ha deciso colui che ieri ha lanciato lo sciopero fiscale:

dovete soffiare con tanta passione sulla casa dei tre porcellini, perché il lupo mannaro deve soffiare con tutte le sue forze, come state facendo oggi. La risposta è molto semplice: bisogna colpire l'uomo del fisco; bisogna tornare alla libertà incontaminata

il licenziamento arbitrario, in tronco, con raccomandata con ricevuta di ritorno, di Enzo Biagi, che è avvenuto senza neppure

che il suo giornalismo - quello del più grande giornalista italiano - era criminoso; è bastato quello perché il direttore generale della RAI passasse immediatamente al licenziamento. Vorrei sapere dove eravate, difensori della libertà, quando Enzo Biagi è stato licenziato;

Dal momento che i cittadini purtroppo credono - ma per fortuna non è vero - che vi sia uno scontro tra le Forze armate ed il potere politico in Italia, vorrei rivolgere

Dal punto di vista della democrazia americana, questo Ministro può dire al militare quello che è detto in questa lettera. Vi potrei ricordare che i generali rimossi dal comando dell'Iraq durante quella terribile guerra sono stati sette: ogni volta che si sono trovati in disaccordo con il Presidente degli Stati Uniti sono stati rimossi entro la giornata, senza che ciò creasse un problema né per la democrazia americana né per le Forze armate americane che sono rispettatissime e hanno tutta l'autonomia di cui abbiamo parlato. parlato. L'autonomia delle Forze armate non significa che il potere politico si ritira come nella marea, per cui a un certo punto, se il mare preme di più, le spiagge si ritirano. L'autonomia delle Forze armate significa che il potere politico è il solo che conta perché è eletto: questa è la democrazia; fuori di questa situazione non c'è democrazia.

da dove viene questo pescaggio profondo? Per esempio, a voi che, come me, siete amici della cultura degli Stati Uniti,

Questo libro narra la storia di tutte le menzogne e falsità nate nei Servizi e nei para-Servizi italiani e trasferite, anche se incoscientemente, anche senza che lo sapessero gli interessati, con il giudizio drammatico delle fonti di *intelligence* americane.

che hanno preparato quella che qui viene chiamata «*The italian letter*», che vuol dire prove false di eventi falsi, come quelli che stiamo qui discutendo. Ma perché non vedere due articoli apparsi

Sul «Corriere della Sera» di oggi si legge: «Nell'archivio segreto del Sismi l'agente Pompa conservava anche un nuovo dossier contro l'attuale premier: atti giudiziari di tutte le inchieste contro Prodi, anche se archiviate, e suoi discorsi come presidente della Commissione europea, con annotazioni negative. Vincenzo Visco, il viceministro che ha perso la delega sulla Guardia di Finanza per il caso Speciale, è il primo politico della lista dei 45 nemici

«E, mollate le toghe, dossier e report vanno a frugare tra i movimenti "girotondini" e associazioni antiberlusconiane. Insomma, più che un ufficio del Sismi, quest'ufficio "pollariano" appare come una specie di agenzia di protezione di Silvio Berlusconi». Allora, ho l'onore di dirvi

ora stanno facendo questa *claque* penosa, l'Italia è nelle mani dello spionaggio; se vincono coloro, tra tutti noi, compresi molti di voi,

noi dell'Italia dei Valori, su questa vicenda abbiamo assunto una posizione che riteniamo abbia contribuito a far sviluppare una discussione che sarebbe auspicabile fosse più serena, perché attiene a questioni importanti della vita di un Paese democratico. Vi abbiamo contribuito con la presentazione di un ordine del giorno, che poi abbiamo ritirato qualche giorno fa, perché nel Consiglio dei ministri di venerdì ultimo scorso si è verificato quello che noi dell'Italia dei Valori chiedevamo, ossia il ripristino di un'imparzialità che ci sembrava negata rispetto ad una vicenda che aveva interessato - e, per certi aspetti, turbato - l'opinione pubblica. Vede, signor Ministro, parliamo di una questione risalente a un anno fa, sulla quale probabilmente non si è voluto far luce, pensando che il tempo potesse in qualche modo occultare qualcosa di non chiaro che era accaduto, ma che è bene diventi chiaro, grazie al contributo che ci auguriamo venga da parte del Governo. Parliamo del rapporto che deve intercorrere fra la politica e l'alta dirigenza, in particolare, della Guardia di finanza.

lo sappiamo sia io sia l'opinione pubblica - che, per quanto riguarda avvicendamenti che dovessero interessare Milano o la Lombardia, nessuna menzione vi era in quel piano e, soprattutto, che gli ufficiali che in quella Regione e in quella Provincia operavano, dedicati dedicati in quel momento a particolari indagini di Polizia giudiziaria, avevano ricevuto l'encomio della magistratura per la quale svolgevano la propria attività professionale. Lei comprenderà che, in quel contesto,

Valori, è relativo ai quattro nominativi non inseriti nel piano di trasferimenti deciso a marzo, incluso successivamente - a su sollecitazione politica o istituzionale, che dir si voglia. Tale piano, però, finiva per riguardare quattro ufficiali impegnati in una particolare indagine in corso, che godevano della fiducia della magistratura e che per quel lavoro avevano ricevuto encomi. Questo è il punto in l'Italia dei Valori ha ritenuto di dover ripristinare, a fronte di versioni diverse della vicenda, una situazione di imparzialità che, a suo avviso, deve sempre impregnare la conduzione della pubblica amministrazione.

Quando ci siamo resi conto, come Italia dei Valori, che una situazione che vorremo fosse sempre di imparzialità veniva turbata e affacciata sulla stampa come ipotesi di turbativa dell'esercizio di funzioni esplicate in un modo che aveva portato anche ad un riconoscimento encomiastico,

correttamente rimettesse il mandato nelle mani del titolare, il ministro Padoa-Schioppa. Questo avevamo chiesto perché pensavamo che potesse contribuire a svelenire gli animi e dare chiarezza all'opinione pubblica. Questo è avvenuto venerdì, per cui ci sentiamo di condividere come Gruppo Italia dei Valori il comportamento del Governo con alcune precisazioni, Ministro. In primo luogo, poteva essere fatto molto prima; lasciar marcire le situazioni non produce mai niente di buono, soprattutto in democrazia. In secondo luogo, va chiarito perché un ufficiale e non un dirigente, un tenente colonnello, è oggetto di questa presunta richiesta di trasferimento; situazione avulsa dal trasferimento dei dirigenti. luogo, perché aver atteso tanto e su sollecitazione di tanta parte dell'opinione pubblica, senza rendersi conto che un gesto nobile avrebbe reso più forte chi lo compiva, un gesto nobile che, al termine delle indagini, avrebbe rafforzato chi lo avesse compiuto in tempi non sospetti. Io sono fra quelli che ritengono che cento torti non fanno mai una ragione. Ho letto stamattina su «l'Unità» un interessante articolo di Rossi, in cui sulla vicenda si fa riferimento al fatto che l'ex ministro Tremonti azzerò di colpo i vertici della Guardia di finanza in epoca in cui aveva questa delega. Bene, credo che sia il modo peggiore per giustificare in questa vicenda quel che è avvenuto o non è avvenuto; dire che altri hanno fatto un errore non legittima mai chi oggi opera a compiere lo stesso errore. Credo, quindi, che sostenendo queste tesi, probabilmente non incontriamo il favore di coloro che ci hanno voluto al Governo per cambiare e innovare rispetto a ciò che avveniva prima. Dire che già Tremonti aveva azzerato senza render conto è un tentativo sbagliato di giustificare quel che è avvenuto. Pensiamo invece che questo dibattito sia una cosa sana perché sta avvenendo nei luoghi deputati a ciò, cioè nelle Aule parlamentari, e riteniamo che questo dibattito - se l'epilogo sarà quello che noi dell'Italia dei Valori

preso atto anche della richiesta che veniva dall'Italia dei Valori e si è congelata quella delega. Secondo noi, si sono, quindi, ripristinate le condizioni di imparzialità e si può andare avanti con serenità e fiducia rispetto all'indagine che la magistratura di Roma ha aperto.

quali sono i contorni che hanno determinato il provvedimento che riguarda il comandante Speciale e un punto sul quale, anche qui, non si può far finta che non sia successo nulla. Dico solo una cosa di carattere personale. È una persona che ha sbagliato nelle prime ore del provvedimento, ma poi, ieri, si è comportato come si comporta e si dovrebbe comportare sempre un servitore dello Stato, annunciando che non avrebbe fatto ricorso al TAR, che avrebbe preso atto del provvedimento, al TAR, che avrebbe preso atto del provvedimento, dicendo una frase che da tempo non ascoltavamo: «Obbedisco». Credo che su questo punto sia necessario che il Governo sia quanto più esaustivo possibile.

ci dicesse cosa non ha funzionato nel rapporto di collaborazione tra il Comandante generale della Guardia di finanza e il vice ministro Visco e ci dicesse anche se un Governo ha la potestà di cambiare un alto funzionario dello Stato, in questo caso il Comandante generale della Guardia di finanza, quando viene meno il rapporto di fiducia. In un delicato sistema di pesi e contrappesi per i militari, da un punto di vista regolamentare, le norme di principio sulla disciplina militare, di cui alla legge n. 382 del 1978 e al regolamento di disciplina, prevedono nei doveri attinenti alla dipendenza gerarchica il dovere di obbedienza nei confronti del Ministro competente e dei Sottosegretari di Stato quando esercitano le funzioni loro conferite per delega del Ministro, mentre vi è piena autonomia del Comandante generale e delle Direzioni generali dell'amministrazione per quanto riguarda la movimentazione del personale. Questo impianto definisce il delicato equilibrio tra ruoli, funzioni e poteri finalizzato a consentire il corretto perseguimento dei compiti d'istituto dei Corpi armati dello Stato, militari e non. Io non ho elementi per mettere in dubbio l'onorabilità del generale Speciale, riaffermata dall'«obbedisco» di ieri pomeriggio, né la correttezza istituzionale del vice ministro Visco, poiché a tutt'oggi nessuno degli organi competenti ha rilevato irregolarità nel comportamento del rappresentante del Governo. D'altronde, il sistema delle garanzie previste per tutti i cittadini, tante volte rivendicato giustamente ed evocato anche dai colleghi dell'opposizione, deve valere anche per chi ha ruoli di governo. Ma se l'onestà, innanzitutto intellettuale, non è in discussione, dobbiamo chiederci cosa non ha funzionato. rispondesse al vero che il Vice ministro dell'economia e delle finanze ha rappresentato, nel quadro degli avvicendamenti degli ufficiali della Guardia di finanza, una soluzione allo stato di criticità di Milano, segnalatagli dal vice comandante della Guardia di finanza e da altri alti funzionari del Ministero, si deve dire che era nel pieno diritto di farlo senza ledere le competenze del Comandante generale e le proprie. È successo altre volte che sono stati avvicendati alti funzionari della pubblica amministrazione, quindi, in un contesto di rapporti di fiducia rispettosi e leali, ovvero di normalità, questa vicenda non avrebbe avuto nessun seguito né il clamore mediatico che ha portato a questo dibattito. Evidentemente vi sono ragioni altre per capire ciò che sta succedendo. Liberando la riflessione dalle tante dietrologie avanzate dagli organi di stampa e da quelle ancora rese possibili dalla sterminata fantasia umana, il problema che ci consegna questa vicenda è il rapporto tra potere politico ed altri poteri in cui si articola lo Stato, ovvero la capacità-potestà della guida politica del Paese e del Governo di cambiare un vertice militare riaffermando il primato del potere politico sugli altri poteri. Un primato ed un potere che nella scorsa legislatura sono stati più volte esercitati dall'attuale opposizione nelle stesse identiche forme attuate dall'attuale Governo. Censurare, inibire, come si pretende oggi il primato del potere politico del Governo sul potere dei Corpi armati dello Stato, è mio parere irresponsabile ed avventuroso per i caratteri del nostro impianto democratico. Rendere precaria la certezza di regole e di trasparenza di rapporti genera sfiducia nei confronti di chi decide e sospetto sul beneficiato; si rischia di alimentare la convinzione che per raggiungere determinati obiettivi occorre essere vincolati a parti politiche, cordate, gruppi di potere. Poiché ne ho sempre avuto stima personalmente, in questo contesto

voglio sperare siano da inquadrare le difficoltà del generale Speciale nell'ambito di questa vicenda, ovvero la necessità anche da parte sua di salvaguardare la propria posizione, altrimenti tutto diventa più oscuro. Tra gli errori di valutazione possono catalogarsi le azioni condotte dal Comandante generale della Guardia di finanza nell'ambito dei rapporti con le autorità cui doveva far riferimento. Un militare della sua esperienza conosce bene le regole della gerarchia. Se si sentiva vittima di ingerenze, di pressioni o di decisioni non condivise con il Vice ministro, perché non si è rivolto al titolare del Dicastero, cioè alla sua persona? Perché fatti di un anno fa vengono alla luce oggi, in un contesto scandalistico ed eclatante ad uso di una parte politica? La legittimità del Governo a sostituire un alto funzionario dello Stato non può essere messa in discussione in discussione senza che si abbia coscienza delle conseguenze di siffatta scelta. Sono convinto che non è utile neanche all'opposizione strumentalizzare la vicenda al fine di mettere in difficoltà il Governo attuale, ipotecando con un pessimo precedente le facoltà dei Governi successivi. In realtà, mi sembra che la lucidità dell'opposizione sia offuscata dall'uso strumentale di ogni soffio di vento dall'inizio della legislatura in poi per cercare di dare la spallata al Governo. Eppure questioni di tale delicatezza, soprattutto quando riguardano le Forze armate e i Corpi armati dello Stato, devono essere affrontate responsabilmente, con grande senso dello Stato e soprattutto con grande equilibrio. I vertici delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato devono restare fuori dalle competizioni politiche. Non per niente nell'unico grande dibattito avvenuto dal dopoguerra ad oggi sulle Forze armate e i loro compiti, che ha prodotto le norme di principio della disciplina militare, cioè la legge n. 382 del 1978, fu sancito che le Forze armate debbano mantenersi fuori dalle competizioni politiche e che ai militari che si qualificano come tali o che indossano l'uniforme sia vietato partecipare a manifestazioni di partito o di organizzazioni politiche. Bisogna proteggere le Forze armate, recuperando quello spirito che consentì di varare una legge condivisa da tutti, che diede luogo al processo riformatore che ha variato i criteri della disciplina militare, trasformando la concezione dell'obbedienza da assoluta in partecipazione consapevole nei vincoli di subordinazione, facendo sì che l'obbedienza diventasse pronta, rispettosa e leale, che ha prodotto le rappresentanze militari e ha portato il mondo militare a più stretto contatto con le istituzioni locali, aprendosi alla società civile. Ecco, istituzioni militari aperte, leali chiare nel loro rapporto con la comunità nazionale e con il Governo, che la comunità nazionale ha insediato a presidio della democrazia e a gestione della cosa pubblica. È con questo spirito, signor Ministro e cari colleghi, che concludo rinnovando piena fiducia nell'operato del Governo e la nostra più totale considerazione della Guardia di finanza per il difficile e delicato compito che svolge, esprimendo soddisfazione per i risultati raggiunti soprattutto nella lotta all'evasione fiscale.

colleghi, molto improvvidamente per la sua parte politica il collega Furio Colombo ha messo in rilievo la caratteristica fondante del dibattito che stiamo facendo oggi, dibattito basato sull'informazione giornalistica mediatica. È vero, collega Colombo, ma per una motivazione altrettanto vera, perché il Governo si è rifiutato di illustrare la sua posizione formale dai Gruppi AN, FI e LNP).* Quindi, stiamo discutendo di ciò che appare sui giornali, perché il suo Governo, collega Colombo, si è rifiutato di venire in Aula all'inizio del dibattito a dire cosa era successo e cosa ne pensava. Io, a differenza di lei, credo che nella TV di Stato sia rimasta un'unica trasmissione non faziosa, quella che lei ha citato, «Porta a porta», e credo che il dottor Bruno Vespa sia un professionista di valore, ma se fosse vero quello che lei dice, collega Colombo, vorrebbe dire che sta seguendo le orme di un suo maestro, e cioè del suo carissimo amico Santoro. Escludo che Vespa voglia diventare come Santoro. Ciò detto come premessa, vorrei limitarmi a due aspetti, sempre sulla base delle informazioni giornalistiche che abbiamo a disposizione, e quindi rivolgere al rappresentante del Governo delle domande. I due aspetti sono: chi sono i soggetti in gioco e quali sono gli oggetti in gioco e in discussione, perché a me non è chiaro. Abbiamo già visto questa mattina, circa i soggetti in gioco, che molto probabilmente, allo stato delle nostre conoscenze oggi pomeriggio, il Paese sta vivendo una situazione surreale nella quale esistono due comandanti generali della Guardia di finanza: uno non revocato e uno nominato per decreto. Ma vorrei capire anche qual è il soggetto, nell'ambito del Governo, che ha la delega sulla Guardia di finanza. Essendo stato io Vice ministro dell'economia, ricordo che, a differenza del Sottosegretario, il Vice ministro dell'economia riceve le deleghe su proposta del Ministro competente, ma le riceve direttamente dal Presidente del Consiglio e dal Consiglio dei ministri. Nel momento in cui un Vice ministro, seppur temporaneamente, rimette le deleghe, evidentemente le rimette a chi gliele ha date, cioè al Presidente del Consiglio e al Consiglio dei ministri. Esiste, in data venerdì 1° giugno, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che affida la delega sulla Guardia di finanza al Ministro dell'economia e delle finanze? E poiché il collega Calderoli stamattina ha sollecitato il Presidente del Senato ad avere a disposizione il verbale del Consiglio dei ministri, io aggiungerei anche la seguente ulteriore il Ministro dell'economia e delle finanze, che siede in quest'Aula, quando e attraverso quale atto ha ricevuto la delega sulla Guardia di finanza?

che un Vice ministro riceve la delega sulla Guardia di finanza: è come se il Ministro dell'interno non avesse la delega sulla Polizia e questa fosse affidata ad un Vice ministro.

per ottenere la delega sulla Guardia di finanza. Quale era allora la motivazione, visto che in quel momento era un atto assolutamente straordinario nella storia della Repubblica italiana? Perché un Vice ministro delle finanze chiede lui stesso, direttamente, per sé, la delega sulla Guardia di finanza? Forse, sempre leggendo i giornali che si sono succeduti, riusciamo a capire perché ha preteso quella delega come fatto straordinario. E allora si capisce l'oggetto. Cari colleghi, l'oggetto è surreale, è inutile che ci nascondiamo dietro a un dito. a un dito. L'attuale Governo ci ha abituato, in quest'Aula, a discutere di tematiche surreali, faccio un unico riferimento, che è, come diceva Manzoni, passato ma non trascorso: questo è un Governo che ha occultato il gettito del 2007 a dicembre e a marzo ha scoperto un tesoretto. È un dibattito surreale.

perché il tentativo di sminuire il ruolo dell'uomo Speciale, palesemente in atto sulla stampa della vostra parte, collega Furio Colombo, significa dimenticare - forse il ministro della difesa Parisi lo ricordava quando ha fatto presente alla sua maggioranza che il caso Visco non si sarebbe chiuso così, senza che nulla fosse - che prima di essere comandante generale della Guardia di finanza, sostenuto proprio in questi giorni dal COCER dei Carabinieri (tanto per dare il clima interno alle varie forze dell'ordine), ha collaborato per anni con un predecessore del ministro Parisi: colui che ha impostato tutta la riforma del sistema di difesa del nostro Paese con il passaggio dal servizio di leva obbligatorio al volontariato. Mi riferisco al ministro Andreatta. Allora, certi comportamenti lo uccidono due volte, non fisicamente, ma in quello che resta, in quella lezione di senso civico, di senso delle istituzioni che questo Governo dimentica il giorno e soprattutto la notte, perché i vertici per mettersi d'accordo sono fatti, come si dice al mio Paese, come i ladri di Pesaro,

cari colleghi, il dibattito che stiamo svolgendo non è sul caso Visco-Speciale, ma su un fatto molto più profondo che non è affatto surreale, ma reale: nella vostra maggioranza si sono formati due comitati di controllo, due patti di sindacato l'un contro l'altro armati che giocano sul sistema bancario, finanziario, industriale e produttivo e ciascuno ha le proprie leve al di fuori di questo Paese. Questo è il tema che stiamo affrontando. Non la questione quasi personalistica tra il generale Speciale e il vice ministro Visco. I due patti di sindacato si scontrano sul serio sin dal primo giorno,

che una parte della vostra maggioranza agì per impedire l'operazione UNIPOL-BNL per poi consentire altre operazioni di aggregazioni bancarie; l'altro patto di sindacato con un'altra aggregazione bancaria. Non prendiamoci in giro: questo è lo scontro di potere in atto all'interno del centro‑sinistra. Chiudo con un'ultima domanda

testimoniando rapporti incestuosi all'interno dei due patti di sindacato tra fratelli e cugini? Sottolineo la parola fratelli, e voi sapete cosa intendo. *(Applausi dai

ho ascoltato molti colleghi esprimere solidarietà alla Guardia di finanza; credo che sia giusto farlo per il compito importante e molto delicato svolto quotidianamente nel perseguimento dell'evasione fiscale. Infatti, sappiamo che solo attraverso l'imposizione fiscale

Con i cittadini militari non possiamo limitarci ai ringraziamenti; dobbiamo prendere atto che c'è bisogno per loro di riforme. Ci sono sofferenze - le sentiamo in questi giorni, esprimono anche questo - tensioni, bisogni individuali e collettivi che non riescono a trovare espressione. Il punto è che, specialmente adesso che abbiamo abolito la leva obbligatoria, organismi con competenze così ampie e importanti per il Paese non hanno dei presìdi di controllo democratico interno con poteri reali. Devono esserci delle strutture che svolgono funzioni così rilevanti che oggi invece non esistono e non hanno reali contrappesi di controllo democratico. Questo è un problema vero e gli attuali organismi della rappresentanza militare - parlo dei COBAR, dei COIR e dei COCER -, come moltissimi delegati denunciano da anni nei siti, nei *blog* e nelle loro corrispondenze, non sono sufficientemente in grado di assicurare funzioni di questo tipo. C'è una frustrazione e un disagio che spetta alla politica rilevare e risolvere. È un problema che noi non possiamo più rinviare. Al Senato la Commissione difesa sta discutendo la riforma della vecchia legge del 1978, che si trascina da tre legislature,

nulla. Voglio dire che c'è bisogno di una riforma della rappresentanza militare; i soggetti che sono chiamati per primi a difendere la democrazia non devono rimanere esclusi dalle regole della democrazia I militari devono vivere e respirare democrazia nei loro organi di rappresentanza e nelle associazioni che anche loro, come prevede la Costituzione, devono poter costituire. Sto parlando del tema della rappresentanza che però è anche il tema della sindacalizzazione, portato avanti con coraggio e determinazione da diversi COCER, tra cui quello della Guardia di finanza è da tempo in prima linea. Questa richiesta di sindacato, vista con sospetto in molti ambienti, nonostante sia presente in diversi Paesi europei - lo voglio dire; noi diciamo di essere un Paese europeo ma in questo campo rimaniamo molto indietro

non ci sono i soldi per le indagini fiscali, per l'utilizzo dei mezzi dei servizio, per la benzina (parliamo di condizioni che conosciamo tutti). Questa situazione ci porta al dibattito svolto durante l'ultima finanziaria, in cui per il comparto difesa si sono raddoppiate le risorse per gli investimenti in armamenti a scapito delle spese per l'esercizio, quali l'addestramento e la manutenzione che sono così importanti perché significano condizioni di sicurezza del personale.

*(LNP)*. Signor Presidente, colleghi, sulla vicenda che ha visto e vede protagonista il vice ministro Visco il Governo ha scritto una pagina vergognosa della sua breve, e mi auguro non ancora lunga, vita e storia. L'Italia, dopo la traumatica rimozione del Comandante della Guardia di finanza (effettuata peraltro senza nemmeno una chiara motivazione), si è trovata davanti ad una scelta: se credere ad un ufficiale che ha sempre servito fedelmente il suo Paese, dando anche in queste ore prova di grandissima dignità (non come invece altri hanno fatto e fanno), oppure credere ad un esponente del Governo. Mi pare che la gente, i cittadini i cittadini (non gli esponenti interessati di questa maggioranza scollata e avventurista) abbiano deciso e che questa scelta sia caduta sul generale Speciale, che è uscito a testa alta, non cedendo alle lusinghe di un incarico alla Corte dei conti, che peraltro non aveva chiesto e che poteva senz'altro essere un ragguardevole viatico dopo l'umiliazione subita. Quando il mio partito, il mio movimento, la Lega, insieme a tutta la Casa delle Libertà (anche se, comunque, giustamente con sfumature diverse), ha chiesto a Visco di farsi da parte, lo ha fatto perché in questo gesto ha visto l'unico modo per ridare al Paese, alla Nazione, la fiducia nel Governo, che altrimenti non ci sarebbe più stata. E invece l'Esecutivo, e con esso la coalizione di maggioranza, ha deciso di andare avanti lungo la miope strada della difesa, contro tutto e tutti, di un suo rappresentante che ha violato il primo e più importante comandamento che è chiamato a rispettare chi entra a far parte del Governo: agire per il bene comune e non solo di una parte o addirittura per se stessi. Qui, colleghi, non si è trattato di un benevolo consiglio dato dal politico a chi con lui ha relazioni di lavoro: qui si è trattato della richiesta di maggiore attenzione nel valutare qualcosa e non si è trattato della richiesta di ancora più profondo rigore nel perseguire chi eventualmente ha violato la legge. Qui, colleghi della maggioranza, si è trattato dell'incredibile richiesta ultimativa fatta da un esponente del Governo di decapitare i vertici territoriali della Lombardia della Guardia di finanza per fini che non si capisce quali siano e che comunque sono senz'altro poco chiari. Appare ancora più strana un'altra cosa. Gli organi di stampa e i media, che negli ultimi giorni hanno dato tanto spazio a questo argomento, non hanno attribuito, a mio avviso, il giusto rilievo al fatto - conosciuto da tutti - che il generale Speciale, venuto a conoscenza dei contatti avvenuti fra il vice ministro Visco e il comandante in seconda, generale Pappa, e il comandante dei reparti di istruzione (vale a dire praticamente il numero tre della Guardia di finanza), generale Favara,

che ben si sono guardati dal darne notizia all'unico titolato a mantenere i rapporti con l'autorità politica, cioè il comandante Speciale stesso. Ora la maggioranza fa quadrato intorno a Visco cerca di trovare il modo di giustificare il suo comportamento davanti al Parlamento e pertanto innanzi all'opinione pubblica. Ma come si può trovare una giustificazione come si po' pensare che l'Italia possa credere che quanto ha fatto Visco rientri nelle normali competenze di un Vice ministro? Se tale comportamento fosse stato messo in essere da parte della coalizione di centro-destra, si sarebbe ricorso ad una sollevazione popolare. Eppure, il tentativo abbastanza, anche troppo palese è il seguente: allargare i confini della vicenda, quindi renderli meno chiari, indefiniti, per poi alla fine, magari, sperare che il tempo renda meno obbrobriosa questa storia. Alcuni esponenti della sinistra paventano l'ipotesi che si sia voluto colpire il vice ministro Visco perché è l'uomo che ha iniziato una battaglia contro l'evasione fiscale, ma non si sono accorti che lo stesso vice ministro Visco ha posto in essere un'altra battaglia, contro la Guardia di finanza. Viene a questo punto spontaneo

maggiormente responsabile, il vice ministro Visco, attingendo alla sua dignità, avrebbe dovuto avere il coraggio e la responsabilità di andarsene, magari per potersi poi meglio difendere da un'accusa, che è essenzialmente politica e morale, ma non per questo

e tanto meno della sua onorabilità, né dell'indipendenza e dell'autonomia dei Corpi armati dello Stato. La Guardia di finanza - come hanno detto altri - ha dato un contributo fondamentale alla lotta all'evasione fiscale i suoi uomini sono fedeli alla Costituzione e professionalmente preparati; ma alcuni dei suoi uomini, anche nel recente passato, non si sono dimostrati degni di questa tradizione: oggi si parla di uno di questi. I fatti di cui stiamo discutendo si sono verificati nel mese di luglio 2006, quasi un anno fa: dopo una discussione sugli assetti interni e su sollecitazione di due generali della Guardia di finanza, tra il vice ministro Visco e il generale Speciale si arriva ad un'intesa sugli avvicendamenti di un gruppo di ufficiali e il 14 luglio il generale Speciale scrive a Visco allegando un elenco di quattro ufficiali della Guardia di finanza in Lombardia che devono essere trasferiti, quelli - per intenderci - di cui Visco avrebbe sollecitato l'allontanamento. Il 17 luglio mattina - tre giorni dopo l'avvocato generale dello Stato presso la procura della Repubblica di Milano, Manuela Romei Pasetti, convoca per le ore 15 del medesimo giorno Speciale e Spaziante per chiarimenti su quella nota: iniziativa fulminea, con tempi di esecuzione tali che lasciano pensare che i generali fossero già pronti dietro la porta. Manuela Romei Pasetti è una toga di un colore simile a quello del cielo, non è difficile pensare che tutto questo sia stato combinato in vista di una sua utilizzazione politica. Si cominciano a configurare i contorni della trappola in cui è destinato a cadere il vice ministro Visco: gli ufficiali elencati non vengono trasferiti, una consultazione interna promossa da Speciale fa emergere un parere negativo. Questi ufficiali sono l'ultima generazione di ufficiali della Guardia di finanza lombarda affermatasi dopo la normalizzazione della Lombardia promossa e realizzata dal ministro Tremonti. Già dal 2001 il Ministro si era ripromesso di occupare la Guardia di finanza lombarda con i suoi uomini fidati, sostituendo quelli che avevano dato tanto fastidio a Mediaset con investigazioni e perquisizioni troppo invasive. Il generale Mosca Moschini, peraltro, non è più al vertice della Guardia di finanza. Il primo passo di Tremonti è la sostituzione del generale Giovanni Maiella, che Mosca Moschini aveva chiamato a sostituire nientemeno che - attenzione - Nicolò Pollari. Maiella è un ufficiale brillante ed integerrimo, responsabile dell'*intelligence* della Guardia di finanza. Nessuno protestò. Nessuna procura chiese il conto di questa destituzione. Ma Tremonti fa di più, modifica la struttura e la dipendenza gerarchica del cosiddetto II reparto, punto di collegamento e di scambio con il SISMI e che Maiella aveva comandato. Le informazioni raccolte non sono più trasferite al Comando generale ma si fermano ai Comandi regionali. Questi diventano i veri centri di potere della Guardia di finanza. L'anno seguente viene sostituita l'intera catena di comando della Guardia di finanza in Lombardia. Nessuno ha sollevato proteste su questo, neanche, a dir la verità, nell'ambito dell'allora opposizione. Il comando interregionale viene affidato a Emilio Spaziante, uomo di Pollari e insediato in un luogo che è l'epicentro dei nuovi poteri economici e politici affermatisi dopo le elezioni del 2001. Il comandante provinciale è Rosario Russo e al Nucleo regionale di polizia tributaria viene assegnato il colonnello Stefano Grassi, collaboratore diretto del ministro Tremonti al Ministero dell'economia. L'occupazione della Guardia di finanza lombarda da parte di Tremonti procede anche negli anni successivi, con il fervido supporto del generale Speciale che nel suo fervore usa procedure non conformi alle regole, non esegue valutazioni attendibili delle persone chiamate agli incarichi, distribuisce encomi, che nella Guardia di finanza significa agevolare le promozioni, e solleva le perplessità di due alti ufficiali della Guardia di finanza che ne riferiscono a Visco. Di qui la richiesta a Speciale degli avvicendamenti. Ma Visco non ha compreso quale sia il grumo di potere opaco con cui ha deciso di confrontarsi: quello della rete delle intercettazioni abusive,

ma siamo di fronte alla manifestazione di un intreccio tra politica e aree deviate degli apparati segreti dello Stato. D'altra parte, cosa sono state le operazioni Mitrokhin, la violazione della *privacy* fiscale di Prodi, il dossieraggio accumulato con le intercettazioni clandestine, gli assalti informatici? Qui c'è qualcuno che sa bene queste cose. VALENTINO *(AN)*. Torniamo ai fatti. Perché il generale Speciale non comunica al Ministro le perplessità della procura? Perchési fa interprete attento di quelle preoccupazioni e denuncia a loro salvaguardia le pressioni del Ministro, mentre in altre circostanze questo è il punto - di fronte ad analoghe preoccupazioni di altre procure, non se ne è dato assolutamente per inteso? Voglio riferirmi alla sostituzione dell'ufficiale

alla quale Speciale non prestò minimamente orecchio. C'è poi il caso della rimozione di Castore Palmerini dal Nucleo di tutela del mercato, che che indagava, relativamente ad un problema di carceri, su Giuseppe Magni, braccio destro dell'allora ministro Castelli, e che si interessava, guarda caso, anche ad una parte del conflitto di interessi della famiglia Berlusconi: in due giorni fu spostato ad un oscuro incarico, nonostante fosse un ottimo ufficiale e vi fosse e vi fosse una presa di posizione di magistrati contro il trasferimento. Allora, è una fortuna

È stata una fortuna che costui abbia rinunciato ad accedere alla Corte dei conti perché avremmo messo la volpe a guardia del pollaio! questa proposta di sistemazione non è stata attentamente considerata ed è un gesto debole cui il Governo è stato indotto, come avete sentito anche negli interventi che mi hanno preceduto, da divisioni interne alla stessa Unione.

Innanzitutto, la Guardia di finanza non c'entra assolutamente in questa vicenda; la Guardia di finanza merita tutto il nostro rispetto per la professionalità e per l'impegno che mette nel proprio lavoro.

È stato affermato che con la revoca del generale Speciale è stato commesso un atto di eversione, è stata commessa una violazione della Costituzione: niente di più falso!

che stabilisce come viene nominato il Comandante della Guardia di finanza. Viene nominato con un atto squisitamente politico non viene nominato dal Capo di Stato maggiore della Difesa o dell'Esercito. È un generale di Corpo d'armata dell'Esercito,

difesa, tra gli ufficiali di Corpo d'armata dell'Esercito non per le sue capacità, ma per la fiducia che questi due Ministri ripongono in quell'ufficiale. Viene poi designato dal Consiglio dei ministri e, quindi, a norma dell'articolo 87 della Costituzione, è nominato con decreto presidenziale.

Questa è la sacrosanta verità. Vediamo dunque quali sono le ragioni che hanno indotto la Presidenza del Consiglio dei ministri a revocare tale incarico.

dai giornali, in particolare dal vostro giornale che ha pubblicato questa vicenda. Una prima volta l'ANSA pubblicò che c'era stato questo trasferimento per bloccare le indagini.

gli ha presentato un elenco di ufficiali da trasferire, i cosiddetti movimenti, e allora il Vice ministro ha che non c'erano gli ufficiali di Milano. Badate che questi movimenti sono assolutamente normali, perché è un principio di buona amministrazione non lasciare molti anni negli stessi posti gli stessi ufficiali,

che si volevano decapitare i vertici di Milano per determinate ragioni, cioè - dicendolo proprio chiaramente - per bloccare le indagini della Guardia di finanza in quella città. Ebbene, è stata dimenticata un'altra cosa da parte di tutti.

perché, per fortuna, il nostro codice del 1988 ha rimediato a una situazione del genere, garantendo che le indagini della magistratura andassero sempre avanti.

le sezioni di polizia giudiziaria. Inoltre, nelle disposizioni di attuazione, all'articolo 14, si è detto chiaramente che i dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria per essere trasferiti dall'Amministrazione devono ottenere il consenso del procuratore della Repubblica e del procuratore generale. Pertanto, non poteva assolutamente succedere che si adottasse un provvedimento del genere per impedire la prosecuzione delle indagini. Non si poteva fare, perché, se lo avessero fatto senza chiedere il consenso della magistratura, avrebbero commesso un reato. Che questo sia ben chiaro: è stato il legislatore del 1989 a dare questa garanzia per l'indipendenza della magistratura e della stessa polizia giudiziaria. Senza contare poi che queste indagini non erano affidate esclusivamente a quei servizi, ma anche alla polizia giudiziaria, che aveva un comandante che conosco personalmente, il colonnello Martino, un uomo di grandi capacità, e quindi non sarebbero state fermate; inoltre, erano condotte anche dal nucleo di polizia valutaria di Milano e di Roma. Quindi, questa è una grossa falsità. falsità. Veniamo al comportamento dell'ufficiale, che deve avere la fiducia del Ministro delle finanze; deve averla perché deve seguire il suo indirizzo politico per fare da tramite con il corpo della Guardia di finanza.

E allora, ecco l'allarme; ecco che si spiega anche l'intervento del procuratore generale, perché si tratta dell'allarme che dà un comandante generale infedele con il Ministro.

quanto stava accadendo a Milano, chiedevano in qualche modo l'attenzione del Governo. Peccato che a quell'interrogazione del 18 luglio 2006 non sia stata data alcuna risposta: ciò avrebbe evitato tanti problemi di cui oggi stiamo parlando. Onorevole Presidente, cari colleghi senatori, onorevole Ministro, il senatore Andreotti, sulla vicenda Visco-Speciale, ha parlato di un clima di squallore. Sono ancora più pessimista, colleghi

sulla vicenda Visco-Speciale, ha parlato di un clima di squallore. Sono ancora più pessimista, colleghi senatori: ho molta preoccupazione. Stiamo vivendo momenti bui della democrazia del nostro Paese. FI).* Questa è la realtà, cari colleghi, perché la vicenda di cui stiamo discutendo nasce da un abuso d'ufficio politico del Governo Prodi e da un arrogante atto di ingerenza, in materia attribuita in via esclusiva alla competenza del comandante generale della Guardia di finanza (alla luce dell'articolo 4 della legge n. 189 del 1959, citata dal senatore D'Ambrosio)

La nostra Costituzione, cari colleghi e soprattutto caro senatore D'Ambrosio, con apposite norme ha delineato lo svolgimento dei rapporti fra Capo dello Stato e Governo e tra Governo e pubblica amministrazione, rapporti in ogni caso da svolgersi nel rispetto del principio di legalità, sottolineo nostra - di democratici dello Stato di diritto. In tale quadro è chiaro e indiscusso il dato per cui non possono essere ammesse potestà dei pubblici poteri, nemmeno politiche, il cui esercizio sia sottratto all'osservanza del principio di legalità. Quando il presidente emerito della Repubblica, senatore Cossiga, afferma che, in caso di contrasto tra politica e amministrazione militare, prevale il parametro politico coglie solo in parte la verità, perché tale prevalenza non può dar luogo ad atti concreti o comportamenti che contraddicano il principio di legalità. Nel caso Visco-Speciale, infatti, ci troviamo di fronte ad un atto o più atti del Consiglio dei ministri (revoca, nomina, avvio di procedura per incarichi esterni all'ordinamento militare) che, essendo illegittimi, non hanno la forza costitutiva dell'effetto giuridico (rimozione del generale Speciale) in funzione del quale gli atti stessi sono stati assunti.

Quindi, non c'è potere politico che in qualche modo possa interferire con poteri assegnati da apposita legge al comandante della Guardia di finanza. Le interferenze esercitate e comprovate dal vice ministro Visco sono, dunque, illegittime sul piano giuridico, ma anche sul piano più strettamente politico per le seguenti considerazioni che mi permetto di fare. Non vi è dubbio che il rapporto tra il Governo e l'amministrazione della Guardia di finanza rientra nella limitata categoria dei cosiddetti atti di alta amministrazione riguardando l'assetto e l'organizzazione dell'ordinamento della sicurezza del nostro Paese, tanto è vero che le decisioni in materia non sono assunte dal Ministro, ma richiedono il consenso dell'intero collegio ministeriale; assumono, pertanto, immediata rilevanza politica (lo voglio ricordare in particolare alla senatrice Finocchiaro) e si può asserire che tali atti costituiscono un parametro di raccordo tra politica e amministrazione che esigono correttezza politica e trasparenza giuridica. Nel caso del comportamento del vice ministro Visco ciò non è avvenuto e non possiamo ridurre l'episodio ad un fatto di mera promozione o mera e normale rimozione a liquidare il tutto al rango di un problema marginale. Il Consiglio dei ministri (dalle scarse e reticenti dichiarazioni che abbiamo letto tutti sui giornali) fa comprendere che si è trattato di un mero avvicendamento al posto di comandante generale della Guardia di finanza. Va precisato che ci sono due tipi di avvicendamento, lo sanno tutti, immagino anche il senatore D'Ambrosio: quello quello ordinario per raggiunti limiti di età o dimissioni dell'interessato e l'altro forzato se si dà luogo a rimozione della carica in assenza delle condizioni citate. La decisione di sostituire il generale Speciale rientra nella seconda ipotesi e, quindi, il Governo ha assunto un atto di sostituzione con altra persona in maniera illegittima perché il posto di comandante generale della Guardia di finanza, per le questioni che hanno detto i colleghi questa mattina e oggi pomeriggio, non è nella disponibilità del Governo, al momento, in quanto il mero avvio della proposta di nomina del generale Speciale a consigliere della Corte dei conti non è sufficiente a trasformare da forzoso a normale l'avvicendamento del generale Speciale che, peraltro, ha ripetutamente negato - anche oggi - il suo assenso alla proposta di essere nominato consigliere alla Corte dei conti. Ed allora, in presenza di un avvicendamento forzoso - aggiungo, solo per motivi politici - scatta l'obbligo, senatore D'Ambrosio, per il Governo di osservare le regole del procedimento sanzionatorio disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 (cosiddetto giusto procedimento), che prevede una serie di garanzie per i funzionari dello Stato contro cui il Governo ponga in essere atti di restrizione della sfera giuridica del destinatario, come nel caso del generale Speciale. Non è dunque sufficiente quello che lei ricordava, senatore D'Ambrosio, la mera perdita di fiducia da parte del Governo, come sostiene qualche Ministro e come è stato sostenuto da lei: la fiducia del Governo non c'entra in queste cose perché ci sono precise disposizioni a garanzia anche delle cariche dello Stato e di chi è a capo di corpi militari, come quello della Guardia di finanza. Da tale punto di vista, gli atti di nomina e di avvicendamento assunti dal Consiglio dei ministri sono illegittimi e contraddittori. Le ragioni sottese alla rimozione (parliamo chiaro: di questo si tratta e non di normale avvicendamento) del generale Speciale, inoltre, non possono giustificare la contestuale e riparatoria assunzione del provvedimento di nomina dello stesso alla Corte dei conti, a fronte della gravita delle accuse fatte dal Governo al generale Speciale

Voglio, infine, concludere con alcune osservazioni circa il rapporto tra Capo dello Stato, Governo e pubblica amministrazione. So, Presidente, che è un fatto delicato, però voglio parlarne lo stesso. Con tutto il rispetto, sincero e convinto, verso le prerogative del Capo dello Stato, ma spinto dalla lealtà che un parlamentare deve avere nei confronti delle supreme istituzioni, devo precisare il mio punto di vista sugli accennati rapporti istituzionali, ricordando anche il pensiero di illustri giuristi e costituzionalisti che sono stati senatori in quest'Aula (parlo soprattutto del senatore Aldo Sandulli). Nella nostra Costituzione il Governo non può essere considerato Governo del Capo dello Stato, ma è altresì vero che il Presidente della Repubblica, per gli atti per cui obbligatoriamente partecipa all'assunzione (parlo in particolare della nomina di alti funzionari, come nel caso previsto dall'articolo 87 della Costituzione), deve essere ritenuto un partecipe non solo nella forma ma anche nella sostanza. Infatti, il risultato giuridico dell'atto di nomina o di revoca di un comandante generale della Guardia di finanza può essere raggiunto con l'intervento (firma) del Capo dello Stato. Tale intervento, a mio modesto giudizio, non può ridursi ad una forma simbolica e dovuta; al contrario, la partecipazione presidenziale all'azione del potere esecutivo rappresenta l'estrinsecazione di una concreta e reale potestà per l'esercizio della quale è essenziale una coscienziosa valutazione degli effetti politico-istituzionali nel nostro Paese. In definitiva, nel caso Visco-Speciale, il Capo dello Stato avrebbe potuto (non dico dovuto) usare la prudenza derivante dall'articolo 87 della Costituzione che lo definisce come Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale. Non ci aspettavamo dal Capo dello Stato sicuramente il rifiuto della propria firma, ma solo un'azione di persuasione preventiva che evitasse la spaccatura del Paese a fronte della pericolosa situazione che sta sotto gli occhi di tutti quanti noi. Peccato, devo dire. Il Presidente della Repubblica ci aveva abituato a «intromissioni» che avevano fatto rinascere speranze ed aspettative per un Paese migliore. Speriamo che il Presidente della Repubblica, Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale, possa riprendere questo cammino per il bene dell'Italia.

è la rappresentazione di un vero e proprio colpo di mano, di un golpe che scuote e offende la coscienza degli italiani, che continuano a chiedersi e a chiederci: chi difende la democrazia?; continuano a chiederci: che torto ha avuto il generale Speciale? La risposta è semplice: ha avuto il torto di rispondere al pubblico ministero, raccontando la verità. Il comandante generale della Guardia di finanza - è paradossale - è stato rimosso perché ha agito nel rispetto della legge. La sinistra dice che non ci sono state interferenze: ma se non ci sono state (che ci sono state: abbiamo letto i verbali su «il Giornale»), se non c'è stato niente di anomalo, perché allora Visco ha rimesso la delega,

Il perché è chiarissimo: quella «rara tempra di galantuomo» di Vincenzo Visco (così l'ha definito lei, signor Ministro), un anno fa ha minacciato il comandante generale della Guardia di finanza, affinché rimuovesse alcuni ufficiali delle Fiamme gialle sgraditi a lui e al suo partito. E perché? Perché «colpevoli» di aver indagato sul caso UNIPOL, facendo venire alla luce intrecci inquietanti tra la sinistra affaristica e il mondo economico-bancario. E nemmeno ora che Visco è stato travolto dallo scandalo e dalle menzogne, Prodi ha ritenuto che fosse arrivato il momento di dirigersi al Quirinale per rassegnare le dimissioni. E dal Colle, in questi giorni, è arrivato un silenzio francamente imbarazzante: quella a cui abbiamo assistito non è una «baruffa politica», una vera e propria emergenza istituzionale e riteniamo che il Capo dello Stato farebbe bene ad intervenire come garante della Costituzione che all'articolo 97 stabilisce che debba essere assicurata l'imparzialità dell'amministrazione e, quindi, la non interferenza fra i poteri dello Stato. Ora la parola è al Senato e qui non è in gioco solo il Governo, non è in gioco solo l'onorabilità del generale Speciale e di tutta la Guardia di finanza. Ed è davvero stucchevole il comportamento ambiguo dell'Ulivo che, per salvare la poltrona, del giorno loda l'operato della Guardia di finanza (ed è giusto che sia così), ma esclude dall'elogio il generale Speciale. La posta è più alta, qui e in gioco la cultura della legalità. Quella cultura della legalità che questo Governo rifiuta, avendo scelto la strada dell'arroganza e della menzogna. Su questa strada ha, come compagni di viaggio, giornali faziosi e schierati, sempre pronti a disegnare scenari misteriosi. Siamo arrivati perfino a parlare di P2 e di servizi segreti; mancano Star Trek e magari la Banda Bassotti che, per conto di Berlusconi, ruba documenti preziosi. Siamo alla fantapolitica per cercare di mischiare le carte, per nascondere agli italiani la realtà delle cose, ma gli italiani hanno capito bene e sono indignati; hanno capito bene che sono governati da un *Premier* bugiardo ed è per questo che lo hanno già ampiamente sfiduciato. La crisi, che si vuole artatamente addebitare alla politica in generale, cercando in questo modo di coinvolgere tutti in unico calderone, è in realtà la crisi di questo Governo, debole con debole con i forti e forte con i deboli, come testimoniano le buste paga dei salari più bassi e dei pensionati. Oggi, però, abbiamo la possibilità straordinaria di dire basta a tutto questo, abbiamo la possibilità di mandare a casa il Governo delle tasse e il Governo degli imbrogli. Non perdiamo, per favore, questa grande occasione.

al di là di aver sentito un'Aula che più che un Parlamento sembrerebbe poco più che uno stadio, dove ormai si tifa o Guardia di finanza o ministro Visco,

Pirandello. Se oggi chiedessimo ad un italiano quanti sono i comandanti generali della Guardia di finanza, questo non potrebbe che ricordare Pirandello: uno, forse nessuno, forse più di uno, centomila.

Questo Governo, prima, e il Ministro dell'economia, dopo, chissà per quale motivo, hanno infilato una serie di provvedimenti con una velocità inconcepibile, di corsa, sbagliandoli dall'inizio alla fine; ci si chiede per quale motivo. Un italiano non giurista (abbiamo sentito fare grandi lezioni in quest'Aula), di fronte al fatto che qualcuno ingerisca ed attribuisca ad un ufficiale di Guardia di finanza di avere debordato nelle indagini, un normale cittadino dice: «Secondo me, le indagini di polizia giudiziaria spettano ai magistrati, che si avvalgono degli uffici di polizia giudiziaria, quindi anche della Guardia di finanza». Al punto che, avesse avuto un briciolo di prudenza, il vice ministro Visco avrebbe dovuto fare una verifica e annotare che addirittura un procuratore di Milano aveva scritto una lettera di elogio a uno di quegli ufficiali per come stava svolgendo quelle quelle indagini. E via via con i bottoni sbagliati, si parte con il primo e si va avanti così. Ma, ministro Padoa-Schioppa (vale per lei come per il suo vice Visco), disponete di uffici, del Consiglio di Stato che vi può dare degli autorevolissimi pareri, avrete probabilmente degli esimi giuristi che lavorano per voi: com'è che avete portato avanti una questione da emeriti dilettanti? È quasi inconcepibile. Indagini nelle quali si ingerisce nelle inchieste, si rimuovono ufficiali senza motivazioni, si dà esecuzione a provvedimenti prima ancora che diventino esecutivi: ma è tutto un caso? Sono diventati degli sprovveduti tutto d'un colpo? È difficile anche da credere, questo. È casuale? Lo abbino ad un altro evento che non può essere casuale: due giorni fa il presidente del Consiglio Prodi si trova a Trento, in un teatro dove recita la sua parte, viene avvertito che dei *no global* avrebbero infastidito il suo intervento, questi entrano impunemente in un teatro, nessun

il principio della casualità. Che brutta figura che ha fatto il Governo davanti al Paese. E tutto questo per fare quadrato attorno ad un Vice ministro in un Governo che vanta 102 posizioni di Governo e di sottogoverno? A noi fa molto più specie - devo dirlo - il comportamento di una certa sinistra che della correttezza vorrebbe farne un baluardo, l'Italia dei Valori, che si piega ad accettare posizioni insostenibili da parte della maggioranza.

altro, non si fa nemmeno il reggimoccolo a un Governo che ormai è come il burro rancido, che non si sa per quanto tempo possa ancora essere buono. Penso che il vice ministro Visco possa essere anche, forse, una persona seria e in questi casi le persone serie lasciano prima che gli si chieda di lasciare, almeno in un Paese normale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi auguro che coloro che hanno, ultimamente e giustamente, denunciato la crisi ed il costo della politica, abbiano ora il coraggio di denunciare anche l'arroganza della politica, l'arroganza della politica, ridotta a cinica e proterva gestione del potere proprio dall'Unione prodiana, il cui fallimento nella funzione dell'esercizio governativo è sotto gli occhi di tutti ed il cui fallimento progettuale è reso evidente dalla lenta, ma graduale implosione della maggioranza di centro-sinistra. Quella che noi oggi, in vario modo e a vario titolo, stiamo valutando è infatti solo una squallida storia di prepotenza, il cui protagonista è un Governo pavido, privo di qualsiasi rispetto delle istituzioni e privo, soprattutto, di qualsiasi senso del pudore. Sì, quella che noi oggi stiamo giudicando è la banale - ma grave - storia di un Governo che ha voluto arbitrariamente rimuovere ed allontanare quegli ufficiali della Guardia di finanza che indagavano *(Applausi (magari riuniti in cooperativa) del Governo, onde evitare ulteriori danni ed imbarazzi a se stesso e alla propria incerta maggioranza. È una storia esemplare di malgoverno e di arroganza ed è una storia talmente chiara, nella sua dinamica e nelle sue ragioni di fondo, da essere perfettamente intesa e compresa dagli italiani, senza bisogno di commenti o spiegazioni, tanto che Silvio Berlusconi (il quale possiede come pochi il dono di entrare in sintonia con gli umori e i sentimenti della gente) ha osservato provocatoriamente: «Ma ve lo immaginate se il mio Governo avesse per caso preso analoghi provvedimenti verso quei finanzieri che indagavano sulle aziende del gruppo Fininvest?

richiama tutti noi ad una comune assunzione di responsabilità verso la Repubblica, la quale non può essere al contempo onorata e irrisa, celebrata e oltraggiata. Si apre perciò una grande questione civile: sapere se è ancora valido l'assetto istituzionale della Repubblica italiana, che ha contenuto le funzioni di Governo nell'indirizzo generale ai Corpi armati e alle Forze di polizia, lasciando a queste il dovere di ordinarsi nel rispetto della legge, o se invece tale assetto è stato di fatto superato, per lasciare alla politica (voluta dall'Unione prodiana) il compito di invadere ogni ambito istituzionale, asservendo tutto e tutti, compresi i Corpi di Polizia. Non è, a mio avviso, una questione dalla quale il Capo dello Stato - lo dico con il massimo rispetto - può chiamarsi fuori. Prigioniero della sua visione arrogante, prepotente e invadente della politica, il Governo Prodi, anziché chiarire pubblicamente e davanti al Parlamento i motivi del clamoroso contrasto sorto tra il vice ministro Visco e il comandante generale della Guardia di finanza Speciale, ha preferito da un lato cacciare quest'ultimo, promuovendolo alla Corte dei conti e dall'altro ritirare le deleghe sulle Fiamme gialle a Visco, dopo averlo sempre protetto e giustificato. Il che è obiettivamente paradossale perché tale scelta ammette implicitamente l'esistenza di ombre inquietanti nell'azione del vice ministro Visco, pur colpendo esclusivamente il comandante Speciale, reo di aver tutelato i propri uomini, oltre che la dignità, l'autonomia e l'operatività della Guardia di finanza. Ora, per difendere l'indifendibile Visco, alcune disperate frange del centro-sinistra si trovano addirittura costrette a ricorrere all'invenzione di congiure e complotti, evocando, sullo sfondo di logge massoniche deviate, un inesistente tintinnar di sciabole; per non parlare della vergognosa diffamazione di cui è fatto oggetto la persona e la carriera del generale Speciale, al quale va tutta la mia incondizionata solidarietà. Sarebbe facile, Presidente, obiettare al Governo tutta una serie di considerazioni che altri colleghi hanno fatto. Prendo semplicemente atto che, in tanta confusione politica ed istituzionale, il presidente del Consiglio Romano Prodi tende sempre più ad assomigliare ad Aiace, che reso folle dagli dei per la sua arroganza, devastò inutilmente il proprio campo - il campo degli Achei - scambiando le pecore per uomini e perdendo

alcun pregiudizio ostile nei confronti dell'onorevole Visco; direi che ho piuttosto simpatia nei suoi riguardi, perché ricordo suo padre che è stato uno dei più diretti collaboratori di un mio antico maestro, l'onorevole Oronzo Reale quando questi era Guardasigilli. Non ho alcun pregiudizio ostile, ma non condivido la sua concezione sul ruolo della politica quale è emersa da questa vicenda. Non indulgo ai facili qualunquismi oggi di moda e non contesto né il ruolo né il primato della politica, ma questi vanno collocati nelle loro giuste dimensioni quando si tratta di rapporti con le strutture burocratiche o con le Forze armate; in una dimensione cioè, come mi ha insegnato Ugo La Malfa, che non interferisca con i compiti e i poteri delle strutture amministrative, rispetto alle quali il potere politico deve limitarsi a dare direttive generali. So che è un confine sottile perché se il politico rinuncia alla sua funzione di indirizzo abdica ai suoi compiti, ma se invece supera questo limite, invadendo le sfere di competenza di altri organi, esorbita dai suoi poteri, realizzando un sopruso. Nel caso dell'onorevole Visco, di cui stiamo discutendo, mi sembra si configuri la seconda ipotesi: l'ipotesi di un potere politico che ha invaso altre sfere, realizzando non in termini penali, ma certamente in termini di responsabilità politica, un abuso di potere. Io non entrerò nei dettagli della vicenda che hanno riguardato la richiesta di spostamento dei vertici della Guardia di finanza in Lombardia né sulle cause che l'hanno ispirata; su questo si sono già ampiamente intrattenuti altri colleghi. Mi limiterò sul punto a dichiarare che considero invero strumentale la campagna posta in atto da un autorevole quotidiano nazionale che, con l'obiettivo di delegittimare i vertici della Guardia di finanza e di sostenere in conseguenza il Vice ministro, che pure dichiarava di volere criticare, ha parlato di una nuova P2 che si sarebbe infiltrata negli apparati dello Stato. Quello che mi preme sottolineare è che in questo caso si è invece espressa una concezione distorta del primato della politica, ma soprattutto che questa non è stata la sola occasione. Sulla base di notizie apparse sulla stampa, essa si era già manifestata in altri due episodi in cui vi erano state invasioni ingiustificabili di ambiti di competenza. Mi riferisco innanzi tutto ad un episodio che risale al 2001 e che è stato rievocato in questi giorni. L'onorevole Visco, allora ministro dell'economia, avrebbe chiesto al presidente della Camera, Luciano Violante, di destituire il capo del servizio studi della Camera dei deputati, reo di avere espresso, parlando a titolo personale in un seminario dell'Associazione Mario Rossi, dubbi sulla tenuta dei conti pubblici ed ipotizzato l'esistenza di un extra-*deficit*. In quella circostanza, solo grazie alle procedure garantiste relative alla nomina dei consiglieri dell'amministrazione della Camera, non fu possibile esaudire la richiesta di Visco. Ne derivò tuttavia una curiosa lettera del Segretario generale della Camera diretta a tutti i dipendenti che li richiamava - ma nasceva dal quel caso - al rispetto dei principi di imparzialità e terzietà nell'esercizio dei propri diritti costituzionali e politici per evitare che l'Amministrazione della Camera si trovasse coinvolta nella competizione tra parti politiche. Fu proprio così, colleghi. Il secondo episodio è quello denunciato sulle colonne de «il Giornale» del 3 giugno dall'ex direttore dell'ANSA, la prima agenzia di stampa italiana, Pierluigi Magnaschi, e relativo al suo licenziamento, sollecitato dal Governo perché reo di aver riportato in un'agenzia del 16 luglio 2006 la notizia che era stata chiesta la decapitazione del vertice dalla Guardia di finanza di Milano in relazione alla vicenda delle intercettazioni telefoniche sul caso UNIPOL. Non è chiaro, in questo caso, se le pressioni fossero giunte dal Vice ministro dell'economia o da altri esponenti del Governo. Quello che comunque è evidente è che la richiesta sarebbe stata avanzata per avere l'ANSA divulgato la notizia di una pressione indebita riferibile all'onorevole Visco. Quindi, quello di questi giorni sarebbe il terzo episodio e, come dicono i processualisti, tre indizi concordanti formano una prova. La prova di una concezione del ruolo del potere politico che va nella direzione esattamente opposta a quella che dovrebbe essere seguita per mantenere un quadro di corretti rapporti tra organi politici e organi amministrativi, tra esponenti di Governo e organi di informazione. La dimostrazione di una intolleranza verso chi dissente, che è propria di una certa sinistra nostrana. Ecco perché l'attuale vicenda trascende dal singolo episodio ed assume una valenza più generale: quella di un pessimo costume cui l'attuale Esecutivo si è abituato e che è pericoloso per un corretto funzionamento delle nostre istituzioni. Un corretto funzionamento che non può certo essere ripristinato fingendo che nulla sia accaduto e revocando contemporaneamente all'onorevole Visco le deleghe relative alla Guardia di finanza solo per superare i contrasti interni che erano emersi nella coalizione. Un corretto funzionamento per cui è indispensabile l'accoglimento della richiesta delle opposizioni di assicurare, non in via transitoria ma definitiva, che il Corpo della Guardia di finanza dipenda a tutti gli effetti dal Ministro dell'economia, ponendo così fine ad un processo di lottizzazione degli apparati dello Stato all'interno delle componenti dell'attuale maggioranza. Non ci illudiamo che l'accoglimento di questa richiesta possa da sola riparare il *vulnus* che si è verificato tra il potere politico e l'Arma: i danni introdotti rischiano di essere di più vasta portata, ma almeno un segnale di ripensamento verrebbe dato. Temiamo, però, che questo Governo e questa maggioranza non vorranno né potranno dare nemmeno questo timido segnale.

onorevoli colleghi questo dibattito si svolge sulla base di notizie di stampa non confermate né smentite dal Governo. È inevitabile che riecheggi una certa aria di chiacchiericcio, come ha notato altro senatore in un intervento precedente, ma la colpa non è del Senato, è del Governo. Non abbiamo, infatti, una versione ufficiale del Governo degli eventi oggetto della discussione in quest'Aula: non sappiamo quale sia la situazione di fatto e non sappiamo neppure quale sia la situazione di diritto. La Corte dei conti non ha ancora registrato il decreto di nomina nel nuovo comandante e nemmeno la revoca del comandante precedente. Voci di corridoio - e a queste voci dobbiamo fare riferimento, visto che non si fa sentire la voce del Governo dicono che il decreto non sarà registrato tanto facilmente, perché vi è un evidente difetto di motivazione. Vorrei dire alla senatrice Finocchiaro che non è politicamente irrilevante sapere se il Governo ha agito in eccesso di potere, e quindi è oggetto di una doppia censura, oppure ha agito all'interno dei suoi poteri ed è oggetto di una censura sola, quella politica. Un Governo che non rispetta la legalità è pericoloso per il Paese assai più di un Governo semplicemente incompetente. Difetto di motivazione. Certo, ben più penetrante è il dovere di motivazione politica che il Governo deve ottemperare davanti al Parlamento.

sappiamo però anche qualcosa di più di ciò che ci ha detto: che il Presidente degli Stati Uniti ha il dovere di motivare davanti alla Camera dei rappresentanti le proprie decisioni e, se non lo fa in modo convincente, se è colto nell'atto di fornire motivazioni false e pretestuose, allora può essere persino il Presidente degli Stati Uniti a trovarsi nella necessità di dare le dimissioni. Mi spiace che tanta sapienza del senatore Furio Colombo sia stata sprecata su di una questione che non c'è: nessuno contesta il diritto del Governo di mandare a casa un generale,

Quali sono le motivazioni reali del dimensionamento del generale Speciale? Che non si tratti di un normale avvicendamento sembra evidente. Quello che ho capito è che il vice ministro Visco voleva imporre il trasferimento d'urgenza, senza osservare le procedure ordinarie, di alcuni ufficiali impegnati in delicatissime indagini che avrebbero potuto coinvolgere importanti personaggi della politica. La procedura ordinaria prevede che gli ufficiali siano interpellati e diano il gradimento alla sede loro proposta; in questo caso ciò non sarebbe dovuto avvenire: è una procedura punitiva, ma non è chiara quale sia la mancanza che avrebbe dovuto essere punita. Sono debitore di questa ricostruzione ad un illuminante intervento del ministro Di Pietro, non è una ricostruzione di parte. Noi ci domandiamo: perché mai il Vice ministro si è interessato con tanta premura di questi trasferimenti? Il Vice ministro ha poteri di indirizzo politico e non di gestione; questi appartengono al comandante generale della Guardia di finanza. Il generale Speciale, non ravvisando ragioni per punire i suoi uomini, li ha difesi. Vorrei dire al senatore D'Ambrosio che il generale Speciale ha interpellato la procura della Repubblica per conto della quale le indagini venivano svolte, la quale ha detto che quelli rimanessero al loro posto; quindi - conformemente a ciò che dottamente ha spiegato il senatore D'Ambrosio - il generale Speciale avrebbe commesso un reato se avesse trasferito quegli ufficiali. Il generale Speciale ha fatto ciò che un dirigente, militare o civile, ha il dovere di fare: ha difeso i suoi uomini contro un'ingiustizia e questo certamente ha dato grande prestigio a lui come persona, ma anche all'istituzione comandante della Guardia di finanza

Nell'assenza di una chiara presa di posizione del Governo, ci tocca leggere i giornali e seguire le ipotesi che ci forniscono. Il quotidiano Torino, notoriamente vicino al Governo, afferma che esisterebbero intercettazioni compromettenti per un membro del Governo in relazione ad una maxitangente distribuita dal dottor Consorte. Leggo da «La Stampa» di Torino di oggi: «D'Alema, i veleni delle spie Telecom e i conti segreti in Sud America». Tengo a dire subito che ho stima del ministro D'Alema, sono convinto che queste sono infami calunnie; voglio segnalare che queste infami calunnie vengono dell'interno della maggioranza e sono il sintomo evidente di un regolamento di conti tutto interno alla maggioranza. Questo sarebbe il segreto che doveva essere protetto ad ogni costo. La colpa di Speciale sarebbe allora - questo il giornale non lo dice ma lo lascia facilmente immaginare - di non avere collaborato alla custodia del segreto. Il giornale «la Repubblica», noto anch'esso per le sue posizioni di organico sostegno alla maggioranza e direi quasi portavoce autorizzato del Governo, ci fornisce un'altra versione, forse alternativa, forse complementare, ma certo ancor più infamante per il Governo. «Il generale Speciale e il generale Pollari sarebbero al centro di una vera e propria congiura per condizionare i poteri dello Stato...». Una specie di loggia P3. «Tale loggia sarebbe protetta dal Ministro della difesa e dall'intero Governo, tanto che il Governo Prodi avrebbe apposto il segreto di Stato alla vicenda del sequestro di Abu Omar, cosa che il Governo Berlusconi si sarebbe invece rifiutato di fare». Sono tutte affermazioni del giornalista D'Avanzo del quotidiano «la Repubblica» non mie. Di nuovo «...Sono convinto che il ministro Parisi sia una persona di specchiata probità e voglio dirgli qui la mia solidarietà contro queste accuse infamanti». Questo Questo è un regolamento di conti tutto interno alla maggioranza. Queste accuse vengono dall'interno della vostra maggioranza. C'è il diritto di aspettarsi querele da parte degli esponenti del Governo citati verso gli estensori di questi articoli. Di tali querele, però, fino ad ora non vi è notizia. Cosa dobbiamo pensare? Una cosa è certa, ci troviamo davanti ad un regolamento di conti. Due dei più importanti giornali che sostengono il Governo contro due dei Ministri più prestigiosi del medesimo Governo. Se il generale Speciale è colpevole di ciò che "la Repubblica" gli attribuisce avrebbe dovuto essere allontanato da tempo. Il ritardo con cui l'allontanamento è avvenuto esporrebbe il Governo al sospetto di essere ricattato dalla rete di potere costruita da Speciale o di essere colluso con essa. Dovrebbe dare le dimissioni solo per questo. Se quelle pagine fossero vere, il Governo dovrebbe dare le dimissioni a prescindere. Attenti Attenti quindi, cari colleghi della maggioranza, a riecheggiare in quest'Aula quelle accuse, perché il significato politico di quello che qualcuno di voi ha detto è che il Governo si dovrebbe dimettere immediatamente.

chi sto citando. «E' necessario che sulla vicenda Visco e Speciale venga fatta chiarezza. È il Governo che in questo caso deve fornire spiegazioni su quanto è successo per cui oggi, nell'Aula di Palazzo Madama, mi aspetto che il rappresentante scelto dall'Esecutivo dissipi i dubbi e faccia chiarezza sulle pressioni che il vice ministro dell'economia Vincenzo Visco avrebbe esercitato sui vertici della Guardia di finanza per la rimozione dei quattro ufficiali impegnati presso la procura di Milano in alcune scottanti inchieste in ambito finanziario. In particolar modo, vorrei fosse fatta luce sulle modalità di sostituzione del generale Roberto Speciale. Nell'incontro straordinario del Consiglio dei ministri che si è svolto ieri mattina....». Chi chiede di sapere queste cose è il ministro Di Pietro, che fa parte di questa maggioranza. Signor Ministro, scricchiolano strutture fondamentali dello Stato, si indebolisce il patto di fedeltà che lega i servitori dello Stato allo Stato che servono ed i cittadini in generale allo Stato di cui sono cittadini. Si preannuncia una stagione di veleni che non può non preoccupare profondamente tutti coloro che hanno a cuore il bene comune del Paese. Si sta levando dal fondo del Paese un'ondata di antipolitica, che minaccia di travolgere il prestigio e la credibilità di tutte le istituzioni. Colleghi senatori, potete dare un voto di sostegno al Governo per mera appartenenza di partito, per paura delle conseguenze, per rimanere ancora un poco nell'illusione di un progetto politico che ormai è fallito, oppure potete avere il coraggio di un gesto di libertà che consenta di aprire una fase nuova nella vita del Paese. Signor ministro Padoa-Schioppa, non copra con il suo prestigio, guadagnato con una vita spesa al servizio dello Stato, un Governo che la manda avanti ad assumersi responsabilità che non le competono. Dia le dimissioni e inviti il Capo del Governo a fare la stessa cosa, perché ci si possa poi mettere attorno a un tavolo per assumere insieme la nostra responsabilità di politici e di cittadini per il bene dell'Italia. *(Applausi dai Gruppi UDC e FI. Congratulazioni).*

Nulla vieta situazioni del genere, ma conoscendo il suo passato di magistrato e le sue doti di persuasione, credo che in questo momento sia perlomeno inopportuno un rapporto del genere e chiedo pertanto che il Senato assuma informazioni sui *pass* di ingresso dei suddetti personaggi.

atto parlamentare intriso di tentazione agitatoria o di derubricare il confronto che si svolge in Aula a livello di un contenzioso da Tribunale amministrativo regionale.

stiamo affrontando una questione fondamentale per il corretto rapporto all'interno delle istituzioni e per il corretto funzionamento di una democrazia parlamentare.

Kelsen aveva una concezione procedurale della democrazia; non a caso il marxismo contesta tale approccio con il concetto stesso di democrazia e oppone la democrazia sostanziale alla democrazia formale. Il buon marxista Visco, che ragiona ancora in questi termini (penso sia uno degli ultimi comunisti rimasti in Italia), in realtà, in realtà, segue un modello di democrazia sostanziale chavista sudamericana, cioè non tiene conto delle regole e ritiene che e ritiene che la democrazia non debba ispirarsi al rispetto di determinate procedure.

Anche l'ex ministro Bassanini ha chiarito, in questi giorni, che il Governo ha il potere di nominare il comandante della Guardia di finanza, ma non i suoi sottoposti. Qual è la dinamica di tutta questa vicenda? Perché il comportamento del vice ministro Visco è eversivo, cioè un comportamento di chi non rispetta le regole e le norme giuridiche?

con l'allora comandante della Guardia di finanza Mosca Moschini circa l'impiego di alcuni sottufficiali della Guardia di finanza; Mosca Moschini rispose a Visco che, per quanto riguardava gli impieghi ed i trasferimenti relativi alla Guardia di finanza, la competenza era sua esclusiva aveva un solo obbligo, cioè quello di informarlo. Il vice ministro Visco è recidivo perché il 21 giugno 2006, nell'occasione della festa della Guardia di finanza, si è occupato

i Governi di centro-sinistra: quando governa il centro-sinistra si stratifica una grande quantità di evasione fiscale e poi bisogna procedere con i condoni.

senza tener conto del fatto che il potere politico ha soltanto la facoltà di nominare il comandante della Guardia di finanza, ma non i suoi sottoposti. Il vice ministro Visco comincia a indire riunioni anomale, eversive - queste sì sì - e conflittuali contro la catena di comando della Guardia di finanza, con due ufficiali, il comandante in seconda Italo Pappa e il comandante della scuola Sergio Favaro. Favaro e Pappa si accordano con Visco alle spalle di Speciale: vogliono far carriera e allora dicono al Vice ministro di esser disposti a violare quei princìpi e quelle norme giuridiche poste a salvaguardia della terzietà del Corpo della Guardia di finanza e, sostanzialmente, a fare in modo che egli entri e dia indicazione negli spostamenti, nei trasferimenti e nelle progressioni di carriera nella Guardia di finanza.

il generale Forchetti, il colonnello Lorusso, il colonnello Pomponi ed il tenente colonnello Tomei, quattro ufficiali che lavorano a Milano. Pappa e Favaro da questo momento in poi diventano una sorta di commissari politici della Guardia di finanza. Avviene però qualcosa di più grave. Il generale Michele Adinolfi, comandante del Primo reparto, scopre che il suo sottoposto, il colonnello Rapanotti, è convocato, all'insaputa del Comandante generale, dai generali commissari politici Favaro e Pappa, che gli dettano i trasferimenti da effettuare. Badate bene che al colonnello Rapanotti viene detto di non parlare di quei trasferimenti con il suo diretto superiore. Non so come faccia

il generale Speciale, perché con il suo comportamento ha inteso difendere la democrazia in questo Paese. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, solo pochi minuti per formulare qualche osservazione sulla grave vicenda che ha coinvolto il Vice ministro dell'economia e delle finanze e il Comandante generale della Guardia di finanza e per rivolgere un appello al Governo sulla politica fiscale. In questa situazione molto difficile, il comportamento del Governo non mi è sembrato lineare. Avrei preferito che le decisioni in merito al generale della Guardia di finanza Speciale fossero state prese una volta chiarita

Approfitto anche per intervenire in merito alla politica fiscale del Governo che non riesco più a condividere e non sono l'unica. Lo si vede dal crescente disagio di tutti i contribuenti (politica fiscale inadeguata per le famiglie, per i dipendenti e per le imprese). La pressione fiscale è insostenibile a causa della indetraibilità dei costi previsti nella legge finanziaria, con effetto retroattivo e il conseguente aumento della base imponibile. Per le imprese, in casi non rari, la pressione fiscale è cresciuta, addirittura, al di sopra del 70 per cento. Ho qui un esempio, che vorrei far mettere agli atti,

Le modifiche apportate nell'ultima finanziaria hanno reso questo strumento totalmente inadeguato a rispecchiare le singole realtà economiche. Mi risulta, infatti, che addirittura più del 70 per cento delle piccole imprese con punte nelle attività marginale del 90 per cento non riescono a rientrare nei parametri stabiliti per l'anno 2006. Signor Ministro, qui ci vuole un intervento immediato per non mettere a rischio tutto il mondo delle piccole imprese, pilastro fondamentale della nostra economia. Gli obblighi burocratici sono ingestibili. Le nostre richieste di semplificazione, di snellimento delle procedure burocratiche quando hanno a che vedere con il fisco rimangono lettera morta. Pensiamo solo alla reintroduzione degli elenchi clienti e fornitori dopo anni dalla loro abolizione; a tutti gli invii telematici previsti, con particolare riferimento all'invio telematico dei corrispettivi; alla richiesta preventiva di autorizzazione alla compensazione IVA; all'invio delle comunicazioni dei dati e delle notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate, e via dicendo. A parole sembra tutto molto semplice, ma dietro ogni provvedimento che prevede obblighi burocratici ci sono dei costi di adeguamento che ogni impresa deve sostenere. Costi non preventivati che, per le piccole e medie imprese, hanno una grossa rilevanza. Per non parlare poi dell'assoluta incertezza legislativa. Vengono cambiate le leggi in continuazione, vengono cambiate con effetto retroattivo e addirittura con circolari e comunicati stampa. Abbiamo esperienza di situazioni paradossali, come il caso di circolari che contrastano con disposizioni approvate dal Parlamento. Faccio l'esempio della circolare ENPALS n. 6 del 20 aprile scorso che è in contrasto con la norma approvata dal Parlamento e, quello che sconcerta di più, è l'atteggiamento del Governo che, nonostante le ripetute proteste di noi parlamentari, non riesce a far rispettare ai propri uffici pubblici competenti una legge dello Stato. uffici pubblici competenti una legge dello Stato. Ci si trova in continua emergenza legislativa testimoniata dall'importanza dei comunicati stampa dell'Agenzia delle entrate che hanno assunto, in più di un'occasione, la funzione di atti normativi perché annunciano proroghe dei termini che in genere sono formalizzate con notevole ritardo lasciando i contribuenti in completo abbandono legislativo. Signor Ministro, concordo pienamente con la necessità di combattere l'evasione fiscale, ma non concordo con il metodo adottato. I risultati non si ottengono aumentando la pressione fiscale fino all'insostenibile e rendendo difficoltose e macchinose le procedure per gli adempimenti. Non dobbiamo inventare niente di nuovo, basterebbe solo copiare dai Paesi a noi più vicini. Dobbiamo: - abbassare la pressione fiscale ad un livello accettabile, - ridurre gli obblighi burocratici, - effettuare controlli mirati, soprattutto nei territori a più alta concentrazione di evasione e non tartassare i contribuenti onesti con controlli oppressivi e sanzioni su formalità. del genere. Bisogna smettere di considerare tutti gli imprenditori come evasori e disonesti!

a meno che non riceva un ordine preciso ed indiscutibile dal mio partito e che in replica non ci sia una chiara risposta del Governo ai problemi da me sollevati.

la questione di cui ci stiamo occupando è estremamente inquietante e delicata. La materia del dibattere scaturisce da atti e atteggiamenti riconducibili a due note personalità, entrambe differentemente applicate al servizio dello Stato e delle istituzioni. Due persone che continuano a fornire sulla nota questione versioni distorte e spesso fra di esse antitetiche. L'una, evidentemente, dice il vero; l'altra, altrettanto evidentemente, non può che dire il falso. E fin qui tutto fila liscio. Ma chi delle due dice il vero? Ecco il punto.

e pongono in evidenza una condotta del Governo confusa e confusionaria, incerta e pavida, reticente e perfino autolesionista. Un Governo che così realizza, una sfilza di veri e propri misfatti e oltraggi all'indirizzo della politica,

Un Governo che attraverso un suo Vice ministro vuole imporre ai vertici del Corpo delle Fiamme gialle il trasferimento di quattro ufficiali, già valorosamente ed impeccabilmente impegnati in delicatissime inchieste. Che vuole fare ciò senza addurre ragioni serie e nemmeno lievi; ragioni che ad oggi non si conoscono, se non per informazioni e illazioni della carta stampata. un pessimo servizio reso dal Governo alle istituzioni, ai cittadini, persino alla sua stessa credibilità. A me tocca dire, sinceramente non con gaudio, tenuto conto del danno ampio e generale perpetrato al Paese, che chi governa deve avere, costantemente e tenacemente, viva e forte la sollecitudine per il bene comune. Il che vuol dire possedere la capacità, fatta di intelligenza e di iniziativa, di decisione e di temperanza per gestire la *polis*; che chi governa deve avere chiaro il convincimento, nei fatti e non nelle chiacchiere, che l'esercizio della politica e la politica stessa inconcepibili senza l'ispirazione e il supporto di forti valori etici. Il che vuol dire che la politica è ben più di una tecnica amministrativa. È opera dell'uomo per l'uomo. sollecitudine vigile e operante per la dignità della persona umana e per i valori che liberano e costituiscono la persona stessa. Chiediamoci come inquadrare in questa riflessione la dignità ed il senso dello Stato delle persone, del generale Speciale e dell'onorevole Visco. A me pare, ripeto, senza voler fare il giudice della situazione, che entrambi i protagonisti escano enormemente malconci; l'uno, in quanto vittima; l'altro, in quanto incauto e sbrigativo aggressore. E non pare esservi dubbio, almeno questo, su chi sia l'aggressore, visto che a dare fuoco alla miccia risulta essere stato il vice ministro Visco,

se il Vice ministro avesse fatto ciò che ha posto in essere in base a motivazioni vere e forti, mediante procedure oculate e trasparenti.

che, proprio perché così, ci fa sentire responsabili non soltanto dei propri atti, ma anche di quelli degli altri. Fa sentire responsabili tutti. E qui è il punto, cari colleghi:

per il suo modo di operare e di rapportarsi con esso, continuando ad alimentare il discredito nella politica, nelle istituzioni politiche ed ora anche verso Corpi essenziali e portanti dello Stato? Può il Governo continuare a far finta di niente e di nulla, attraendo e coinvolgendo nel recinto della responsabilità oggettiva verso il Paese anche le forze politiche dell'opposizione, a motivo e a causa dei danni e del discredito da esso perpetrati alla politica mediante la sua insipiente ed ibrida conduzione della politica e dell'attività governativa? È stato scritto che l'atmosfera è per il Governo da ultimi giorni di Pompei. Non lo so e personalmente non sono affascinato dallo sport dell'esercizio previsivo. Concludo, osservando che il convoglio del Governo, dopo questo episodio, è proprio giunto ad una stazione di confine: o trova la forza,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il cuore di tutto il dibattito di questi giorni si incentra, paradossalmente, su fatti pubblici e incontestabili: le pressioni indebite sul Comandante generale della Guardia di finanza da parte del vice ministro Visco, fatti che avrebbero dovuto portare ad una sola possibile soluzione: le dimissioni del Vice ministro e la sua incriminazione per abuso d'ufficio. Ciò è, infatti, testimoniato dalle missive. Basta citare, al riguardo, la lettera con la quale il vice ministro Visco ha, *per tabulas*, imposto perentoriamente a Speciale di concertare ogni decisione futura direttamente con i due sottoposti, i generali Italo Pappa e l'allora capo dei reparti d'istruzione Sergio Favaro, persone che il Vice ministro aveva appena incontrato. La circostanza rappresentava, di fatto, una sorta di esautoramento del Comandante generale. Il comportamento del Vice ministro è stato peraltro reiterato, com'è noto, appena tre mesi fa. Il 16 marzo scorso Visco scrisse: «Devo peraltro ribadire nell'occasione che eventuali ulteriori ipotesi di designazioni dovranno avvenire solo all'esito di un preventivo e approfondito confronto sulle motivazioni delle stesse con l'autorità politica». Ciò, quindi, in pieno dispregio di quanto ha previsto la normativa del decreto Bassanini, che ha scisso la responsabilità politica da quella amministrativa. Proprio questa lettera fa cadere tutte le accuse rivolte agli ufficiali, ovvero di essere vicini all'ex ministro Giulio Tremonti o di essere frutto di una gestione privatistica del Corpo. È vero proprio il contrario. Emerge infatti che Visco ha inteso e intende la Guardia di finanza come un Corpo militare sul quale può esercitare ogni ingerenza. Ed alla fine, dobbiamo amaramente constatare che è andata proprio così; pressione dopo pressione, lettera dopo lettera, ingerenza dopo ingerenza, il generale Speciale è stato messo alla porta. A Visco sono state tolte le deleghe, ma solo temporaneamente, finché, si spera, la magistratura non farà chiarezza. Appare allora chiaro come il Comandante generale della Guardia di finanza si sia reso colpevole solo di aver tutelato le sue prerogative istituzionali e la dignità delle Fiamme gialle dalle illegittime interferenze del vice ministro Visco. Si colpisce un servitore dello Stato che ha avuto il torto di difendere i propri uomini e di pretendere il rispetto delle regole anche da parte della politica. Siete attestati su una pericolosa deriva di autoreferenzialità e ci esponete a una pessima figura in ambito internazionale.

approfondisca meglio: qui si parla di UNIPOL e non di missioni o guerre. Inoltre, porre la questione di come Berlusconi parli l'inglese è un atto saccente o piuttosto un sentimento d'invidia per non aver fatto ciò che il presidente Berlusconi ha realizzato con l'incontro a Pratica di Mare, che consentì il superamento della "guerra fredda". Chieda al suo Presidente del Consiglio, che l'inglese lo parla molto bene, cosa sta facendo. Non pare che ad oggi stia ottenendo brillanti risultati in politica estera. Comunque, dobbiamo nuovamente affermare di essere nel pieno di una grave emergenza democratica. Non possiamo credere che non ci siano più in questo Paese istituzioni indipendenti in grado di arrestare questa deriva autoritaria di un Governo irresponsabile. Si tratta, peraltro, di una decisione senza precedenti. I comandanti del Corpo, salvo casi di conclamata corruzione, sono infatti sempre cessati per raggiunti limiti di età. La decisione della rimozione d'imperio è invece sempre un atto traumatico, che va ponderato mille volte e va adottato solo in casi estremi. A ciò va aggiunto che sono peraltro numerosi i dubbi di legittimità Basti dire solo questo, esso è stato assunto in un Consiglio dei ministri semideserto: il ministro d'Alema ha preferito dedicarsi ad altro, forse alla vela, e altri Ministri hanno invece semplicemente disertato la riunione.

Forse un ristoro economico? No. Egli ha rifiutato l'*excusatio non petita* della nomina alla Corte dei conti ed ha semplicemente chiesto di tutelare l'onore, suo e del suo Corpo, manifestando il desiderio di restare in carica almeno fino al 21 giugno, giorno della festa della Guardia di finanza. Riprendo qui alcune parole pronunciate dal COCER della Guardia di finanza, che afferma: «Speciale resterà nei nostri cuori: oggi sarà sereno perché ha dimostrato a tutti la sua rettitudine». Ancora, si legga quanto scrive il COCER dei Carabinieri, il quale, pur non essendo direttamente coinvolto nella vicenda, segnala come la destituzione sia «un atto gravissimo». Il COCER dei Carabinieri ricorda come, se il Governo si vanta molto del famoso tesoretto, questo lo si deve anche agli uomini comandati dal generale Speciale. Insomma, dalle dichiarazioni, dai fatti, dai comportamenti emerge un'altra pagina buia della più becera gestione del potere che sta operando questo Governo. Al generale Speciale ed ai militari delle Fiamme gialle non possiamo che ricordare, in questi bui momenti, il motto araldico del Corpo della guardia di finanza, che, fin dal 1933, consiste nella antica frase latina «*nec recisa recedit*», ovvero «neanche spezzata retrocede». L'onore del Corpo e del suo comandante è stato infatti spezzato

Signor Presidente, il nostro dibattito ruota attorno ad un interrogativo preliminare, ma all'interno delle istituzioni, ed in particolare all'interno dei Ministeri, qual è il rapporto corretto tra il vertice politico e il vertice tecnico? Può darsi che la linea di confine non sia così netta e non sarebbe male se il Parlamento la approfondisse nelle sue linee generali. La legge ci dà una mano: il decreto legislativo prima ricordato del 30 marzo 2001, agli articoli 4 e 16 che non leggo per rispetto nei confronti dell'Aula -, indica la linea di confine. Nella vicenda Visco questa linea di confine è stata superata il Vice ministro ha dolosamente sbagliato nel pretendere il trasferimento nominativo e contestuale di quattro alti ufficiali della Guardia di finanza lombarda: giuridicamente non gli competeva, non compete neanche allo stesso Ministro dell'economia. Ha dolosamente sbagliato a insistere perché il trasferimento avesse luogo in termini tassativi; ha dolosamente sbagliato nel prospettare, neanche tanto implicitamente, pregiudizi alla carriera del generale Speciale, nell'ipotesi di mancato adempimento di quelle pretese; ha dolosamente sbagliato nell'omettere la necessaria consultazione dell'autorità giudiziaria di Milano che si avvaleva della collaborazione del lavoro degli ufficiali che pretendeva di trasferire. Sono circostanze incontestabili, riferite in modo formale, in un verbale, dal generale Speciale non al giornale della famiglia Berlusconi, ma all'autorità giudiziaria di Milano e finora non smentite né da Visco, né dal Governo; riferite su iniziativa della autorità giudiziaria, non su denuncia del Generale; riferite da un soggetto che non è un collaboratore di giustizia che ha bisogno di riscontro, ma da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. In quanto tali, queste parole, valide fino a rigorosa prova contraria e questa prova contraria finora non c'è stata. Non entro nel merito delle ragioni per le quali quei trasferimenti venivano pretesi (le comunichi Visco). Dico solo che se non ci fosse stata la consapevolezza del carattere illegittimo della richiesta, Visco, a fronte della motivata resistenza del Comandante della Guardia di finanza, avrebbe insistito perché quanto lui pretendeva fosse eseguito, invece non lo ha fatto. Sono circostanze che rivelano un modo di fare illegittimo. Prima è stata ricordata la lettera del 16 marzo 2007, che individua non un fatto occasionale, ma un sistema interpretato in modo dolosamente sbagliato. Questi tentativi di prevaricazione, in quanto condivisi nei fatti dal Governo, ne hanno generati altri fino all'illegittima destituzione del Comandante generale della Guardia di finanza; si dirà - lo dice la maggioranza-: «Ma come? Il Governo non può sostituire i vertici delle Forze di polizia»? Ci mancherebbe altro: il Governo in carica ha sostituito il Comandante generale dei Carabinieri e i tre vertici dei Servizi di informazione e sicurezza. Qualcuno ha protestato per queste nomine? Se oggi protestiamo, Presidente, è perché il Comandante della Guardia di finanza è stato rimosso per punirlo della sua legittima resistenza ad un ordine illegittimo. Se oggi protestiamo, cari colleghi della maggioranza, è perché l'avallo al pasticcio che è stato combinato ha un significato grave. Coincide con l'affermazione di un principio che è in dispregio a tutte le disposizioni vigenti. Il principio è che il capo di una forza di polizia deve sempre e soltanto sottomettersi agli ordini del vertice politico, altrimenti viene cacciato. Secondo l'ordine del giorno firmato dai Capigruppo della maggioranza, il Senato dovrebbe condividere e sanzionare questo principio. Chiedo ai colleghi della maggioranza: non siete preoccupati come noi di questa deriva di arroganza e di protervia? Veramente volete votare questo ordine del giorno? Lo dico con preoccupazione. Nella passata legislatura, per cinque anni, ho avuto l'onore di esercitare al Viminale la delega per la pubblica sicurezza; se si avalla questo precedente, domani un Ministro dell'interno, chiunque esso sia, o addirittura un sottosegretario - il Vice ministro è un Sottosegretario che poi ha qualcosa in più dal Consiglio dei ministri, ma mantiene il rango di Sottosegretario - potrà ordinare al Capo della polizia, chiunque esso sia, il trasferimento di un questore che indaga su vicende sgradite e se non lo fa viene destituito. *(Applausi dal Gruppo* *FI)*. Volete veramente votare un principio del genere? Si dirà: «Il Governo è salomonico» perché sostituisce il generale Speciale e sospende le deleghe a Visco. Il Governo è illogico e ingiusto: sostituisce Speciale in modo definitivo e senza motivazioni al momento, mentre sospende temporaneamente la delega a Visco. Se il Senato avalla quanto accaduto, sappia che la sospensione di Visco terminerà lunedì della prossima settimana. Cari colleghi, vogliamo darci appuntamento martedì 12 giugno, alle ore 10, alla Scuola di polizia tributaria con sede a Ostia? È prevista la cerimonia di chiusura dell'anno di studi 2006-2007 con la consegna dei diplomi agli ufficiali che hanno frequentato il corso biennale di polizia tributaria. Alla cerimonia è annunciata la presenza del nuovo comandante generale della Guardia di finanza e di chi?

compirà un atto di esercizio della propria delega; quindi, già da oggi siamo certi che la sospensione durerà non più di cinque giorni a partire da questo momento. È ammissibile che la presa in giro giunga a tanto? Veramente si ha voglia di fare finta di nulla? Veramente hanno voglia di farlo coloro, come il senatore Villone ed altri con lui, che hanno criticamente fortemente l'operato del Governo? Il rispetto per le istituzioni passa per una chiara presa di distanza dalla condotta tenuta dal vice ministro Visco. Il Senato ha questa sera la facoltà di scrivere una pagina di dignità in una vicenda squallida, contrassegnata dalla prevaricazione e dall'arroganza. Non lasciamoci sfuggire, colleghi, questa occasione.

L'aggressione contro Visco è tutt'uno con l'attacco generalizzato contro il Governo. Si tratta di un attacco pretestuoso ed infondato. Vorrei partire da una domanda che riguarda il passato: è vero o no che con il Governo Berlusconi intere catene di comando della Guardia di finanza, a cominciare dalle sedi periferiche del II Reparto, addetto all'*intelligence*, sono state azzerate e sostituite?

Sapevamo di queste sostituzioni; avevamo ragione di credere che esse fossero legate ad apprezzamenti discrezionali e politici ispirati dallo stesso Tremonti; non abbiamo voluto polemizzare poiché le polemiche pubbliche sull'uno o sull'altro funzionario di apparati dello Stato non fanno bene alle istituzioni, anche quando vi sia la fondata persuasione che quei funzionari siano condizionati dalle sponsorizzazioni politiche che li accompagnano. Inoltre, nel 2002 furono sostituiti il comandante regionale della Lombardia, il comandante provinciale di Milano, il comandante del nucleo regionale di polizia tributaria di Milano. Anche qui scelte discrezionali, discutibili, ispirate a criteri non trasparenti di valutazione delle qualità professionali dei singoli. Tutto ciò avveniva mentre si rafforzava, negli stessi anni, un gruppo dirigente nella Guardia di finanza strettamente legato da mille vincoli ai funzionari di vertice del SISMI e mentre nello stesso SISMI si sviluppavano gravi comportamenti illegittimi. Una catena di pesanti illegittimità abbiamo visto all'opera nei cinque anni passati. Ricordo, in proposito, le attività delittuose che facevano capo alla sicurezza Telecom e ad una rete di agenzie investigative private alcuni mascalzoni - in concorso con pubblici ufficiali. Una rete di malaffare e di intrighi che bisognava e bisogna - mi rivolgo agli illustri rappresentanti del Governo - spazzare via. Mi colpisce il fatto che, in continuità con le nomine del 2001, e poi degli anni successivi, e in continuità con il metodo invalso ai tempi del Governo Berlusconi, il generale Speciale, nominato da quel Governo, abbia continuato nell'ultimo anno a compiere nomine con metodo del tutto discrezionale e senza criteri, su una base molto semplice ed elementare, quella dell'*intuitus personae*, che, fuori da ogni regola, è tale da condurre all'arbitrio. Un altro elemento grave di arbitrio, nelle decisioni del generale Speciale, è stato determinato dalla distribuzione degli encomi, indirizzata ad una serie di soggetti prescelti, spesso non si sa perché. La concessione di encomi è così estesa, dettata da motivazioni soggettive e tale da predeterminare gli avanzamenti, da far sì che gli ufficiali encomiati, vicini al capo, possano scavalcare decine e decine di colleghi ed essere ingiustificatamente premiati. A questo genere di arbitrio si ispira l'ultima raffica di nomine disposte dal Comandante generale, avviate a marzo e - se non sbaglio - definite conclusivamente appena pochi giorni fa. Ebbene, l'arbitrio non poteva e non può essere tollerato. Nello stesso tempo, è singolare e preoccupante che, nella scelta dei suoi collaboratori più stretti, lo stesso generale Speciale abbia dimostrato concretamente quanto potesse essere fallace la discrezionalità, quanto fuorviante l'*intuitus personae*, se è vero che nei confronti di uno degli ufficiali a lui più vicini, suo aiutante, è stato richiesto dall'autorità giudiziaria il rinvio a giudizio per un grave reato di peculato. Non credo che si debbano qui citare i nomi delle persone collegate a questo sistema di governo del personale e di direzione della Guardia di finanza. Giudicherà la magistratura, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle regole.

Vorrei ancora rivolgere qualche domanda, che riguarda più direttamente gli ufficiali della Finanza di Milano, le vicende di un anno fa e la campagna politica di oggi. La lettera inviata il 14 giugno dal generale Speciale al vice ministro Visco proponeva una serie di avvicendamenti, già concordati con il Vice ministro, tra i quali vi erano quelli riferiti alla sede di Milano, che solo più tardi sarebbero stati contestati. Quella proposta, riguardante anche Milano, era forse illegittima? No davvero, altrimenti lo stesso generale Speciale non avrebbe dovuto inviare e firmare quella lettera. La sostituzione di quegli ufficiali poteva bloccare o deviare le indagini in corso? Certamente no, e comunque quelle indagini non riguardavano UNIPOL. La motivazione era semplice: in sedi così delicate, la rotazione ragionevole è un bene, è una risorsa positiva. Immediatamente dopo arriva l'attacco mediatico, promosso dalla destra ed incoraggiato dal generale Speciale. I trasferimenti da Milano, nonostante la procedura regolarmente avviata, non si sono poi attuati. Vorrei sottolineare che stiamo parlando di trasferimenti non avvenuti. Si è scatenato, a quasi un anno di distanza, un attacco tanto duro quanto immotivato contro Visco. La regolarità del procedimento seguito avrebbe dovuto essere difesa dallo stesso Comandante generale che vi aveva partecipato. Tanto più che i trasferimenti in discussione non erano avvenuti. Niente di tutto questo. È invece avvenuto il contrario. Il generale Speciale ha consegnato al giornale di proprietà della famiglia Berlusconi un verbale reso davanti all'avvocato generale presso la Corte d'appello di Milano, contenente affermazioni irrilevanti sotto il profilo giudiziario, prive di riscontro e di fondamento, rivolte contro il Vice Ministro ed il Governo. Esistono ragioni sufficienti per affermare che il rapporto di fiducia tra il Governo e il Comandante della guardia di finanza si è rotto. Il decreto di sostituzione è perciò del tutto legittimo e sarà regolarmente registrato. Signor Presidente, cari colleghi, è corretto e giusto che il Governo democratico del Paese fissi il proprio indirizzo, assuma le proprie decisioni. Esso ha il compito di garantire che le istituzioni militari (e tra queste la Guardia di finanza, che secondo la legge istitutiva dipende direttamente dal Ministro delle finanze e comunque i suoi vertici sono nominati dal Governo) siano dirette ed organizzate a tutela del bene comune, a tutela della sicurezza e della dignità della Repubblica.

Signor Presidente, colleghi, faccio una premessa da liberale quale sono.

svolgendo un ragionamento pacato che non dovrebbe mai mancare in un'Aula di un Parlamento democratico. Ripeto, sono un liberale, ho il senso dello Stato, grande rispetto per le istituzioni e grande rispetto anche per gli avversari. In un momento come questo, di crisi preoccupante, che non è solo politica ma in qualche modo investe le istituzioni, sento il dovere di non alzare i toni, come è stato fatto soprattutto - bisogna riconoscerlo - dalla parte della maggioranza, ma di tenerli (lo ripeto nuovamente) al livello della ragione. Mi atterrò all'essenziale della questione che stiamo discutendo, anche perché prima di me altri colleghi ne hanno illustrato, a favore a favore o contro, i vari aspetti. Interverrò inoltre brevemente, perché il tempo a mia disposizione non è poi molto ampio. Qual è la sostanza della questione? Un potere politico - in questo caso un Vice ministro - ha preteso di invadere un potere che non gli spetta per legge, per consuetudine, per tradizione, ledendo l'autonomia organizzativa della Guardia di finanza: questo è il vero problema.

ma è la sua cultura politica che lo ha portato dove è andato in questo caso: questo è il punto. Ma non c'è dubbio che l'onorevole Visco ha dato prova di avere una concezione autocratica dello Stato e delle istituzioni in genere. Non mi dilungherò citando verbali, lettere o testimonianze, già qui abbondantemente citate. Per rimanere all'essenziale - come ho detto

che «eventuali designazioni dovranno avvenire solo all'esito di un preventivo e approfondito confronto con l'autorità politica». Quel "solo" - badate - vale un "Perù" di provocazioni e interferenze. Qui non possono esserci dubbi: c'è una violazione di norme giuridiche e siamo in presenza di un comportamento politico inammissibile;

ma non di imporre disposizioni, trasferimenti, promozioni o altro. Ce lo dice, badate, l'onorevole Bassanini

Nessun dubbio, dunque, che siamo in presenza di principi e norme di legge violati; tralascio di considerare il modo con cui queste violazioni sono avvenute. Ripeto, Visco ha una sola giustificazione, che è la sua cultura politica, la sua concezione delle istituzioni e dello Stato.

a tutto il Governo, perché è il Consiglio dei ministri che ha approvato le misure adottate contro il comandante della Guardia di finanza, e segnatamente

Il Presidente del Consiglio non c'è, ma voglio lasciare traccia di una responsabilità molta grave che gli addebito: di aver preso una decisione assurda, illegittima, comportandosi tra l'altro nelle sue reazioni verso l'esterno con una certa arroganza e addirittura in taluni casi anche con insolenza verso gli avversari, verso l'opposizione. È chiaro che la maggiore responsabilità è sua, ma, signor Ministro dell'economia, lei ci ha messo del suo in questa brutta vicenda, e glielo dico con rammarico perché ho stima di lei per il suo *curriculum* personale: glielo ho già detto, l'ho anche scritto diverse volte e abbiamo avuto già modo di confrontarci nella Commissione di vigilanza RAI.

in cui dice testualmente: «Mi ha chiamato il ministro Padoa‑Schioppa, mi ha detto: siamo arrivati ad un punto in cui bisogna prendere una decisione, allora la cosa migliore sarebbe che lei presentasse una lettera di dimissioni e noi in cambio avremo un occhio di riguardo, le troveremo una buona sistemazione». Ma le pare che si tratti una questione così grave e delicata in questo modo, signor Ministro? Lei non ha smentito il generale Speciale. Questa è la Repubblica italiana, che con tutti i suoi difetti merita di essere onorata, non è il regno di Curlandia! Ma è mai possibile che avvengano fatti del genere? È questo un modo di affrontare una questione tanto grave e delicata? Mi meraviglia, signor Ministro - glielo dico con rispetto e considerazione -, che un uomo come lei si sia lasciato andare a proposte che, me lo lasci dire, somigliano davvero a un baratto. Mi creda, signor Ministro, sono addolorato per lei perché verso di lei, come sa - l'ho scritto più volte nei miei commenti settimanali e gliel'ho anche detto a voce in altre occasioni - ho sempre dimostrato rispetto e considerazione. L'onorevole Prodi in un'intervista ha detto che le cose sono state fatte nel modo giusto.

ministro Visco ha preteso di invadere competenze non sue, il presidente Prodi si è comportato e si comporta con assoluto disprezzo dei più elementari principi istituzionali e di giustizia; onorevole ministro Padoa-Schioppa, non so se per ingenuità politica o per convenienza personale - voglio pensare non per questa seconda ipotesi -, si è reso complice di un grave caso che non ha precedenti.

a discutere sulle vicende che hanno portato il vice ministro Visco alla temporanea rinuncia ad alcune delle sue deleghe e alla sostituzione del Comandante generale della Guardia di finanza. Sono questioni importanti che attengono all'indirizzo generale dell'azione di Governo in tema di politica, di sicurezza,

abbia fatto fronte con assoluta correttezza alle responsabilità di direzione politica del Corpo della Guardia di finanza che la legge gli attribuisce. Da nessuno, anche nel corso di questo dibattito, è stata messa in dubbio l'assoluta legalità del comportamento del vice ministro Visco. Anche i critici più severi dell'operato del Governo hanno sollevato osservazioni ed anche alcune censure di carattere politico o tutt'al più gestionale-amministrativo. Non ho sentito formulare rilievi specifici che sottintendessero violazioni di legge o gravi irregolarità formali. Questo è il punto fermo da cui dobbiamo partire. partire. Onorevoli senatori, premessa la piena legalità dei comportamenti, in tutte le democrazie del mondo, quando viene meno il rapporto di fiducia tra un'autorità militare ed il Governo, il generale lascia al suo posto e il Governo resta. Questo è successo anche nel caso di cui stiamo discutendo e mi preoccupa che l'opposizione possa sostenere che sarebbero state preferibili soluzioni diverse. Infatti, in una democrazia parlamentare soluzioni diverse dalla riaffermazione del pieno ed indiscusso potere governativo a designare, sostituire e nominare i vertici delle Forze armate sono l'anticamera dell'eversione. Per di più, vorrei invitare l'opposizione a prestare molta attenzione ai profondi sentimenti delle nostre Forze armate e della Guardia di finanza, la cui lealtà la cui lealtà democratica e il cui assoluto e convinto rispetto dei poteri del Governo democratico della Repubblica sono fortunatamente molto saldi e radicati. Lo stesso generale Speciale ha reso testimonianza di questa lealtà democratica dicendo "obbedisco", parola che a me, al contrario del senatore Calderoli, fa molto piacere che il generale Speciale abbia pronunciato. Devo dire, con molta franchezza, che la documentazione pubblica sull'ultimo anno del comando del generale Speciale non mi consente di condividere molte delle forme con le quali ha esercitato le funzioni di comandante generale, né la sostanziale assenza di una sua collaborazione con il Vice ministro delegato a guidare politicamente il Corpo. Questi miei giudizi sull'ultima fase del comando del generale Speciale non mi impediscono di esprimere un sincero apprezzamento per la dignità con la quale, sia pure dopo alcune interviste che io giudico imprudenti, ha accettato la decisione del Governo di avvicendarlo al comando e ha anche preferito concludere la sua carriera da comandante della Guardia di finanza piuttosto che da consigliere della Corte dei conti. In terzo luogo, l'opposizione di centro-destra ha voluto politicizzare una vicenda così delicata come quella dei rapporti tra il Comandante della Guardia di finanza ed il Governo. Questo è un modo di fare politica

ed alla protesta della piazza; che senso ha parlare di emergenza democratica o di eversione; che senso ha manifestare con i megafoni e con gli *slogan* davanti al Senato; come è possibile parlare con una leggerezza veramente eccessiva di colpo di Stato e di *golpe*. Vi sembra, senatori dell'opposizione, che queste espressioni siano correttamente utilizzabili oggi in Italia? Italia? Il dibattito sulle vicende delle ultime settimane non sarebbe corretto se non ne comprendessimo le connessioni con la situazione generale del nostro Paese. Sarebbe molto grave se non sapessimo cogliere il valore emblematico della vicenda, il cui significato, se correttamente inteso, va molto al di là delle pur delicatissime attività della Guardia di finanza. L'odierno dibattito pone all'attenzione del Parlamento questioni che travalicano il comportamento delle autorevoli personalità pubbliche che ne sono coinvolte. I veri problemi su cui oggi il Senato dovrebbe soffermarsi sono quelli che stanno a monte della crisi attuale e che in qualche modo l'hanno determinata e ne costituiscono l'origine prima. Signori senatori, oggi il nostro Paese vive finalmente una stagione economica molto favorevole; tutti i parametri hanno un segno positivo. Ciò nonostante, la politica non riesce ad affrontare le grandi crisi strutturali che ci rendono fragili e che generano insicurezza e precarietà. L'economia va bene, ma abbiamo ancora tanto piombo sulle ali. Penso - lo voglio ricordare qui, in Senato - alla crisi strutturale del nostro Stato e di gran parte dei suoi organi, alla crisi del sistema politico e delle istituzioni rappresentative perché so e tutti voi sapete che sono queste crisi profonde ad aver reso possibile che una tensione pericolosa tra chi rappresenta il Governo della Repubblica e chi comanda un corpo militare tanto delicato come la Guardia di finanza si sia trascinata per tanto tempo, sino a produrre il dibattito di oggi pomeriggio. Vorrei segnalare al Senato che la gravissima debolezza del sistema politico sta ponendo le basi perché si apra nel nostro Paese una brutta stagione (simile ad un'altra che abbiamo già vissuto) nella quale i giudizi dell'opinione pubblica, guidata dalla semplificazione dei *media*, potrebbero finire con il prescindere totalmente dalla verità dei fatti, dagli interessi generali, dalla costruttività e persino dalla correttezza dei rapporti tra le persone, tra le parti politiche ed anche tra gli stessi Gruppi parlamentari. Sono di questa mattina ricostruzioni giornalistiche che creano un clima velenoso che oggettivamente rischia di alimentare la destabilizzazione del sistema politico e che può frenare sia la costruzione del Partito democratico (e questo interessa noi), ma anche l'approvazione di una buona legge elettorale, che tutto il Paese, anche l'opposizione, si attende con ansia. Bene hanno fatto, io credo, i Democratici di Sinistra a smentire nettamente l'affermazione calunniosa secondo la quale ad alcuni loro dirigenti nazionali sarebbero ascrivibili conti bancari esteri. Non ho mai avuto dubbi, e non ne ho ne ho nemmeno oggi, sull'onestà politica e morale della dirigenza dei DS: lo voglio riaffermare solennemente nell'Aula del Senato. Ma dobbiamo dirci con chiarezza, onorevoli senatori, che se al termine di questo nostro dibattito tutto dovesse rimanere come prima, se non fossimo stati nemmeno capaci di realizzare quel minimo di collaborazione tra maggioranza e opposizione che è necessario per far funzionare il nostro Senato, questo vorrebbe dire che intendiamo prolungare condizioni di insicurezza del nostro Paese, moltiplicare le sue fragilità, promuoverne promuoverne e non curarne i malesseri. Mi rivolgo, quindi, in primo luogo a tutti i senatori e a tutti i deputati, ma voglio indirizzarmi personalmente anche al capo della maggioranza, al primo ministro Romano Prodi, e al capo dell'opposizione, all'onorevole Silvio Berlusconi, perché soltanto se noi, senatori e deputati, e i due *leader* Prodi e Berlusconi riusciremo e riusciranno loro a parlare senza pregiudizi e strumentalità, solo se sapremo occuparci di più del bene comune, sarà possibile cambiare il modo con il quale maggioranza e opposizione stanno oggi svolgendo il loro lavoro politico. Silvio Berlusconi in particolare - è assente da quest'Aula perché è deputato, ma lo voglio nominare - può fare molto per cambiare il clima politico italiano e paradossalmente può farlo oggi più da capo dell'opposizione di quanto lo abbia fatto da capo del Governo, quando la sua azione era condizionata dal ruolo che svolgeva, assillata dal contesto, frenata dalle esigenze degli alleati. Oggi l'Italia non ha bisogno né di pasticci politici, né di compromessi disonorevoli; anzi, oggi più che mai è necessario oggi più che mai è necessario che maggioranza e opposizione tengano con chiarezza i rispettivi campi. Ma l'Italia, se non vuole perdersi, ha bisogno assoluto che quando sono in gioco l'interesse nazionale e il futuro del Paese, maggioranza e opposizione, sindacati e imprenditori, laici e cattolici cessino le guerre di posizione, abbandonino la tecnica del veto reciproco, dimentichino gli anatemi e sappiano dimostrare di sapere

quando ricordava: «Questo Paese non si salverà e la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera, se non crescerà un nuovo senso del dovere». Onorevoli senatori, se oggi Aldo Moro fosse qui tra noi, ci inviterebbe a riflettere sul fatto che il primo luogo dove dev'essere fatto prevalere il senso del dovere è proprio il Parlamento, è proprio il Senato*.

delle finanze*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ho ascoltato con attenzione chi ha preso la parola in questa giornata. Non tutto ciò che è stato detto è strettamente pertinente al tema. Non lo sono le preoccupazioni espresse in discussione generale e presentatemi anche personalmente dal Gruppo Per le Autonomie per la pressione fiscale e gli oneri burocratici nei confronti delle piccole e medie imprese. È un tema all'attenzione del Governo, sul quale sarò pronto a un approfondimento. Ma qui ora cercherò di rendere conto degli atti compiuti da me e dal Governo nella vicenda che riguarda i vertici della Guardia di finanza e i rapporti tra questi e il Governo della Repubblica nella persona del vice ministro Vincenzo Visco. Al Consiglio dei ministri, riunitosi d'urgenza il 1° giugno scorso, ho proposto la sostituzione del comandante generale della Guardia di finanza, ben consapevole della responsabilità che mi assumevo compiendo un sì grave passo. Ho esposto i motivi che mi inducevano a compierlo. Di concerto con il Ministro della difesa, ho proposto che nuovo comandante generale fosse nominato il generale di Corpo d'armata Cosimo D'Arrigo, in sostituzione del comandante generale Roberto Speciale. Il Consiglio dei ministri ha deliberato conformemente alla mia proposta. Nella stessa riunione ho sottoposto al Consiglio dei ministri...

e delle finanze. ...*aderendo a una richiesta dell'interessato, riprendevo nelle mie mani la responsabilità della Guardia di finanza.

dell'esempio che il Senato della Repubblica può e deve dare, per la sua grande responsabilità, sempre, tanto più quando ci raccordiamo direttamente con i nostri elettori.

finanze*. Presidente, gli italiani non sanno che ho ascoltato tutto quello che è stato detto nel corso di tutta la giornata seduto in questa sedia.

Signor Presidente, vorrei fare una premessa.

L'obiettivo dominante del mio comportamento in questa delicatissima circostanza è stato restituire serenità e fiducia al Corpo della Guardia di finanza. Ho servito io stesso nelle Forze armate e so quanto essenziale sia per chiunque ne faccia parte, senza distinzione di grado, la sicurezza dell'ordine a cui appartiene e la certezza di avere superiori sul cui corretto comportamento non possa nutrire dubbi. Altrettanto essenziale è una piena consapevolezza del rapporto corretto che deve esistere tra ordine militare e ordine politico. Quell'obiettivo dominante assume, nel caso della Guardia di finanza, una rilevanza particolarissima, perché essa non è un corpo che opera in tempi di pace per prepararsi all'eventualità che le pace possa venire meno. No, essa è un corpo militare impegnato qui e oggi in una difesa attiva contro chi compie illeciti e delitti di natura finanziaria, primo tra questi l'evasione fiscale. È dunque nelle condizioni tipiche di una forza combattente, bisognosa di un sovrappiù di certezza morale e di fiducia, senza le quali è impossibile battersi. Dal momento in cui un anno fa assunsi la responsabilità di Ministro dell'economia e delle finanze, ho sempre assunto quale criterio di partenza il migliore utilizzo possibile delle situazioni ereditate. La continuità delle istituzioni è un bene prezioso. Sulla base di questo criterio ho affrontato le situazioni dell'Alitalia, della RAI, dei dipartimenti del mio Ministero Ho deciso di intervenire quando mi sono convinto che il buon governo imponesse di correggere situazioni divenute ormai insostenibili. Con questo animo ho affrontato la vicenda della Guardia di finanza. Affronterò ora due questioni: in primo luogo, la legittimità del potere che l'Esecutivo ha usato; luogo, il ricorrere delle condizioni di fatto che hanno reso indifferibile esercitarlo. Sulla prima questione ricordo che la nomina di un nuovo comandante generale della Guardia di finanza e la contestuale revoca di quello in carica sono espressione di un potere del tutto legittimo in mano al Governo della Repubblica. Su questo punto sono concordi anni e anni di dottrina e di giurisprudenza. La nomina, come anche il mantenimento nella carica del comandante generale - ma lo stesso principio vale per tutti i vertici delle istituzioni militari e civili -, è qualificata come una decisione, e quindi un atto, di altissima amministrazione da assumersi in base ad una molteplicità di criteri che devono tutti ed ineludibilmente tendere all'obiettivo di garantire il perseguimento dei principi costituzionali che impongono il buono e corretto andamento della pubblica amministrazione. In linea generale, il buon andamento dell'amministrazione dello Stato si realizza concretamente allorquando, all'unisono, professionalità, assoluto rispetto dei ruoli e delle regole, inflessibile autonomia di azione nell'ambito di dette regole, serena e costruttiva dialettica istituzionale nell'alveo delle rispettive competenze, non disgiunta da impeccabile stile comportamentale, si riscontrano nei soggetti chiamati al rispetto e all'attuazione dei citati principi e della nostra Carta costituzionale. Laddove l'assenza o anche la carenza di uno solo dei requisiti personali ed oggettivi che ho appena richiamato possa sostanzialmente pregiudicare la funzionalità di una branca dell'amministrazione dello Stato, non credo si possa disconoscere la legittimità e l'opportunità di un intervento risolutivo ed adeguato, per quanto incisivo esso possa essere. Se poi innestiamo tali comportamenti e tali considerazioni sulla vicenda di cui ci stiamo interessando, non ho dubbi né perplessità sulla fondatezza sostanziale e formale dei provvedimenti da me proposti ed assunti all'unanimità dal Governo. Nel caso specifico, l'atto di nomina è caduto su un soggetto di indiscussa competenza e professionalità. La riunificazione in un unico contesto della revoca e della nomina configura una struttura provvedimentale binaria ben nota alla dottrina e alla prassi amministrativa. Nella sostanza, come chiarirò nel seguito, si è realizzata una discrasia permanente tra l'esercizio della funzione di direttiva e di indirizzo intestata all'autorità di Governo e le funzioni di gestione e di organizzazione intestate al vertice militare. Questa situazione doveva essere corretta d'urgenza per restituire piena funzionalità al corpo della Guardia di finanza. Passo ora alla seconda questione, per esporre i profili salienti che a giudizio mio e del Governo hanno reso inevitabile l'esercizio del potere legittimo che ho ora descritto. Esaminando con attenzione tutti gli elementi che ho potuto ottenere, ho rilevato gravi manchevolezze su due piani: i rapporti tra Comandante della Guardia di finanza e potere politico, e l'esercizio del comando all'interno del Corpo. In primo luogo, manchevolezze nei rapporti tra il comando di un corpo e l'autorità di Governo. Tutta la vicenda è stata caratterizzata dall'assenza di una comunicazione serena e cooperativa, da mancanza di trasparenza, di prudenza, di riservatezza, oltre che da quel venir meno alle regole...

e delle finanze*. Tutta la vicenda è stata caratterizzata dall'assenza di una comunicazione serena e cooperativa, da mancanza di trasparenza, di prudenza di riservatezza, oltre che da quel venir meno alle regole etiche e deontologiche che si chiama omissione. Una continua distorsione di regole e procedure ha finito per deformare l'autonomia, che è indubbia prerogativa del corpo, in qualcosa di diverso che chiamerei separatezza, quasi che fosse venuto meno l'essenziale legame tra autorità di Governo e vertice del corpo al servizio dello Stato. Gli inviti del potere politico ad usare prudenza e a non sconvolgere regole consolidate dall'uso sono stati definiti minacce o abusi d'ufficio.

Ma minacce non erano, il che spiega perché non siano state prese sul serio dalla stessa procura generale nella dichiarazione resa pubblica dal procuratore generale di Milano, dottor Mario Blandini, il 23 maggio 2007. In quest'ordine di mancanze va inserito l'episodio chiave della vicenda. Il 26 giugno 2006 il comandante generale proponeva una serie di nomine che coinvolgevano un vasto numero di sedi, ma faceva eccezione per Milano, presso la quale vi erano peraltro alcune permanenze di alti ufficiali più lunghe della media. Il 13 luglio 2006 il vice ministro Visco, dopo aver sentito anche i due ufficiali generali più anziani del Corpo per avere maggiori elementi di informazione, faceva presente al generale Speciale una duplice esigenza: primo, rendere più armonico il proposto piano di impieghi degli ufficiali prendendo in considerazione anche la sede di Milano, ovvero operando un ridimensionamento del piano stesso; secondo, ristabilire la giusta armonia anche all'interno del Corpo coinvolgendo il Consiglio superiore e comunque le cariche di vertice che affiancano il comandante generale nella sua azione di comando laddove sono in discussione le decisioni di maggiore rilevanza. Risulta in modo chiaro che il generale Speciale non ha mai riferito al Vice Ministro che il procuratore di Milano, con lettera del 1° giugno, aveva auspicato, nell'interesse di indagini in corso, la continuità dell'azione di comando di due colonnelli soggetti ad avvicendamento. Emerge dai documenti in modo obiettivo che il Vice Ministro non ha mai imposto alcun provvedimento *(Ilarità viceversa, nell'esercizio dei suoi legittimi poteri di direttiva ha prospettato l'opportunità di coinvolgere anche la sede di Milano negli avvicendamenti proposti e sul piano del metodo ha consigliato di seguire la prassi, cioè di consultare il Consiglio superiore. *(Commenti del senatore Storace)*. Il complesso di questi fatti dimostra un comportamento reticente e non cooperativo nei confronti dell'autorità di Governo. Il rapporto tra Corpo della guardia di finanza e autorità di Governo è stato dunque guastato anche da mancanza di collaborazione, comunicazione e trasparenza da parte del comandante generale. *(Commenti Subito dopo che tra il comandante generale e il vice ministro Visco si erano definite le linee guida per gli avvicendamenti alla Guardia di finanza di Milano, il comandante generale interrompeva la procedura che lui stesso aveva iniziato comportandosi come se quella procedura non esistesse: di sua iniziativa e rompendo ogni comunicazione imboccava per proprio conto ed in segreto una strada del tutto imprevista. *(Commenti del senatore Collino)*. Il 14 luglio veniva avviata in apparente consenso la procedura di trasferimento degli ufficiali di Milano;

A partire da questo momento la stampa diventa il canale attraverso il quale filtrano tutte le vicende che riguardano il comandante generale mediante la pubblicazione di lettere e note ricevute o indirizzate alle autorità, compreso il Vice ministro. Infine, la condotta del comandante generale nei confronti del Vice ministro è stata segnata da una mancanza di riservatezza molto grave. *(Commenti dai È inqualificabile che le telefonate tra il comandante e il Vice Ministro fossero fatte ascoltare con il sistema del vivavoce da due collaboratori del generale: il colonnello Carbone e il maggiore Cosentino. Va detta qui una parola chiara sul preteso nesso tra il caso UNIPOL e questa vicenda. Contrariamente a quanto cerca di far credere una campagna di stampa in corso da circa un anno, il nesso manca di ogni riscontro. Che gli instancabili corifei di questa tesi non abbiano saputo a tutt'oggi citare un solo fatto a sostegno del loro canto è di per sé una forte ragione per pensare che il nesso con UNIPOL sia inesistente. Se vi sono prove in contrario le si producano, le esaminerò senza pregiudizio. Concludo. La giusta autonomia del Comandante generale è degenerata in separatezza.

Mentre sulla scena ci si comporta in un modo, dietro le quinte si annodano rapporti con la magistratura e con la stampa. Il secondo ordine di manchevolezze riguarda l'esercizio del comando all'interno del Corpo. Norme e prassi di correttezza sono state non di rado disattese, con conseguente sconcerto dei comandi e perdita di autorità, anche morale, verso i collaboratori più stretti e i subordinati.

Il secondo ordine di manchevolezze riguarda l'esercizio del comando all'interno del Corpo. Norme e prassi di correttezza sono state non di rado disattese, con conseguente sconcerto dei comandi e perdita di autorità, anche morale, verso i collaboratori più stretti e i subordinati. gennaio 1999 n. 34 «il Comandante generale si avvale del Consiglio superiore della Guardia di finanza per le questioni di rilevanza strategica concernenti l'organizzazione, il personale, le operazioni e la pianificazione, a medio e lungo termine, per l'acquisizione e l'impiego delle risorse. Il Comandante generale, invece, non ha consultato in modo costante e sistematico il Consiglio superiore

Entro il Corpo erano notati, con dispiacere, il non puntuale rispetto delle regole e la mancata valutazione degli effetti giuridici delle decisioni prese.

che separa il Comando dal Corpo, che viene meno ai criteri della lealtà e della trasparenza. Quel che è apparso chiaro al Governo è che esistevano, dentro al Corpo e nei suoi alti gradi, sconcerto, profondo malumore, malessere, aspri contrasti. Stati d'animo e giudizi che derivavano da precise mancanze in quella che, a giusto titolo, si chiama arte del comando, opacità dei comportamenti, gestione personalistica e anomala per quanto riguarda gli ufficiali dell'area dirigenziale

e delle finanze*. In questo contesto va considerata la valutazione condivisa dai generali Pappa e Favaro di una gestione complessivamente personalistica del Corpo nella quale si evidenziava una politica dei riconoscimenti e degli encomi attuata spesso senza rispettare le procedure e con una pubblicità interna parziale e limitata. e limitata. Va segnalato che l'aiutante di campo del generale Speciale ha ricevuto un numero enorme di encomi solenni nonostante il fatto che sul suo capo penda una richiesta di rinvio a giudizio per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, peculato e soppressione, distruzione e occultamento di atti.

Al senatore Vegas offro una citazione altrettanto illuminante di quella che egli mi ha gentilmente offerto stamani. Dice Eraclito: «Combattere a difesa della legge è necessario per il popolo proprio come a difesa delle mura». Ritengo di avere combattuto a difesa della legge affinché la difesa della mura continui a svolgersi nel modo migliore. In democrazia la priorità del potere politico rispetto alle gerarchie civili e militari è un dato costitutivo. Naturalmente questo non significa entrare nel concreto dell'attività operativa dei funzionari e degli alti ufficiali che devono mantenere la loro autonomia, ma il prefetto non rimane al suo posto neppure un giorno se il Ministro dell'interno provvede a sostituirlo. E in guerra come in pace può essere sostituito un comando militare: McArthur fu sostituito in Corea da Truman in piena guerra. Là dove sono i funzionari, i generali o i colonnelli

accoglie l'ordine del giorno G11, a firma dei Capigruppo della maggioranza, mentre invita i presentatori degli altri ordini del giorno a ritirarli; diversamente il parere è contrario.

il Ministro ci leggesse, la copia del decreto del Presidente della Repubblica inviato alla Corte dei conti. Quelle che ha riferito sono state valutazioni di carattere politico. Vogliamo vedere le carte, se è possibile.

Da una parte, mi pare chiaro che ci sia un forte interesse a mettere in difficoltà il Ministro che ha il compito di combattere l'evasione fiscale. Ciò mi sembra tanto più grave quando gli ultimi dati parlano per il 2006 di una evasione fiscale e contributiva di oltre 125 miliardi e quando l'Agenzia delle entrate ci dice che il 95 per cento dei contribuenti visitati e controllati risulta non essere in regola col fisco.

Credo anche, tuttavia, che rimangano molti punti interrogativi sull'insieme di queste vicende e - ritengo sia opinione di molti - che avranno ulteriori risvolti politici. Non credo tanto a uno scontro tra poteri occulti di cui hanno parlato i giornali; vedo più concretamente uno scontro tra poteri economici e finanziari e relative cordate politiche che riguardano molte forze, comprese alcune dell'attuale maggioranza; vedo concreti processi dentro i quali si ridisegnano i poteri nella società capitalista. La mozione di apprezzamento dell'operato della Guardia di finanza, proposta dalla maggioranza e che voterò, mi sembra quindi debole, perché funzionale solo a rintuzzare, anche se va fatto, 1'attacco del tutto strumentale e scomposto della destra. Assai più significativa sarebbe stata una discussione sul riordino degli apparati in cui affrontare ad esempio il problema della smilitarizzazione proprio della Guardia di finanza, ma anche una discussione sugli altri apparati di sicurezza, i cui vertici -come quelli della Polizia di Stato - saranno rinnovati a giorni nel più totale silenzio e nella più disinvolta quanto inquietante continuità. *(Applausi della

il caso Visco - così ne parlano ormai tutte le testate giornalistiche e i *media* nazionali - è scoppiato con tale forza da avvelenare, costi quel che costi, il clima politico del nostro Paese. Abbiamo ascoltato ieri su tutti i telegiornali le irresponsabili dichiarazioni del capo dell'opposizione (che si è visto poi costretto a ridimensionare), che ha minacciato azioni contro lo Stato, ancor più gravi se consideriamo che vengono da un ex Presidente del Consiglio che aspira a tornare alla guida del Paese. A ben guardare, vi è caso e caso: un conto è, infatti, la vicenda del Vice ministro dell'economia, conclusasi con la restituzione della delega sulla Guardia di finanza. Ben altro conto sono, invece, l'attacco strumentale, la tempesta di parole spudorate e le polemiche scatenate dall'opposizione, all'unico scopo di montare nel caos mediatico di giornali e una contrapposizione fra istituzioni dello Stato: un tentativo squallido di creare i presupposti per incrinare il rapporto di fiducia tra Governo e Guardia di finanza; un tentativo di bassa politica di giocare con le istituzioni ed il senso dello Stato; un'operazione del centro‑destra maldestra e grossolana, nella quale abbiamo sentito l'ex ministro Tremonti rimproverare al Governo Prodi di varare provvedimenti *ad personam* *ad personam* e Berlusconi rispolverare antichi pallini, come il riconteggio delle schede elettorali o accusare - lui, proprio lui! - il centro-sinistra di conflitti d'interesse. Cari colleghi, tornando con i piedi per terra, bene ha fatto il nostro Segretario e ministro della giustizia Clemente Mastella a richiedere un documento di apprezzamento e di solidarietà alla Guardia di finanza, che restituisca serenità e tranquillità al Corpo, che - lo sottolineo - è e deve restare un'istituzione *super partes*, che va garantita da ingerenze e soggezioni a fatti di tipo politico. Se un merito può essere ascritto a tutta questa vicenda è, semmai, quello di aver reso evidente a tutti la necessità che al vertice della Guardia di finanza - come già avviene per i Carabinieri - sia scelto, in futuro, un generale proveniente dai quadri della Guardia di finanza Siamo qui, cari colleghi, per un ordine del giorno che è stato sottoscritto da tutta la maggioranza e che va votato da tutta la maggioranza. Davanti alla pretestuose e strumentali manovre di un'opposizione che gioca allo sfascio dello Stato,

Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dinanzi al Paese, quest'oggi, vi è lo spettacolo di un potere definito dal generale Speciale con l'inquietante appellativo di regime, che non esita a commissariare il Comandante generale della Guardia di finanza e, quindi, a coprirlo di infamie dopo 46 anni di onoratissima carriera militare al servizio del Paese. è un metodo, noto a molti, tra cui al generale Speciale ma anche al generale Pollari, che utilizza quotidianamente l'aggressione dell'avversario come sistema e perfino la strategia del complotto come elemento inquietante per allargare un confronto politico privo di argomenti che non siano l'arroganza e la prevaricazione. La vicenda di cui ci occupiamo oggi, signor Presidente, è chiarissima: bisognava avvicendare alcuni ufficiali di grado dirigenziale a Milano per azzerare un'intera catena investigativa. Una sola domanda andrebbe rivolta al vice ministro Visco, ed è questa: egli sostiene di avere operato in forza delle proprie deleghe sulla Guardia di finanza riguardanti il reimpiego di ufficiali in grado dirigenziale, generali e colonnelli. Ebbene, signor Ministro dell'economia, oltre all'indebita ingerenza che, secondo la ricostruzione del generale Speciale, tendeva a commissariarlo, come giustifica l'anomalia legata al fatto indiscutibile che tra le immotivate richieste di trasferimento veniva ricompresa quella del tenente colonnello Vincenzo Tomei, Comandante del gruppo Servizi di polizia giudiziaria del nucleo di Milano, che, rivestendo un grado non dirigenziale, non doveva né poteva essere comunque considerato nella procedura riguardante l'impiego dei dirigenti? Si trattava, signor Ministro, di dirigenti presenti in servizio da meno di un anno e, per il generale Forchetti, da appena tredici mesi: erano forse indegni? O lo era - e lo è - il generale Speciale, cui nessuno - ripeto, nessuno - ha fornito uno straccio di motivazione rispetto al proprio richiesto avvicendamento? «Denuncio la volontà di esautorarmi dalle mie precipue, potestà e responsabilità», ha scritto il generale Speciale; è questa la verità a cui credo e crederò fino alla fine di questa vergognosa vicenda.

dire agli italiani che non sempre lavoriamo nelle condizioni in cui ci hanno costretto a farlo stasera. Stiano tranquilli, il Senato è capace di ben altre discussioni e con altre modalità. *(Commenti dai banchi dell'opposizione).*

Noi quella mozione non la voteremo e voglio spiegare i motivi per i quali ci orientiamo in questa direzione; in quella mozione c'è un processo già celebrato e una sentenza già emessa. A noi non sta a cuore - così come è avvenuto e si è visto - precostituire giudizi negativi sui rappresentanti del Governo, sta a cuore, invece, quando temiamo che l'imparzialità non sia più salvaguardata, fare quello che abbiamo fatto nei giorni scorsi come Italia dei Valori. Valori. Nel momento in cui due pezzi importanti dello Stato dicevano cose diverse ed ambedue, a cominciare dal vice ministro Visco, mantenevano le funzioni, bisognava ricostruire e ricostituire la la regola fondamentale sulla quale uno Stato si regge e si governa bene: l'imparzialità della pubblica amministrazione. Noi, quindi, non siamo per una condanna preconcetta per il vice ministro Visco, siamo però - e ringraziamo il Governo per averlo realizzato venerdì venerdì - per il fatto che fino a quando le circostanze non saranno tutte conosciute nella loro entità, sia in punto politico, sia sotto l'aspetto di altre autorità che stanno indagando, quella delega - solo e soltanto la delega relativa alla Guardia di finanza

Chi ha il coraggio di mettere in piazza subito le ragioni, se le ha, e ha il coraggio di privarsi di una funzione sovraordinata, laddove venga messa in discussione la propria imparzialità, esce sempre bene e forte quando questa sarà stabilita in altre sedi. Credo che venerdì questo il Consiglio dei ministri l'abbia fatto e noi dell'Italia dei Valori ci ritroviamo nella mozione di maggioranza che condivide l'operato del Consiglio dei ministri. Abbiamo restituito, signor Presidente e signori colleghi, l'imparzialità in una vicenda che ci faceva correre il rischio complessivamente, come Paese, come Nazione italiana, di essere poco credibili. Siamo soddisfatti di aver contribuito con il nostro ordine del giorno a determinare le condizioni per le quali c'è stato il dibattito che oggi abbiamo svolto in forme civili, con dovizia di particolari, per restituire credibilità alle istituzioni, al Senato, in primo luogo, ma anche al Governo, che ha avuto la capacità di adottare il provvedimento di venerdì scorso, ricostituendo l'imparzialità che è l'unico modo attraverso il quale noi, che esercitiamo una pubblica funzione, possiamo essere ritenuti classe dirigente dai cittadini. Questo è avvenuto e su di esso ci ritroviamo noi dell'Italia dei Valori con la mozione presentata dai Capigruppo di maggioranza. Oserei dire, signor Presidente, signor ministro Padoa-Schioppa, con oggi abbiamo dimostrato che la nostra maggioranza non è omertosa, riesce a parlare con chiarezza e a trasmettere. Ci rammarichiamo che ciò sia avvenuto un po' tardi, forse andava fatto un po' di tempo un po' di tempo fa; probabilmente non sarebbe montata una questione come quella che è montata negli ultimi giorni perché è legittimo per tutti sospettare perché è legittimo per tutti sospettare e avere dubbi, se non si dice con chiarezza il perché e il per come si è operato in un certo senso. Abbiamo appreso dalla sua relazione, signor Ministro, qual è stata la valutazione in sede di Consiglio dei ministri; lei ha fatto una distinzione tra autonomia e separatezza e ci ha posto come evidentemente creatasi una separatezza del Corpo o del Comandante del Corpo piuttosto che un'autonomia che gli è dovuta per legge. Pensiamo che il generale Speciale negli ultimi giorni abbiamo contribuito a svelenire il clima, rispetto alle prime dichiarazioni rese. E vi abbia contribuito dicendo «obbedisco », parola che da tempo non sentivamo nelle nostre discussioni e nel rapporto tra servitore dello Stato e lo Stato. Ci auguriamo e siamo convinti che abbiate visto giustamente: non si trattava più di autonomia, ma di separatezza per quello che avveniva. Siamo convinti che la scelta sia stata fatta in modo oculato. Siamo qui a sorreggervi nella vostra azione. Siamo qui unicamente - e concludo - a rammaricarci. La tempestività in democrazia non è una variabile. È una cosa importante.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo Per le Autonomie mi preme sottolineare, innanzitutto, la necessità che su questa vicenda sia fatta la più completa e celere chiarezza. Il ritiro della delega al vice ministro Visco è stato un segnale necessario e positivo da parte del Governo. Chiediamo fin d'ora che le competenze della Guardia di finanza siano conferite e rimangano definitivamente nelle mani del Ministro competente. Sulla vicenda è ora necessario che la procura della Repubblica faccia il proprio lavoro con serenità e che, qualora emergano aspetti non condivisibili, l'Esecutivo e lo stesso vice ministro Visco prendano le opportune decisioni. Ma questo caso non deve interferire sulle procedure e sul diritto del Governo, sancito dalla Costituzione, di scegliere il comandante della Guardia di finanza. L'ha fatto anche l'ex presidente Berlusconi ed è corretto che, quando viene a mancare il rapporto di fiducia, il comandante possa essere sostituito. Criticabili sono, invece, gli atteggiamenti intrusivi nelle nomine dei singoli riparti. Riteniamo, quindi, che se la destituzione del generale Speciale rientra nell'ambito dei diritti-doveri di un Ministro, la stessa non debba essere messa in discussione, anche se riteniamo che nell'intero caso vi sia stato un *deficit* di trasparenza. Se, al contrario, le scelte fossero state motivate da un voler interferire nelle indagini delle Fiamme gialle, tutto ciò apparirebbe come un fatto gravissimo. Dall'altra parte, il comandante della Guardia di finanza non deve usare la sua posizione come strumento politico. Lo stesso comandante non deve passare le linee ai giornali o fare telefonate in viva voce per poi usarle contro il Ministro. Un Ministro può essere censurato, ma devono esser usati i metodi previsti dalla legge. Al centro dell'attenzione mi permetta che in questo dibattito, diventato politico - in cui l'opposizione vuol far cadere il Governo - poniamo come Gruppo Per le Autonomie e chiediamo l'attenzione per misure nell'ambito della politica fiscale, urgente da affrontare. Premetto che condividiamo l'obiettivo di ridurre l'enorme debito pubblico ed il *deficit* finanziario per liberare risorse per la crescita. Ritengo, però, che la politica fiscale del Governo, a partire dalla rigorosa e pesante legge finanziaria, abbia messo troppo sotto torchio le piccole, medie e microimprese. Queste aziende sono parte essenziale del sistema produttivo e sono state chiamate a contribuire al rilancio dell'economia con aggravi fiscali spesso non più sostenibili. richiediamo, pertanto, ma per tutto il Paese - noi forse perché siamo più sensibili, legati al territorio di una economia molto prospera in Provincia di Bolzano, anche se ritengo che il problema sia nazionale - che nella prossima manovra finanziaria si tenga conto delle difficoltà delle piccole imprese, soprattutto artigiane e commerciali. Forti perplessità nascono, inoltre, nei metodi adottati dalla Guardia di finanza nei controlli. Condividiamo in pieno - su questo non c'è dubbio - la necessità di combattere con forza l'evasione fiscale, stimata da 200 miliardi di euro, ma nel contempo giudichiamo assai esecrabile che nelle sedi delle imprese si arrivi con i mitra spianati e con metodi vessatori, che creano difficoltà fanno insorgere malumori e paura non solo tra le piccole e medie imprese. Inoltre, tolgono ai giovani la voglia di fare impresa.

È di questa mattina la notizia che una azienda è stata chiusa dalla Guardia di finanza perché non aveva emesso scontrini per 59 euro. È stata chiusa perché momentaneamente non aveva la disponibilità della carta necessaria.

Nelle Regioni del Sud, in primo luogo, ma anche in quelle del Nord, lo sappiamo tutti, esiste un forte sommerso. Condividiamo l'obiettivo di un sistema più giusto, facendo pagare tutti e con meno aggravi, però i metodi non si trasformino in terrorismo fiscale. I cittadini vivono una forte incertezza perché il nostro sistema si basa esclusivamente su misure punitive e sanzionatorie. In altri Paesi europei, con risultati molto più efficienti, basta guardare l'Austria, la Germania e la Svizzera, gli organi competenti fanno soprattutto prevenzione e consulenza nei confronti delle piccole imprese, coinvolgendole in una cultura contributiva corretta. I titolari vengono ascoltati e con gli stessi vengono concordati incontri per verificare i libri contabili e capire dove ci possono essere deficienze, senza che in queste consultazioni vengano applicate sanzioni.

un metodo di prevenzione e consulenza che noi come Gruppo Per le Autonomie chiediamo venga adottato anche nel nostro Paese. Il Governo deve dotarsi di una politica di consulenza, accoppiandola ad una semplificazione delle procedure, per un fisco non persecutorio ma sempre più amichevole. Dobbiamo dare serenità e fiducia ai cittadini e queste due condizioni passano anche per un'adeguata politica fiscale. Il voto amministrativo al Nord è stato un campanello di allarme, rafforzato anche da quello che dice la gente, che invita tutti ad una svolta Credo che tali riflessioni siano necessarie in questa Aula visto che tale dibattito si è trasformato in un acceso scontro, in cui l'opposizione cerca di far cadere il Governo Prodi. Non riteniamo che una crisi di Governo in questo difficile momento sia la ricetta migliore per il nostro Paese. I cittadini infatti si aspettano una ripresa del Paese, riforme che sono però ostacolate dalla difficile situazione venutasi a creare proprio in questo ramo del Parlamento, frutto di una legge elettorale distorta, distorta, ma anche, signor Presidente e signor Ministro, e lo dico anche alla maggioranza, da un Governo e da una maggioranza poco coesi, che dovrebbero ritrovare una loro unità per il rilancio dell'economia, la lotta alle vecchie e nuove povertà, la riforma della previdenza e le liberalizzazioni. Accogliamo con soddisfazione, signor Ministro, le rassicurazioni che ella ha fornito rispetto alle preoccupazioni da noi espresse in merito alla pressione fiscale e agli oneri burocratici nei confronti delle piccole e medie imprese. manovra finanziaria - mi permetta il termine - lacrime e sangue, sono presenti i presupposti per il rilancio del Paese. Gli indici sono positivi, il PIL sta salendo, il *deficit* è già diminuito, è diminuita la disoccupazione e anche il tasso di inflazione. Dobbiamo sfruttare questa fase economica favorevole impegnandoci tutti insieme per il bene comune. È per questi motivi che il Gruppo Per le Autonomie non ritiene opportuno che si faccia cadere il Governo. Non sono utili in questa fase scontri di posizione, ma occorrono equilibrio e responsabilità che devono coinvolgere sia la maggioranza che l'opposizione, perché il teatro che abbiamo vissuto pochi minuti fa ha fatto di nuovo distaccare i cittadini da queste istituzioni in cui noi crediamo fortemente. Non è possibile fare un scenata simile davanti a tutto il Paese e dividere e dividere anche questo Parlamento e il Paese, che vuole riforme, vuole innovazione, vuole che il Governo possa finalmente agire, fatto impedito da simili dibattiti. dibattiti. Con le aspettative esposte, rafforzate dalle assicurazioni del Ministro di studiare e di volerci anche incontrare per ridurre il peso fiscale per le piccole e medie imprese

Signor Presidente, esprimiamo fiducia convinta e stima per il vice ministro Visco, sperando che la magistratura, nel più breve tempo possibile, stabilisca le responsabilità in capo a tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda torbida e velenosa. Riteniamo che Visco risulterà estraneo, riteniamo che il Vice ministro abbia avuto un comportamento ineccepibile, per quanto riguarda i rilievi di carattere giudiziario, istituzionale e politico. Esprimiamo fiducia e stima per la Guardia di finanza, per il ruolo importante che svolge contro l'evasione fiscale, per la prevenzione e per gli accertamenti fiscali, per il controllo delle frontiere contro il contrabbando e per la prevenzione dell'immigrazione clandestina. Non possiamo esprimere fiducia e stima per il generale Speciale, perché ha utilizzato un normale avvicendamento ai vertici della Guardia di finanza della Lombardia e di Milano per trasformarlo in un caso politico, in modo maldestro e irrispettoso nei confronti delle istituzioni. Ha lasciato le sue impronte digitali (ovviamente in modo metaforico) nella campagna de «il Giornale» costruita contro il vice ministro Visco; forse c'entrano qualcosa le iniziative e le norme adottate le norme adottate da questo Governo contro l'evasione fiscale e la campagna contro il Governo Prodi.

si è atteggiato a vittima, ha contestato la legittimità del provvedimento di trasferimento a suo carico, ha contestato il trasferimento alla Corte dei conti per poi ritornare indietro, quando la campagna si è sviluppata in quelle ore.

non è la politica che ha interferito, ma è il generale Speciale che ha influenzato e strumentalizzato un caso per trasformarlo in caso politico. Pensiamo che non solo avrebbe dovuto lasciare il suo incarico, ma il Governo avrebbe dovuto aprire un regolare processo disciplinare nei suoi confronti; il Governo avrebbe dovuto essere più presente e più rigoroso in questa vicenda. Si è aperto un conflitto tra istituzioni, sull'autonomia e sull'indipendenza del loro rapporto. Credo che bisognasse coinvolgere l'organo costituzionalmente competente, cioè la Consulta, altro che pressioni della politica sulla Guardia di finanza! È esattamente il contrario: è il comportamento del generale Speciale e dei suoi alti collaboratori che ha contribuito a determinare questa situazione. Per noi la vicenda potrebbe essere chiusa qui, anche perché la mozione della destra che chiedeva di revocare le deleghe al vice ministro Visco non ha più ragione di essere, perché le deleghe sono state sono state ritirate. Allora, perché questo dibattito? Credo che continui la strumentalizzazione politica sostenuta da una campagna di stampa-spazzatura odiosa e cattiva. Bisogna fermarsi, lo chiedo a tutti i Gruppi parlamentari; bisogna fermarsi, ma la destra vuole a tutti i costi la spallata che non arriverà. E allora si insiste su una strada avventurista e destabilizzante; si coinvolgono le più alte cariche dello Stato e lo stesso Presidente della Repubblica. Si dice che il Presidente della Repubblica è, Capo delle Forze armate dimenticando ovviamente non si dimentica, perché lo sapete benissimo - che ha per quanto riguarda la Guardia di finanza solo un ruolo di indirizzo e dimenticando che per quanto riguarda i rilievi di carattere politico la competenza è del Parlamento, non certo del Presidente della Repubblica e meno male meno male che è così. Nei regimi democratici è così. Forse, la destra si dimentica di queste cose e si dimentica che per quanto riguarda gli aspetti di carattere giudiziario la magistratura deve fare il suo corso. corso. Presidente, anche la destra conosce queste regole di base che attengono al funzionamento dei regimi democratici. Allora, perché si è tentato di coinvolgere il Presidente della Repubblica? Si utilizzano, ritengo, le istituzioni a fini politici; non si ha ritegno a chiamare in causa il Presidente della Repubblica; la destra mostra in questo caso, come in altri, ancora il suo DNA profondo, antistituzionale, populista ed intollerante nei confronti delle regole democratiche. C'è una verità che va al di là, Presidente, della cosiddetta vicenda UNIPOL. Credo che qui non c'entra niente il merito; forse non c'entra neanche il collegamento dei vertici della Guardia di finanza di Milano e della Lombardia con l'ex ministro Tremonti. A me pare che viene fuori una concezione della lotta politica barbara, oscura, astiosa e vendicativa. Probabilmente è vero che i rapporti tra il generale Speciale e il vice ministro Visco non erano buoni questo è innegabile - ma mi chiedo: con quale legittimità il generale Speciale ha deciso il trasferimento e la promozione di alte cariche della Guardia di finanza proprio nelle stesse ore nelle quali egli veniva spostato? Con quale legittimità e con quale autorità il generale Speciale protestò nel giugno scorso quando c'è stata la festa del corpo della Guardia di finanza perché aveva saputo che il vice ministro Visco avevo avuto l'incarico per il discorso ufficiale? Con quale autorità con quale legittimità si contesta il fatto che il potere politico svolga, nel modo più trasparente e legittimamente, le proprie funzioni? Ritengo che bisogna ritornare al rispetto delle regole, delle istituzioni, alla divisione dei ruoli e all'autonomia reciproca. La destra fa male a difendere Speciale ed a investire il Capo dello Stato.

Vogliamo che i cittadini conoscano tutti i fatti; vogliamo capire e giudicare e i cittadini vogliono capire e giudicare: capire chi ha qualcosa da nascondere, capire chi ha strumentalizzato e capire chi invece è un galantuomo ed è onesto.

Signor Presidente, anch'io signor Ministro, come lei, ho da fare una premessa per chiarezza: non siamo d'accordo su nessuna delle giustificazioni che lei ha portato per la rimozione del generale Speciale le dimostreremo anche perché. Siamo qui questa sera perché i Capigruppo della minoranza hanno sentito l'obbligo civile e morale di intervenire affinché il Governo si impegni a rispettare le procedure giuridiche e amministrative esistenti in tema di revoca e conferimento di incarichi pubblici. Ciò, all'orecchio del cittadino comune che ci sta ascoltando, peraltro, come del resto al nostro, ha sicuramente un suono strano: chiedere al Governo di rispettare la legge di cui egli stesso è garante è un paradosso, di cui solo l'attuale maggioranza può rendersi protagonista. Stiamo parlando dell'ormai ben nota quanto triste vicenda che ha visto coinvolto il vice ministro dell'economia Visco e il generale Speciale, rimosso dal suo incarico di comandante generale della Guardia di finanza. Noi, al contrario del Governo, vogliamo affrontare tale vicenda da un punto di vista prettamente legittimistico. Vogliamo infatti dimostrare come l'azione governativa di avvicendamento dei vertici della Guardia di finanza in questa occasione si sia rivelata assolutamente illegittima, secondo i principi del nostro diritto. Premesso il legame di dipendenza che lega, *ex* articolo 1 della legge n. 189 del 1959, il Corpo della Guardia di finanza Guardia di finanza al Ministro dell'economia, il quale legittima quest'ultimo ad esercitare i poteri di nomina e revoca del suddetto vertice; è però necessario porre l'accento sui limiti che connotano tale potestà. Prima di tutto bisogna ricollegarsi all'ormai consolidata dottrina che disgiunge gli atti prettamente politici dagli atti di alta amministrazione, ai quali anche lei, signor Ministro, ha fatto riferimento. È del tutto pacifico, infatti, che gli atti politici costituiscono l'espressione della libertà politica, connessa dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato, per soddisfare esigenze unitarie ed indivisibili

volere insistere su questo passaggio. Decisamente diverso è invece l'atto di alta amministrazione che come *species* del *genus* atto amministrativo espleta una funzione di raccordo tra funzione politica e funzione amministrativa e, pur essendo certamente caratterizzato da un'ampia discrezionalità, è sempre da considerarsi un atto amministrativo che, come tale, deve sottostare alle regole previste dalla legge che lo disciplinano. Una volta specificata tale classificazione, è possibile identificare la natura giuridica dell'atto di nomina e, di riflesso, quello di revoca, oggi in questione. Tali atti, infatti, sebbene nella disponibilità dell'organo governativo, non sono volti a esplicitarne i fini politici ma, essendo atti funzionali allo svolgimento di un'attività prettamente amministrativa, e come tale vincolata nel fine, debbono sottostare alle disposizioni in tema di procedimento amministrativo e quindi essere adeguatamente motivati a fronte di un contraddittorio tra le parti. Non vogliamo però addentrarci in un linguaggio troppo tecnico, adatto per lo più alle aule dei giuristi; vogliamo essere concreti perché i cittadini comprendano chiaramente che vi sono delle leggi che specificatamente regolano il procedimento amministrativo. Tali leggi sono state votate da questo Parlamento proprio per tutelare dei principi fondanti del nostro ordinamento quali la trasparenza e la legittimità della pubblica amministrazione. Tali leggi esistono proprio affinché non si possano verificare situazioni ambigue e imbarazzanti - oserei dire come queste in cui le censure di illegittimità non si limitano alla sola, anche se grave, violazione dell'obbligo di motivazione, ma suscitano non pochi dubbi in ordine alle molteplici vicende che hanno ruotato intorno a tutta la questione. Allora ci chiediamo: non sarà che queste motivazioni politiche vadano da noi ricercate presuntivamente in assenza totale di altri chiarimenti da parte del Governo nell'ambito delle indagini in corso a Milano, indagini a cui partecipano i valenti uomini, a detta della stessa procura milanese per iscritto, della Guardia di finanza, oggetto dell'imputato illegittimo trasferimento a cui Speciale si è opposto fermamente? Come è infatti possibile credere che sia solo un caso che i generali e i colonnelli della Guardia di finanza che Visco voleva sostituire facessero parte dalla catena di comando che si occupava della scalata UNIPOL su BNL? Come è possibile non pensare che si volesse posizionare degli uomini di fiducia in quei ruoli chiave, incontrando, per sua sfortuna, un ufficiale integerrimo che ha posto gli alti valori democratici del nostro Paese al di sopra delle illegittime pressioni provenienti da un Ministro,

un atto che non persegue certamente gli interessi pubblici di cui lo stesso deve essere istituzionalmente garante, un atto a cui tuttavia l'Esecutivo ha tentato di porre rimedio *in extremis* offrendo un'allettante poltrona alla propria vittima. Non è solo l'onorabilità di un alto funzionario dello Stato ad essere stata lesa o l'immagine di una carica importante del nostro Paese, come quella di Vice ministro. Sono stati messi in gioco, se possibile, valori ancora più elevati, come lo stesso principio democratico che infonde l'ordinamento del nostro Paese, come la credibilità delle sue istituzioni ed il ruolo svolto da tutte quelle norme che regolamentano i rapporti tra i poteri dello Stato. La nostra preoccupazione è alta. Un abuso di tali poteri potrebbe, infatti, costituire un pericoloso precedente per la vita della nostra Repubblica, per la sopravvivenza del nostro sistema democratico, così come previsto dalla Costituzione e dalle leggi che da essa derivano. Ora, noi comprendiamo, compatiamo quasi questo Governo che ogni settimana rischia di cadere per la sua cronica incapacità di costruire atti idonei a produrre benefici per questo Paese, ma mai potremo giustificare una azione illegittima, tanto in termini amministrativi quanto politici, utilizzata al fine di andare avanti purchessia, un comportamento così contraddittorio ed a tratti illogico di questo Governo, che lascia tutti noi ed i cittadini stessi, a dir poco spiazzati. Sarebbe, infatti, interessante capire come questo Governo può giustificare in modo ragionevole e coerente un provvedimento di alta amministrazione con cui rimuove il generale Speciale e, contemporaneamente, nominarlo consigliere della Corte dei conti, un ruolo di alto prestigio istituzionale. Insomma, se era da punire,

A sottolineare l'ipocrisia della vicenda è stato lo stesso "punito", il generale, rifiutando la promozione presso quella stessa Corte che non ha voluto o non ha potuto registrare l'atto di rimozione per la sua probabile illegittimità. Proprio Proprio questa mattina, l'autorevole collega Finocchiaro ha suggerito a tutti noi di non perderci in inutili cavilli giuridici e di fatto a prendere atto che siamo di fronte ad un atto politico. E allora? Dove troviamo scritto che un atto politico del Governo può essere illegittimo? In questo giunge in nostro "soccorso" un altro esimio collega, il senatore Cossiga, il quale ci richiama due famosi precedenti; quello del generale De Lorenzo e quello del generale Ciglieri. Vorrei far presente come le vicende in questione siano non solo assolutamente inconfrontabili, ma distanti come il giorno e la notte: la notte di De Lorenzo ed il giorno del generale Roberto Speciale. In questa vicenda, non siamo di fronte ad anni bui che richiedono di mettere in campo scelte difficili da giustificare, ma al contrario, oggi, per tutelare quanto costituito, si richiede e si pretende trasparenza e chiarezza. Le incongruità sono tipiche di questa maggioranza. Molti autorevoli esponenti della stessa - mi riferisco a Bertinotti, a Di Pietro e a Mastella - hanno chiaramente manifestato disapprovazione per l'intera vicenda e per il comportamento del vice ministro Visco, ma daranno il proprio appoggio a questo Governo che non rispecchia più nessun valore e tantomeno la volontà dei cittadini. Il pubblico dei cittadini che ci ascolta questa volta, nonostante la pesantezza dei discorsi spesso pronunciati in quest'Aula (rinunciando a seguire la partita della nostra nazionale), sta sicuramente facendo il tifo nella speranza che questa sera, come è già accaduto altre volte in questi dodici mesi, il Governo delle contraddizioni non abbia la maggioranza politica richiesta dal Presidente della Repubblica e che, quindi, come promesso, quest'ultimo ne prenda finalmente atto. *(Applausi dai Gruppi DCA-PRI-MPA e FI).* Diciamo questo "con" gli italiani, ma soprattutto "per" gli italiani, poiché siamo fermamente convinti di essere interpreti di un sentimento diffuso

Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, come Presidente del nuovo Gruppo parlamentare Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo ho sottoscritto l'ordine del giorno della maggioranza e i dodici senatori del nostro Gruppo lo voteranno. Consideriamo questo voto alla stregua di un atto di fiducia che ci viene chiesto dal Governo. Siamo convinti che questa maggioranza e questo Presidente del Consiglio devono adempiere per l'intera legislatura al mandato che è stato conferito dagli elettori e per questo compiamo un atto di coerente e leale sostegno al Governo. Il nostro giudizio sulla vicenda, collimante con quello testé formulato dal ministro Padoa-Schioppa, è stato espresso nel suo intervento dal senatore Paolo Brutti. semmai da domandarsi, come ha già fatto il senatore Paolo Brutti, tale essendo il giudizio del Governo, se fosse opportuna la destinazione del generale Speciale alla Corte dei conti. È questa anche l'occasione per ribadire la nostra solidarietà e il nostro sostegno alle Forze armate e alla Guardia di finanza, come ha fatto la senatrice Silvana Pisa a nome di Sinistra Democratica: migliaia di persone che si impegnano con grande professionalità, a volte a rischio della vita, per assicurare la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità, a cominciare da quella tributaria (altro che sciopero fiscale: l'onorevole Berlusconi si deve rassegnare a pagare le tasse come tutti i cittadini). Attenzione, però, questa vicenda si svolge nel contesto di una situazione di crisi nel rapporto tra la nostra maggioranza, il nostro Governo e larghi e crescenti strati della società italiana e dell'opinione pubblica; questa vicenda però si svolge anche nel contesto di una più generale crisi di credibilità del rapporto tra la politica nel suo insieme e i cittadini. Si aggiunge, in queste ore, un flusso di veleni, di insinuazioni, di annunci di torbide vicende. Signori del Governo, occorre reagire, e subito. Le strumentalizzazioni fuori di luogo e i toni esagitati del centro-destra - ai quali abbiamo assistito anche poco fa in quest'Aula - rischiano di accrescere il dissenso e la critica nei confronti della politica in generale. C'è un'antipolitica crescente nel Paese, che rischia di determinare, essa sì, una vera emergenza democratica. L'emergenza democratica c'è se si diffonde e consolida l'idea che le istituzioni rappresentative e le forze politiche, tutte, di destra e di sinistra, non sono in grado, prima ancora che di dare una risposta, di ascoltare la protesta che cresce. La risposta non può essere quella di cedere alle suggestioni di Governi extraparlamentari, di soluzioni estranee al sistema delle forze politiche, le quali si misurano sul voto dei cittadini. La risposta all'antipolitica sta nella buona politica: una politica diversa - per intendersi - da quella che appare in televisione tutte le sere. La buona politica è possibile, lo constatiamo noi della Sinistra Democratica con la straordinaria ed entusiastica partecipazione di giovani, di donne, di lavoratori alle iniziative che stiamo svolgendo in tutta Italia per dare vita al nostro nuovo movimento. C'è una grande domanda di partecipazione in Italia; c'è una grande richiesta di un'altra e buona politica, una politica che affronti con i cittadini quelle che per i cittadini, e non per il Palazzo, sono le vere questioni da affrontare e cercare di risolvere. C'è un profondo disagio sociale, particolarmente acuto nel Mezzogiorno, per le crescenti diseguaglianze, per il precariato, per le differenze in termini di reddito e di dignità sociale che si accompagna all'insoddisfazione manifestata dal ceto medio produttivo soprattutto del Nord Italia. E poi c'è un'altra grande questione aperta in Italia: la nuova questione morale. A cosa assistono i cittadini? Ad esempio, al silenzio di fronte all'accusa rivolta al Governo dal quotidiano «la Repubblica», che parla di connivenze con un'ipotizzata nuova P2. Davanti ad un'accusa cosi grave e inquietante non si può tacere: una risposta deve essere data. Ne ha parlato il senatore Massimo Villone, con parole in cui ci riconosciamo. E ancora: i cittadini ci sentono parlare di ridurre le loro pensioni, mentre noi parlamentari continuiamo a usufruire di ingiustificati privilegi pensionistici. E ancora i cittadini vedono che davanti ai costi abnormi e agli sprechi della politica - finalmente diventati un tema al centro dell'attenzione - invece di fare qualcosa di concreto, è in corso un assurdo rimpallo tra Governo, Regioni e Comuni su chi debba cominciare a tagliare per primo. Sinistra Democratica, con questo mio intervento, chiede al Governo alcuni atti precisi e concreti per segnare un'inversione di tendenza che consenta di recuperare il consenso perduto e di rilanciare l'azione del Governo Prodi. In primo luogo, chiediamo la coerenza con il programma elettorale. Il primo atto della riforma della politica è non rinnegare, quando si è al Governo, ciò che si è promesso agli elettori. Siamo ben consapevoli, essendo forza di Governo, della necessità di fare i conti con gli equilibri finanziari e con il debito pubblico, ma non possiamo dare l'impressione di avere, da un giorno all'altro, cambiato l'ordine delle priorità indicate dal cittadino nel momento in cui si è chiesto il suo voto. Anche da qui nasce l'antipolitica, dalla sensazione di un tradimento tra ciò che si detto prima e ciò che si fa poi. In secondo luogo, chiediamo al nostro Governo di bloccare il flusso dei veleni. Per bloccare il flusso dei veleni c'é un solo metodo: totale e assoluta trasparenza. Trasparenza, non segreti. È confermato oggi che nell'ambito delle indagini condotte dalla procura di Milano sul sequestro di Abu Omar è stato sequestrato un *dossier* redatto dall'ex funzionario dei Servizi Pio Pompa, un *dossier* illegale che viene indicato come finalizzato all'obiettivo dell'aggressione e della diffamazione di magistrati, giornalisti ed esponenti politici. Sull'indagine che riguarda anche questo *dossier* il Governo ha posto il segreto di Stato. Chiediamo al Governo di ritirare il segreto di Stato sulla vicenda Abu Omar e di ritirare il ricorso avanzato alla Corte costituzionale contro la Procura della Repubblica di Milano. Chiediamo al nostro Governo di fare pulizia: è vero o no quello che scrive "la Repubblica", che quello stesso Pio Pompa di cui si parlava svolge le funzioni di dirigente del personale presso il Ministero della difesa? E se è vero, è sostenibile questa situazione? Non va egli stesso immediatamente rimosso? In terzo luogo, chiediamo di affrontare con determinazione il tema dei costi abnormi e degli sprechi della politica. Dobbiamo cominciare a farlo dal centro, dal Governo e dal Parlamento. Ministro Santagata, nessun Governo formato da 102 persone può avere la credibilità per chiedere agli altri soggetti istituzionali gli indispensabili tagli e riduzioni negli scandalosi sprechi e la riduzione drastica dell'esercito di quasi mezzo milione di persone che oggi in Italia vivono di politica e intorno alla politica. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC e LNP).* Sinistra Democratica, con questo mio intervento, chiede al Presidente del Consiglio - come abbiamo già fatto negli incontri avuti con lui e con il ministro Chiti - un drastico snellimento della struttura di Governo. La Spagna prima e oggi anche la Francia dimostrano che un Governo può benissimo funzionare con quindici ministri, con un numero di donne pari a quello degli uomini, con pochi Sottosegretari. Il ministro Fabio Mussi ha già dichiarato pubblicamente e ufficialmente che è pronto a fare un passo indietro. Noi della Sinistra Democratica, che pure rappresentiamo la terza forza parlamentare della maggioranza, non chiediamo posti per noi: non nel Governo, non nei consigli di amministrazione, non nella RAI, ma chiediamo ad altre forze politiche non di fare come noi, ma almeno di sottoporsi ad una seria cura dimagrante (fa anche bene alla salute). Così come chiediamo a maggioranza e opposizione di avviare subito l'esame dei disegni di legge costituzionali per la riduzione del numero dei parlamentari. Sinistra Democratica propone di stabilirlo subito in 400 deputati e 200 senatori; poi sviscereremo la complessa questione del superamento del bicameralismo paritario. Solo partendo da noi, dal Governo e dal Parlamento tutto, avremo l'autorevolezza di chiedere agli altri soggetti istituzionali di fare la loro parte e anzitutto alle Regioni, che non possono pretendere di sottrarsi all'esigenza di moralizzazione della politica italiana in nome di un malinteso federalismo. Concludo. Per rilanciare la coazione in cui crediamo, per ridare serenità al Paese, per ritrovare una coesione sociale che rischia di perdersi, per restituire tranquillità alle istituzioni servono fatti politici: fatti nuovi, concreti e concludenti. questione morale e questione democratica sono oggi legate. Attenzione: rischiamo un'implosione del sistema. È mia ferma opinione che solo questa maggioranza politica è in grado di dare una risposta che eviti quell'implosione. Sinistra Democratica chiede concrete decisioni politiche ed istituzionali che parlino all'Italia e non al Palazzo, che ridiano a milioni e milioni di cittadini la fiducia e la speranza di una politica di segno nuovo, attenta ai problemi reali degli uomini e delle donne in carne ed ossa. Il nostro impegno a sostenere il Governo di centro-sinistra, con le nostre proposte, le nostre sollecitazioni e la nostra volontà unitaria, rimane fino in fondo a partire dal voto favorevole che ci accingiamo ad esprimere. Coraggio, amici del Governo, possiamo e dobbiamo dimostrare al Paese che meritiamo di governare. La Sinistra Democratica farà fino in fondo la sua parte.

attraverso la diretta televisiva, grazie alla quale oggi è possibile tornare all'*agorà*, luogo ideale ed insostituibile della democrazia diretta. Oggi si consuma una vicenda legata all'ennesimo atto di prevaricazione, di incapacità, di confusione e di dilettantismo con cui questo Governo sta calpestando le istituzioni e le buone prassi amministrative. La lista è lunga. Si è cominciato dalla notte delle elezioni in cui i *leader* dell'attuale Governo sono scesi in piazza e si sono autoproclamati vincitori delle elezioni stesse. Si è continuato con la totale occupazione di tutte le poltrone disponibili: le *Authority*, l'*Antitrust*, l'ANAS, la Cassa depositi e prestiti, le Ferrovie dello Stato, le attività portuali, gli enti cinematografici, l'Agenzia delle entrate. sottolineo l'operazione per la quale la sinistra ha eletto Segretario della Camera dei deputati un individuo condannato per terrorismo, con grave spregio dei sentimenti delle vittime. Prodi, in questa inesauribile sete di poltrone, ha nominato il Governo più numeroso della storia della Repubblica, com'è stato testé ricordato: 105 tra Ministri e Sottosegretari. Non contenti, nell'autunno del 2006, hanno fatto approvare una legge secondo la quale è possibile rimuovere anche i dirigenti di minore importanza al fine di sostituirli con persone gradite. Vorrei ricordare ai cittadini in ascolto che però, siccome neanche loro hanno avuto il coraggio di licenziare funzionari muniti di regolare contratto,

La vicenda di cui parliamo si inserisce in questo filone autoritario. Riesaminiamola brevemente per i cittadini che ci ascoltano. Nell'estate 2006 il vice ministro dell'economia e delle finanze Vincenzo Visco, in totale spregio delle leggi, delle prassi e delle consuetudini, è intervenuto sul comandante generale della Guardia di finanza Speciale, imponendogli con arroganza - come attestano le risultanze scritte e testimoniali - di sostituire tutti i vertici della Guardia di finanza lombarda; arrivato addirittura a minacciare Speciale, con una telefonata di cui ci sono i testimoni, di gravi conseguenze se non avesse ottemperato immediatamente ai suoi ordini. Allora, signor Ministro, inqualificabile non è la testimonianza dei generali, ma inqualificabile è la telefonata del vice ministro Visco! *(Applausi Allora, la domanda che ci si pone è una e inevitabile: perché Visco fa ciò? Perché c'è questa necessità assoluta di sostituire immediatamente i vertici lombardi?

frase lascia il re nudo e denuncia i traffici poco chiari, gli intrecci sotterranei che esistono tra la sinistra e la finanza rossa dimostrando che, al di là dei proclami moralistici, la sinistra non ha mai rinunciato a trafficare sul piano degli affari, con un'intollerabile commistione tra politica, interessi economici e finanziari. Vedo, signor Ministro, che lei china la testa, forse si vergogna di quello che sto dicendo. Ride, beato lei che ha da ridere, come Prodi; ridono sempre, chissà perché, nel Paese in cui sono ridono sempre. Cuor contento il ciel l'aiuta. Bisognava intervenire, dare una lezione agli ufficiali non allineati, occorreva occupare e normalizzare anche la Guardia di finanza. Visco però ha fatto molto male i suoi conti, ha trovato sulla sua strada un uomo con la schiena diritta, un soldato, un servitore dello Stato che non si è piegato alla vostra prepotenza politica! Quindi, non c'è stata nessuna rimozione immotivata per quanto riguarda gli ufficiali cui l'onorevole Visco aveva fatto

Per un anno tutto tace; anzi, affinché serva da lezione, il direttore dell'ANSA, che aveva osato dare per primo la notizia del contrasto tra Visco e la Guardia di finanza, viene licenziato in tronco;

due affermazioni gravissime. In prima battuta ha dichiarato che il generale Speciale ha usato la magistratura: dovrà tornare in quest'Aula a rendere conto di queste parole, signor Ministro,

se lei avesse ragione, il suo comportamento sarebbe ancora più grave, perché significherebbe che avete lasciato al suo posto, in una posizione di assoluta delicatezza e importanza, un alto ufficiale infedele e non rispettoso della Costituzione, in quanto non ha ottemperato alle direttive dell'autorità politica; non soltanto, ma gli avete proposto la promozione in un importantissimo ente come la Corte dei conti! Anche questo dovrà venire a spiegare in Aula: perché ad un ufficiale infedele avete proposto una promozione! Dovrà venire qui a spiegarcelo, signor Ministro.

Vede, signor Ministro, anch'io ho passato duri momenti, magari anche in Aule più turbolente di quella di stasera (lo sanno i colleghi che erano qui), siccome sono sempre stato convinto di essere nel giusto, sono sempre venuto a sostenere le mie idee guardando negli occhi i senatori: dov'è il vice ministro Visco? Perché è scappato? Perché non è qua a guardarci negli occhi?

Visco rimette momentaneamente le deleghe e a te Speciale, diamo la poltrona comoda sulla quale stare. Vi è andata male anche questa volta, perché avete trovato un uomo con la «U» maiuscola, che non ha accettato un compromesso di questa natura. e AN).* Credo che ormai la vostra protervia vada di pari passo con la vostra incapacità: state gettando nel caos il Paese e le istituzioni.

Grazie.

della questione. Ad esso farò riferimento tra qualche minuto, non prima, però, di averle ricordato il fatto che, molti anni fa, ebbi la fortuna di conoscerla in Banca d'Italia, quando era vice segretario generale, persona molto stimata di un'istituzione molto stimata, in un momento nel quale si temeva che vi fossero azioni giudiziarie non condivise nei confronti dei vertici di quella Banca. Mi

che non gradisce che il Governo della Repubblica insulti i rappresentanti del popolo. Ella, in questo momento, al Senato della Repubblica ha riferito cose che abbiamo grande difficoltà a ritenere, non dico vere, ma verosimili, per una ragione molto semplice.

Avete idea di cosa sia la Corte dei conti? Vi rendete conto che è un'istituzione dignitosa della nostra Repubblica e non una discarica in cui mandare tutte le fecce umane? Si rende conto, Ministro, che lei, attaccando Speciale (come ha fatto stasera), ha di fatto insultato politicamente la Corte dei conti in modo drammatico? Si rende conto che il popolo italiano, quale sa che questo è il Governo che ha messo le mani nelle tasche degli italiani, ragionevolmente aveva un vice ministro Visco che ha tentato di mettere le mani sulla Guardia di finanza? Questo è il problema che abbiamo di fronte a noi: la gente crede che Visco ha tentato di usare la Guardia di finanza per fini di parte. Ma si è chiesto, lei, perché c'è il vice ministro Visco, signor Ministro dell'economia? Ha capito perché in quel gigantesco assemblaggio di Ministri e Sottosegretari è stato messo accanto a lei,

senza successo fino ad ora - di avere il resoconto stenografico delle dichiarazioni del ministro Padoa-Schioppa al Senato: se risultasse vero ciò che mi sembra di aver ascoltato, pur nel clamore durante la dichiarazione del Ministro, che ha insultato il Senato della Repubblica, direi che non può il Governo insultare il Senato della Repubblica e il Presidente del Senato ha il dovere di difendere la dignità del Senato.

Se il resoconto stenografico risulterà riportare frasi del ministro Padoa-Schioppa di insulto al Senato della Repubblica, in questo caso avremo modo di avviare un nuovo dibattito insegnare al Ministro che esiste nel nostro sistema un rapporto tra Governo e Parlamento che non consente al Governo di insultare il Parlamento. Può darsi che il Ministro non lo sapesse, queste cose gliele spiegheremo, mica è una cosa difficile. Può darsi che, venendo dalla Banca d'Italia, avesse una conoscenza economica e non una conoscenza giuridica di questo tipo. Non è una cosa grave, essendo un Ministro tecnico è possibile che conosca una parte del suo mestiere e non tutto. Non è una cosa scandalosa. Stasera ha dimostrato, per esempio, di non conoscere per niente il diritto costituzionale, ma non è una cosa grave: il Ministro dell'economia, infatti, non è il Ministro delle riforme istituzionali,

che esiste nel nostro ordinamento costituzionale una pluralità di organi raccordati con il Governo, il quale non ha il potere assoluto, come poteva avere Gengis Khan nei confronti di tutti gli altri subordinati; il ministro Padoa-Schioppa ha parlato da ministro del Governo di Gengis Khan. Queste cose - bisogna farlo capire - non sono consentite nel nostro ordinamento. Vi è la magistratura, vi sono le Forze armate, i diplomatici, le forze di polizia, le religioni, le autorità universitarie, tutte istituzioni autonome rispetto all'indirizzo del Governo, nei confronti delle quali non vi è la separatezza, ma l'autonomia. È una questione molto seria e, da questo punto di vista, l'ignoranza costituzionale del Ministro è motivo di mia grande preoccupazione di essere governato da un Governo al cui interno il governo dell'economia è affidato ad una persona che non conosce le regole essenziali dei rapporti con le altre istituzioni. Questo è un fatto molto grave, è una questione di grande preoccupazione, in ordine alla quale noi vorremmo onestamente poter avere con il ministro Padoa-Schioppa un confronto un po' più sereno di quello che abbiamo avuto alla luce delle cose che ci ha detto qui stasera. In questo momento a Napoli - ma non solo lì

C'è chi lo vota, ma vorrebbe meno tasse per i poveri imprenditori dell'Alto Adige; c'è chi lo vota volendo una riduzione del costo della politica; c'è chi lo vota dicendo che il Governo sarebbe dovuto intervenire prima; c'è chi lo vota dicendo che Speciale andava cacciato molto prima. Mi chiedo, alla fine, se siamo in presenza di un ordinamento costituzionale serio: ma che razza di voto è quello che avremo tra poco? Un voto nel quale concorrono a dire sì persone che hanno le più svariate motivazioni, soltanto perché hanno paura delle elezioni? Questo è il problema. Occorre che gli amici e i colleghi capiscano che le elezioni non sono un fatto sconvolgente, ma una eventualità normale e pertanto la paura delle elezioni non può motivare argomenti a favore di un Governo con i voti più contraddittori tra loro. Per queste ragioni,

Ma oggi, dopo quello che è avvenuto, vorremmo votare la nostra mozione, nella quale chiediamo che il Governo rispetti la legge, in base alla quale la Guardia di finanza dipende dal Ministro delle finanze e non dal Vice Ministro delle finanze. È possibile chiedere al Governo di rispettare la legge o questo è un fatto eversivo? Lo dico ai colleghi della maggioranza. Chiediamo che il Governo rispetti la legge. Questo chiede l'opposizione. Questo Governo, che ha messo molte mani,

Noi vorremmo evitare che il Governo continuasse nella linea di incostituzionale comportamento nei confronti di tutte le istituzioni autonome. Credo che non chiediamo troppo. Capisco che Padoa-Schioppa possa non capire queste argomentazioni di ordine costituzionale: venga un Ministro che possa capire di questi argomenti e ne parleremo tranquillamente. *(Applausi dai Gruppi

con riferimento all'attacco che le destre hanno mosso nei confronti del Governo e agli insulti rivolti al ministro Padoa-Schioppa, a cui va la nostra solidarietà che un grande concittadino mio e anche del senatore D'Onofrio diceva: «Ogni limite ha una pazienza». Lo diceva Totò. Ecco, Ministro: ogni limite ha una pazienza. Quindi, l'attacco rivolto con toni violenti e con argomenti spesso mortificanti, come abbiamo visto oggi e che i telespettatori hanno potuto hanno potuto notare, è una pagina aspra, dura, preoccupante della vita del Parlamento italiano. Le destre alimentano e coprono politicamente sottofondi bui della nostra Repubblica, loschi figuri legati ai servizi deviati; utilizzano agenzie di spionaggio private, che lavorano insieme ad autorità pubbliche in attività illegittime (questo sta dimostrando); incostituzionali centrali di sovversione di poteri forti. È un armamentario che, purtroppo, la storia della democrazia italiana ha conosciuto e che riemerge torbidamente in una fase di difficoltà, di crisi del Parlamento e della partecipazione democratica. Si tenta di trasformare la politica, il Parlamento in inerti appendici di poteri forti, di cui vediamo solo la punta dell'*iceberg*, ma che sotto la superficie nascondono agenzie di spionaggio private, di intercettazioni, di sofisticate ed il legittimo uso della e LNP)*. E voi tutti lo sapete! Sono le destre a creare, quindi, la vera emergenza democratica; come, del resto, nella scorsa legislatura (lo dico a chi sembra avere poca memoria), alimentati dal Governo Berlusconi, assistemmo agli spettacoli tristi (e, per certi versi, grotteschi) della Commissione Mitrokhin, che indagava - figurarsi - sul fatto che Prodi fosse o meno un agente del KGB della Commissione Telekom-Serbia. Pagine tristi ho detto: chi non ricorda le vicende di Scaramella e di tanti suoi amici faccendieri e spioni? Il nostro allarme democratico è forte, perché si vuole iniettare nelle persone il veleno dell'insicurezza, della paura, della impossibilità di essere governati. Si avvelenano i pozzi, signor Presidente *(Commenti dei senatori Storace e Baldassarri)*, che sono poi i pozzi dell'intera società, per deprimere la partecipazione e far emergere populismo plebiscitario. È questo il vero senso della «spallata», che, ancora una volta, tenta Berlusconi e che noi oggi respingiamo, come ha ricordato la senatrice Gagliardi nel dibattito. E Berlusconi, il grande teorico dell'evasione fiscale, attacca Visco, che considera simbolo della lotta all'evasione fiscale. Pagare tutti le tasse per pagare meno è, evidentemente, una concezione lontana da coloro che hanno costruito la politica fiscale sui condoni, sul rovesciamento della progressività costituzionale, facendo pagare meno tasse a chi più ha. Anche questa è una questione democratica: di fronte ad un'evasione fiscale, contributiva, a cui si accompagna l'elusione, che è 14 volte più alta della media europea (sono indagini ufficiali europee), che equivale annualmente a più finanziarie, che è furto di risorse nei confronti delle classi popolari, che è abbattimento dello Stato sociale e dei servizi pubblici, spingere allo sciopero fiscale, come ha fatto ieri Berlusconi (salvo poi vergognarsene e ritirare le sue affermazioni, ma aveva parlato in diretta televisiva, quindi lo hanno sentito tutti: Berlusconi ha chiamato allo sciopero fiscale), è un attacco allo stesso spirito pubblico

Personalmente ho sempre ritenuto che la Guardia di finanza andasse smilitarizzata e condotta ad un livello massimo di specializzazione; ma ne apprezziamo comunque il ruolo, la funzione, l'operatività.

È evidente che fra il Governo e il generale Speciale si è rotto un rapporto di fiducia. Se il Governo si rende conto che il responsabile di un corpo militare ha commesso errori gravi o atti che ledono il rapporto di fiducia istituzionale, è suo dovere rimuoverlo. Il nostro voto è quindi un atto di fiducia in questo Governo affinché vada avanti, ritrovando una «connessione sentimentale» - come avrebbe detto Gramsci - con il suo popolo. Il Governo sfuggirà agli agguati berlusconiani solo se crescerà il suo consenso sociale. il Governo è debole; se il popolo dell'Unione soffre, si passivizza, si frantuma, si astiene (come ha fatto nelle recenti elezioni amministrative in quartieri operai, proletari, popolari). Il nostro popolo si attende dal Governo segnali precisi di «risarcimento sociale»; la domanda è alta, qualificata, sacrosanta, dopo anni di sacrifici, anni nei quali la centralità del lavoro è stata messa in un cono d'ombra. Occorre un'inversione di tendenza, una redistribuzione delle risorse. Se lo aspetta chi non arriva a fine mese con lo stipendio o con la pensione, chi paga affitti o mutui impossibili, chi non regge più la tensione

Il Governo ha modo e tempo per recuperare. Ma deve fare, da subito, scelte decise; a partire dal Documento di programmazione economico-finanziaria e dall'impostazione della nuova finanziaria. Lotta alla precarietà, aumento delle pensioni basse (non solo minime), salari, stipendi, condizioni di lavoro, salario sociale per ragazze e giovani disoccupati sono alcune delle priorità immediate da iscrivere nell'agenda del Governo; insieme alla tutela dell'ambiente, dei servizi, fondandosi sul paradigma dei beni comuni (acqua pubblica, salute, istruzione, formazione, come griglia di ricostruzione di una più complessa socializzazione). Non possiamo sottovalutare la situazione: la crisi della politica è ormai crisi della rappresentanza; vi è un vuoto politico generale, in Europa e in Italia, ma vi è un vuoto politico grande a sinistra. Questo vuoto politico deve essere colmato da una nuova soggettività organizzata, da una forza di sinistra, in forma confederata, io penso, che unisca le forze, politiche e sociali, delle sinistre alternative. Un percorso, finalmente, di unità, non più di divisioni e frantumazioni, come troppe volte la sinistra ha subìto. Riteniamo che questa sia un'operazione socialmente indispensabile, ma anche di straordinaria innovazione e cultura politica. Vogliamo costruire una sinistra unita, che affronti i grandi temi del lavoro, della condizione di vita, della democrazia, a partire da una legge elettorale che contenga, tra l'altro, come punto qualificante, l'equilibrio della rappresentanza di genere (un uomo, una donna; una donna, un uomo): questa è l'unica vera democrazia. Oggi respingiamo l'attacco strumentale delle destre proprio perché, già da domani, governo e maggioranza possano attuare il programma dell'Unione. È questo l'impegno del Gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea. Grazie

il 3 luglio del 2002 l'onorevole Scajola si dimetteva da ministro perché un giornalista aveva carpito in ascensore una frase dello stesso Ministro. Il 18 febbraio del 2006 il senatore Calderoli si dimetteva da ministro perché aveva indossato un indumento non ritenuto consono dall'opposizione per un Ministro. Il 10 marzo del 2006 l'attuale si dimetteva da ministro per alcune illazioni riportate da giornali senza avere nemmeno ricevuto un avviso di garanzia; il ministro Storace non era nemmeno parlamentare. Tutti e tre, per non danneggiare il Governo di cui facevano parte. Il vice ministro Visco, preso con le mani nel sacco nel tentativo di trasferire degli ufficiali con la complicità sua, signor Ministro, perché stavano indagando su imprese a lui vicine (leggi UNIPOL), oltretutto poco abile, perché nemmeno è riuscito ad ottenere il trasferimento degli stessi ufficiali, è rimasto al suo posto Per usare un termine militare, signor Ministro: fulgido esempio di attaccamento alla poltrona. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).* Apprendiamo, inoltre, che il Governo è intervenuto per far sostituire il direttore dell'ANSA, dottor Magnaschi, perché si era permesso (udite! udite!) di dare la notizia dell'indagine da parte della Guardia di finanza nei confronti dell'UNIPOL. I fatti sono noti: il generale Speciale è stato rimosso (anche su questo c'è poca chiarezza: c'è chi dice che non è stato rimosso, chi con un atto di prevaricazione improvviso proprio di un regime e da vittima è stato trasformato in colpevole: colpevole di non aver commesso il fatto. Mentre il Vice ministro è stato graziato per aver tentato di commettere il fatto e sanzionato con la semplice remissione temporanea della delega sulle Fiamme gialle, pagata la quale potrà ritornare senza colpo ferire a calcare la scena del delitto,

il Presidente del Consiglio ha tentato persino di comprarsi la dignità del generale Speciale, offrendogli in cambio un prestigioso incarico alla Corte dei conti. Gli italiani si sono fatti un'idea precisa sulla responsabilità del vice ministro Visco in questa gravissima e per certi versi inaudita vicenda, un'idea solida, fondata su dati e riscontri concreti sulla illegittimità commessa. Non ci interessa in questa sede - ha ragione la collega Finocchiaro - e non è compito del Senato stabilire se nel comportamento nel comportamento dell'onorevole Visco si possano ravvisare reati amministrativi, penali o civili che siano; ci interessa l'aspetto politico, aspetto politico che è molto rilevante, di inimmaginabile gravità per gli effetti destabilizzanti che esso genera. Non abbiamo qui il tempo per ripercorrere tutti i fatti che dimostrano le pressioni, le ingerenze, l'azione invasiva della sfera delle competenze esclusive del comandante generale della Guardia di finanza esercitate dal Vice Ministro; i colleghi Ramponi, Mantovano, Saporito, Baldassarri lo hanno fatto oggi durante il dibattito. Ma c'è di più, colleghi senatori: le ingerenze dell'onorevole Visco non sono finite nel luglio del 2006 con i falliti trasferimenti dei vertici lombardi delle Fiamme gialle, sono proseguiti anche nel marzo 2007 per una vicenda anch'essa riportata ampiamente sul quotidiano «il Giornale». Questa è la prova del nove che dovrebbe impedire a Visco di restare un solo minuto ancora al Governo. Cos'altro si aspetta per dimissionare un personaggio che voleva porre

nei colleghi dell'attuale maggioranza potrebbe prevalere ancora la spinta all'autoconservazione, ma noi auspichiamo che il buon senso di tanti senatori - e non mancano nel centro-sinistra spiccate personalità - consenta loro un sussulto di coraggio per staccare la spina al Governo Prodi. Salverebbero il Paese da una deriva, dal degrado incontrollato; probabilmente, potrebbero allo stesso tempo salvare anche la loro coalizione dal disastro cui la sta portando l'irresponsabilità del presidente Prodi, che è arrivato privilegiare la politica delle vendette e a colpire l'istituzione militare. Vincerete forse tra poco qui in questa ma non so se vincerete a Genova, a Lucca, a Pistoia, a Latina, a Piacenza dove, domenica, sarete chiamati al ballottaggio.

Mi riferisco, tra le altre, in particolare a quella del presidente Bertinotti che ha preso atto delle conseguenze politiche pesanti che la cattiva gestione della vicenda Visco-Speciale Visco-Speciale comporterà sul Governo e sulla coalizione. Ci sorprendono, invece, alcune dichiarazioni del ministro degli affari esteri, onorevole D'Alema, che tenta di accreditare la tesi che il centro‑destra è diviso sul percorso da effettuare dopo la caduta dell'attuale Governo. Non parteciperemo, signor ministro D'Alema, e soprattutto non useremo mai le notizie riportate oggi da un quotidiano nei suoi confronti. Non è nella nostra cultura buttare fango sull'avversario; ci viene persino voglia di esprimere tutta la nostra solidarietà. Vogliamo il confronto politico e solo quello. D'Alema esca dal fortino in cui l'ha imprigionato l'onorevole Prodi; operi con il coraggio, che certamente non gli manca, nell'interesse dei cittadini. Quando insieme ai suoi più avveduti alleati deciderà di staccare la spina, chiudendo un'esperienza parlamentare per il Paese - ma voglio aggiungere suicida anche per il nascente partito democratico e per tutta la sinistra

nuocere a voi stessi - di questo potremmo anche gioire - e portare il Paese verso una deriva incontrollata e incontrollabile e per questo non possiamo certo gioire. La vicenda Visco è, dunque, gravissima e la ribadiamo, ma non vorrei che la si facesse passare come una questione a se stante, un semplice incidente di percorso del Governo; sarebbe riduttivo rispetto alla situazione generale disastrosa che Prodi, il suo Governo e la sua maggioranza hanno determinato. La vicenda Visco è solo lo specchio attuale di un Esecutivo diviso e politicamente debolissimo, entrato in rotta di collisione con la stragrande maggioranza degli italiani. Siamo convinti che se non fosse stato così debole, Prodi non avrebbe posto in essere un atto inaudito come la rimozione senza giusta causa del comandante della Guardia di finanza. Se il Governo fosse stato forte avrebbe tolto le deleghe al vice ministro Visco. La politica ha una sua logica. Onorevole Ministro, lei quest'oggi ha usato un termine nel suo intervento: «La Guardia di finanza ha bisogno di un sovrappiù di certezza morale». Qual è il sovrappiù, onorevole Ministro? Ordinare il trasferimento di ufficiali che stanno indagando sugli amici? Con il suo intervento lei è stato capace

dalla Guardia di finanza e assoggettare la stessa e la Corte dei conti per governare senza controlli. Lei afferma inoltre nel suo intervento di ritenere di aver combattuto in difesa della legge. Signor Ministro,

Non me ne voglia, signor Ministro, per quello che sto per dire ma l'impressione che questo Governo dà non è quella di un Governo coeso, composto da Ministri che dialogano e poi decidono, bensì quella di un Governo formato da complici che a vicenda intervengono per nascondere le rispettive marachelle. Eppure è un Governo composto da uomini politici di grande esperienza, anche bravi in politica - li combattiamo perché abbiamo idee diverse - e certamente protagonisti della vita politica di questi ultimi anni. Basterebbe riflettere su questo perché uomini di tal fatta restano in questo Governo con un Ministro come lei che oggi ha dimostrato di essere la vergogna di questo Paese. MATTEOLI *(AN)*. Lei non ha chiarito nulla; ha solo pronunciato frasi pesanti contro il generale Speciale al limite dell'offesa:

ad elezioni anticipate. Qualora ciò non fosse possibile siamo disponibili ad un confronto, ma solo quando questo Governo avrà sgomberato il campo, e solo allora.

questa vicenda parte dal lontano 1997, quando l'allora ministro Visco provò già - era comandante generale della Guardia di finanza il generale Mosca Moschini - ad occuparsi di progressione di carriere ed impiego del personale della Guardia di finanza. qui una lettera del ministro Visco dell'epoca attraverso la quale chiedeva in punta di piedi, riconoscendo di non essere competente ad occuparsi di questa materia, di essere preventivamente informato di quello che avrebbe fatto il comandante generale dell'epoca.

Questo Governo, per la prima volta nella storia, decide di delegare i rapporti con la Guardia di finanza ad un proprio Vice ministro. Signor Presidente, non era mai successo; non ci sono precedenti anche perché credo che la norma

tanto è vero che arriva ad una situazione di confronto duro con un galantuomo, il generale Speciale, che paga la colpa di avere difeso la Guardia di finanza dall'ingerenza di un potere politico. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e ministro Visco, che contesta al generale Speciale di avere comunicato troppo tardi gli atti di impiego del personale, arriva a scrivere del personale, arriva a scrivere che eventuali, ulteriori ipotesi di designazione dovranno avvenire solo all'esito di un preventivo e approfondito confronto sulle motivazioni delle stesse con l'autorità politica.

gli atti del tentativo di decapitazione dei vertici della Guardia di finanza della Lombardia, signor ministro Padoa-Schioppa, ci aspettavamo di più da lei: lei è un grande economista, ma probabilmente non un perfetto politico, perché si è prestato a rendere voce ad un Governo che si è reso protagonista in questi giorni dell'atto più efferato contro la tenuta delle istituzioni del nostro Paese.

(lei o il suo *dossier*) che il Corpo di comando della Guardia di finanza della Lombardia andava rimosso perché permaneva in quei ruoli da troppo tempo. Non è così: parlano gli atti. Ebbene, il Vice ministro, avendo addirittura deciso di occuparsi di questi trasferimenti di autorità, perché andava punita quella Regione, Regione, all'insaputa del comandante generale della Guardia di finanza convoca i bracci destri di quest'ultimo (il vice comandante ed un altro generale) chiedendo loro di suggerire al comandante generale la decapitazione dei vertici della Guardia di finanza. Ebbene, queste sono le lettere di questi due galantuomini che dichiarano di essere stati convocati dal Vice Ministro e di avergli detto che non avevano elementi per potere giustificare quei trasferimenti. Questo è su carta.

Lei ha detto, signor Ministro, che il generale Speciale non si è avvalso mai del Consiglio superiore della Guardia di finanza per la realizzazione dell'impiego del personale. Signor Ministro, ma noi conosciamo le funzioni di questo Consiglio superiore della Guardia di finanza, questo Consiglio superiore della Guardia di finanza, che si occupa di ben altro, quando si parla di personale: si occupa di aspetti ordinamentali del personale, vale a dire di stabilire gli organici e le metodologie di progressione di carriera, e non di trasferimenti e di promozioni. Il generale Speciale, quando si è occupato di questa materia, ha avuto sempre il consenso - previa concertazione - di tutti i generali di corpo d'armata, che hanno messo nero su bianco l'adesione all'impiego del personale. Le regole non sono state mai violate da questo galantuomo.

Ebbene, apprendiamo in quest'Aula, in questa casa degli italiani, che oggi l'imputazione penale costituisce la morte della carriera di una persona quando ancora deve essere condannata. *(Applausi dal Gruppo FI).* Che grande garanzia effettivamente sancisce questo Governo. Per non parlare del decreto, signor Ministro: un grande pasticcio - ci consenta - privo di precedenti. Avendo dimenticato di fare una revoca espressa del generale Speciale, vi siete inventati un atto che conterrebbe una revoca che non c'è. La verità è un'altra. Voi, presi dalla frenesia di realizzare questo esasperato strappo delle regole, di mandare a casa il generale Speciale (perché oggi, altrimenti, sareste caduti attraverso i voti della vostra stessa maggioranza che avrebbe votato contro il Governo), avete compiuto un atto privo di motivazioni. Non si capisce per quale motivo sia stato esautorato il comandante generale della Guardia di finanza, quando quest'atto è un atto di alta amministrazione, come lei stesso lo ha definito, e lei sa bene che la Corte costituzionale ha previsto che per gli atti di alta amministrazione occorra una motivazione che vada al di là della perdita del rapporto di fiducia tra potere politico e comando generale. Occorre valutare attentamente l'azione del comando generale, non basta la perdita di fiducia perché il comando generale della Guardia di finanza non può essere asservito alla volontà politica di un Governo che, attraverso il proprio Vice ministro, voleva attuare un disegno. disegno. La verità è una sola: attraverso l'utilizzo, gli spostamenti, le promozioni, i trasferimenti di ufficiali della Guardia di finanza si decide se trasferire quel comandante in quel ruolo in cui ci si occupa o no di polizia giudiziaria e attraverso eventuali spostamenti si punta ad avere uffici amici che occupandosi di polizia giudiziaria possano avere un controllo delle indagini della magistratura, un controllo indiretto della magistratura, un asservimento indiretto della magistratura, attraverso la conoscenza preventiva delle sue indagini.

non un servitore dello Stato, un pericolo per lo Stato, così come è stato disegnato da questo Governo tanto da meritare la defenestrazione nel giro di due ore, ma come lo si può mandare alla Corte dei conti, un organismo che si occupa del controllo della spesa pubblica, della spesa di tutti gli italiani? C'è qualcosa che non capiamo, che ci sfugge, signor Ministro, e lo dovete spiegare al Paese, perché voi al Paese purtroppo questa spiegazione non l'avete data. Il Paese è preoccupato, perché si trova in balia di un Governo che esercita il proprio potere istituzionale per risolvere i propri problemi di sopravvivenza; questo è il dramma che vivono gli italiani. Allora, avete sacrificato prima un galantuomo, che cade sull'altare della sopravvivenza del vostro Governo, prima ancora avevate compiuto un altro strappo offendendo la dignità del nostro Paese, quando per salvarvi avete chiesto al Presidente dell'Afghanistan di trattare con i talebani per liberare dei terroristi pur di non cadere e rimanere a casa. *(Applausi dai Gruppi FI, ricordiamo tutti e che il nostro Paese pagherà e sta pagando, perché la dignità internazionale che avevamo acquisita in cinque anni di nostro Governo non ce l'abbiamo più e ce la possiamo scordare perdurando questo Governo. Vede, signor Ministro, è sufficiente girare il Paese, non basta commentare i dati delle precedenti elezioni amministrative che vi hanno dato una forte segnale, il Paese non è più con voi; e non basta che lei all'inizio del suo intervento si sia preoccupato di recuperare i voti di qualche dissidente di un partito di maggioranza che lamenta l'eccessiva pressione fiscale: hanno la nostra solidarietà i colleghi che lamentano questo stato di cose e si associano a tutta l'opinione pubblica che non ne può più. DCA-PRI-MPA).* I cittadini si identificano in un Governo quando si sentono rappresentati da quel Governo, non quando si sentono offesi da un Governo che li tassa e li vessa. Infine, per concludere, l'ipocrisia e le contraddizioni di un Governo che presenta in quest'Aula del Parlamento un documento attraverso il quale si elogia il ruolo della Guardia di finanza, ma non i suoi uomini: è una minaccia di epurazioni? Noi siamo con la Guardia di finanza, noi siamo con gli uomini della Guardia di finanza, con tutti coloro i quali quotidianamente rischiano la vita per la collettività, per gli interessi del Paese: viva la Guardia di finanza, viva gli uomini della Guardia di finanza!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, ho riflettuto su questa dichiarazione di voto, non certo perché avessi dubbi sulla correttezza dell'agire del Governo, né tanto meno su quella dell'agire del vice ministro Visco,

Scusatemi del richiamo. Prego, senatrice mi ha confermato nel giudizio e mi ha rassicurato ulteriormente. Condivido quella decisione politica, la condivide il mio Gruppo, apprezzo la responsabilità istituzionale del vice ministro Visco che ha rassegnato le deleghe, condivido peraltro interamente l'intervento del senatore Zanda, di cui questo vi prego

In questa discussione si ha la sensazione di aver smarrito un quadro comune di riferimento, un comune affidarsi ad un sistema di regole che disegna i poteri, i doveri, le responsabilità, gli ambiti di competenza, che in qualche modo assesta una storia, un percorso, un processo che ha attraversato il tempo delle istituzioni repubblicane e che prescinde dalla maggioranza. Una storia comune che regola ogni conflitto, anche il più aspro, e che mostra sempre la via d'uscita rispetto alla crisi, al contrasto, e che ci impedisce di varcare il recinto permettendoci di evitare l'impazzimento della discussione e le sue conseguenze sul sentimento di fiducia e di affidamento dei cittadini nelle istituzioni e nella politica. Credo che ogni critica, anche quella asprissima, ad una decisione politica debba stare dentro un quadro regolato altrimenti è l'impazzimento, ma è anche qualcosa di più preoccupante. Colleghi, non voglio dare lezioni, offro solo una riflessione che che forse potrebbe rappresentare la parte più fruttuosa della discussione odierna. Mi perdonerà il senatore Calderoli se per spiegarmi meglio prenderò le mosse da una sua dichiarazione di stamattina. Oggi il senatore Calderoli ha affermato che il problema è che non si può prescindere da un ruolo di Napolitano (sic). «Emerge proprio oggi» - dice il collega Calderoli - «che l'atto con cui si è proceduto a questa nomina è un decreto del Presidente della Repubblica che può firmare o non firmare un atto. Inoltre, la Guardia di finanza è un corpo che appartiene alle Forze armate e il massimo vertice delle Forze armate è il Capo dello Stato. È la Costituzione stessa che lo dice». Una dichiarazione che molti dei nostri concittadini, e probabilmente molti dei nostri colleghi, assumono come fondata su un sistema di regole e che invece non è affatto fondata sul sistema di regole vigenti e rischia di portare la discussione fuori dal quadro di riferimento che disciplina la materia e che dovrebbe disciplinare la discussione tra di noi. Non si tratta, come dice il presidente D'Onofrio, di ignoranza istituzionale. Sono ben certa che il senatore Calderoli conosca perfettamente le regole che disciplinano la questione e che volutamente le ignori, ignori la Costituzione, ignori le leggi, ovvero le tradisca.

formale e che la responsabilità dell'atto sia tutta del Consiglio dei ministri e che il Presidente della Repubblica non può rifiutare l'emanazione se non per attentato alla Costituzione. Inoltre, tutti sappiamo che la Guardia di finanza non è un Corpo che appartiene alle Forze armate, ma è un Corpo di polizia ad ordinamento militare - lo dice la legge - che dipende direttamente dal Ministero delle finanze e non della difesa e il comandante della Guardia di finanza non è componente del Consiglio supremo di difesa, presieduto dal Capo dello Stato, né del Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate. Queste cose, colleghi, le sapete meglio di me. Ma allora perché rompere il recinto di una discussione regolata da ciò che è scritto nella legge e nella Costituzione? Perché coinvolgere in un dibattito, legittimamente aspro, poteri, funzioni, istituzioni che non hanno relazione con l'oggetto politico del dissenso? Secondo me non ne viene affatto una maggiore forza alla vostra argomentazione, ma ne viene confusione, distruzione, smarrimento nei cittadini. La questione che sto ponendo, colleghi, e che vale identicamente per voi e per noi, è che fuori da una contesa regolata da un sistema politico e istituzionale c'è solo il pericolo di un cedimento complessivo del sistema democratico. Quel sistema resta in equilibrio solo se le regole governano anche il conflitto altrimenti l'equilibrio, divenuto instabile, è ristabilito ogni volta in maniera diversa e non dai poteri previsti dall'ordinamento ma in base a rapporti di forza non controllabili, imprevedibili, talvolta addirittura spuri. Voi volete giudicare politicamente l'operato del Governo: fatelo! Siamo qui per questo da stamattina. Abbiamo preteso noi, questa mattina, contro alcuni di voi che volevano rinviare il dibattito, che la discussione si facesse qui, pubblicamente, davanti a tutti gli italiani con la diretta televisiva. Lo abbiamo chiesto proprio per tale motivo, perché questo è il luogo: il luogo: il recinto disegnato dalla Costituzione e dai Regolamenti parlamentari; qui dove si celebra il vostro diritto ad esporre le vostre ragioni e dove il vostro attacco al Governo può essere più chiaro, più trasparente e più diretto; che, in democrazia, è il luogo della responsabilità di maggioranza, di opposizione e di Governo. Davvero stupisce che questa mattina alcuni Gruppi del centro-destra non volessero più il dibattito odierno, ma noi siamo qui e voteremo con le regole che governano il lavoro, il funzionamento e l'espressione democratica del voto delle Aule parlamentari. Voglio

il ruolo ed il lavoro della Guardia di finanza e delle Forze armate. Per tale motivo, l'opposizione non ha reso un buon servizio alla Guardia di finanza tentando di arruolare il generale Speciale nelle sue fila.

e se ciò cui abbiamo assistito negli ultimi giorni e qui stasera, in quest'Aula, durante l'intervento del ministro Padoa-Schioppa, e davanti agli italiani, non ne sia la prova conclamata.

Prima di passare alla votazione, per la quale prego i colleghi di prendere e e mantenere i propri posti per rendere più facile l'esercizio del diritto di voto, ricordo che le mozioni e gli ordini del giorno saranno posti ai voti secondo l'ordine di presentazione. Per il voto dei documenti resta stabilito che esso si riferisce alle parti eventualmente non precluse o assorbite da precedenti votazioni.

Presidente, avremmo preferito, anzi ne saremmo stati ben soddisfatti, se il vice ministro Visco avesse avvertito l'esigenza di venire in Parlamento a spiegarci il perché dei suoi comportamenti, anziché affidarsi a una relazione del ministro Padoa-Schioppa. Ciò non è avvenuto, anche se in passato Ministri di altre legislature, in presenza di mozioni di sfiducia, hanno assunto hanno assunto l'iniziativa di difendersi davanti al Parlamento quando erano sfiduciati dalla loro stessa maggioranza, pensi un po'. Questo silenzio è imbarazzante e lo definirei quasi assordante, perché certo non fa onore alla storia della nostra democrazia e al ruolo del nostro Parlamento. del nostro Parlamento. Con questo atto chiediamo al Governo di ritirare al vice ministro Visco tutte le deleghe, non soltanto quella relativa al rapporto con la Guardia e di attenersi al rispetto delle regole procedimentali per quanto riguarda l'adozione di un provvedimento di revoca di un Comandante generale della Guardia di finanza,

questo caso non sia in ballo la vita del Governo, tuttavia con questa mozione si esprime fiducia all'operato della Guardia di finanza e ai suoi vertici che, per dichiarazione dello stesso Ministro, è oggi presieduta da persona diversa

ma ai colleghi della maggioranza che hanno la possibilità di ragionare con la loro testa: si tratta di dare o meno la fiducia alla Guardia di finanza. Non chiedo un voto a favore, ma per lo meno non prendano parte a questa votazione, se non se la sentono.

Questo vizio di urlare proprio non riusciamo a togliercelo. Non ci riesco io, sono un incapace io; continuo a dirlo, non ci riesco!

e a promuovere una politica di riduzione fiscale e di sostegno delle fasce più deboli». Cosa possa esserci di strumentale in un ordine del giorno del genere, qualcuno me lo spieghi.

Presidente, lei ha giustificato il mancato assorbimento della votazione precedente, dicendo che l'apprezzamento e la solidarietà sono due cose diverse.

che influenza questa votazione, da cui dipende la vita di questo Governo. Presidente, non vi è dubbio che quell'ordine del giorno è precluso e non capisco nemmeno il perché

è stata una giornata di dibattito; ci sono state le dichiarazioni di voto, i vari voti e non vi è dubbio che la maggioranza ha ottenuto, durante le votazioni, un risultato positivo per quanto la riguarda. Non vedo perché lei debba fare la forzatura di mettere in votazione un ordine del giorno precluso. Allora, Presidente, mi consenta: se lei insiste nella votazione e non vuole annullare la votazione stessa perché è stato un voto illegittimo, si riunisca la Giunta per il Regolamento perché non ci possono essere precedenti precedenti di questa natura. L'ordine del giorno è precluso, lo è per tutti e deve esserlo anche per lei. Non è possibile uscire da questo dibattito, facendo votare un ordine del giorno sicuramente precluso. Voglio dire ai colleghi della maggioranza che vincere è bello, ma se si vuole supervincere, si rischia di perdere, perché hanno vinto la loro battaglia. Glielo riconosco; ancora una volta ottenuto la maggioranza in questo consesso. Non è possibile, però, andare oltre e chiedere un voto su un ordine del giorno sicuramente precluso. Presidente, questa è una provocazione peggiore di quella che ha fatto il ministro Padoa-Schioppa oggi.

per il voto dei documenti resta stabilito che esso si riferisce alle parti eventualmente non precluse o assorbite. Un ordine del giorno esprime solidarietà ed apprezzamento alla Guardia di finanza;

significando all'Aula che si mette in votazione la parte non cassata. Lo deve chiarire, perché in questo modo lei ha messo in votazione un principio sul quale l'Aula si era già pronunciata.

Per il voto dei documenti resta stabilito che esso si riferisce alle parti eventualmente non precluse o assorbite

credo che la sua ultima decisione sia quella corretta e anche perfettamente in linea con quanto ha dichiarato prima. (*Commenti dai

Avete dichiarato che votavate contro un provvedimento in quanto strumentale, ma non esiste l'approvazione su un testo strumentale o non strumentale. Vi siete presi la responsabilità legittima

questa maggioranza non apprezza la Guardia di finanza. Questo è il dato.

Signor Presidente, in questa confusione non mi risultava molto chiara l'argomentazione che lei aveva adoperato in un primo momento, primo momento, relativa al fatto che il contenuto dell'ordine del giorno (qui non stiamo ragionando di una norma, ma di un ordine del giorno presentato dalla maggioranza), parole «condivide l'operato del Governo ed esprime pieno apprezzamento», ovviamente allude ad un contenuto politico diverso da quello recato dall'ordine del giorno presentato per carità, lei ha deciso, signor Presidente, e noi ci rimettiamo alla sua decisione, ma poiché mi pareva che questa fosse una notazione che era sfuggita ai colleghi dell'opposizione, mi premeva farla rilevare. Voglio dire, tra l'altro, che i colleghi dell'opposizione gioiscono, e io capisco che ciascuno si accontenta,

e che lei non ha il diritto di ignorare sistematicamente le domande di presa di parola da parte di membri di questo Gruppo. Mi pare un atto molto grave. In secondo luogo, vorrei far osservare che sarebbe stato bello chiudere questo dibattito col Parlamento unito nell'esprimere apprezzamento alla Guardia di finanza *(Applausi dal Gruppo FI)*, che mette il suo impegno per salvaguardare il patto fiscale degli italiani. È gravissimo che possa sorgere il dubbio che venga orientata a violare questo patto contro i nemici e ad applicarlo con maggiore *souplesse* verso gli amici. La maggioranza questo non lo ha voluto e non può sottrarsi a tale responsabilità. La maggioranza ha rifiutato la possibilità di esprimere insieme l'apprezzamento alla Guardia di finanza. Di più, la maggioranza esprime un principio mussoliniano: fu Mussolini, se ricordo bene, a dire che quello che fa l'opposizione è irrilevante, anche se ci proponeste le cose che diciamo noi, non vanno bene per il semplice fatto che le proponete voi. L'opposizione non è considerata come oggetto di un dialogo, anche aspro, in visione di un bene comune del Paese, ma come qualcosa con la quale non ci si deve contaminare: non importano i contenuti, importano solo le firme di quelli che propongono il documento. Del resto, l'attuale Governo ci ha già abituati al fatto che è possibile venire in Italia e chiedere di comprare Telecom e sentirsi dire di no, tornare insieme con gli amici del Governo e allora ci si sente dire di sì. Credo che la maggioranza abbia fatto qualcosa di dannoso per l'interesse del Paese e abbia leso il prestigio e la dignità del Senato. chiarimento ulteriore; io richiamo quello che è stato dichiarato prima dell'inizio del voto: che per il voto dei documenti, resta stabilito che esso si riferisce alle parti eventualmente non precluse e assorbite. Non c'è dubbio che l'ordine senatore Calderoli, esprimeva apprezzamento e non è stato approvato. Allora il documento approvato, che dice chiaramente (non c'è ombra di equivoco su questo):

Signor Presidente, riteniamo opportuno recuperare la proposta del senatore Buttiglione e invitiamo il Senato a far proprio unanimemente l'apprezzamento per la Guardia di finanza.

Signor Presidente, vorrei, se fosse possibile, intervenire.

Sono sensibile agli argomenti che sono stati qui proposti dal collega Buttiglione. Vorrei rappresentare al Presidente del Senato un problema che pongo come mio personale e che riguarda i miei diritti di parlamentare. Sono qui, in quest'Aula; condivido un ordine del giorno nella sua unitarietà e intendo votarlo poiché in esso sono contemporaneamente espressi due concetti che non possono essere separati l'un dall'altro. Se mi chiedete di condividere un documento che sia amputato dell'approvazione delle scelte del Governo, io non lo voto, ma se mi chiedete di approvare e votare un documento che sia amputato di una parte che io considero essenziale, voi negate il mio diritto di parlamentare di formulare un voto che contempli l'insieme di quell'ordine del giorno.

rispetto alle dichiarazioni che sono nei Resoconti del Senato, equivoco non ci può essere formalmente.

contestare il diritto del senatore Massimo Brutti a votare un ordine del giorno che raccolga ambedue le sue considerazioni, ma ritengo che in termini procedurali la sua decisione sia ineccepibile, perché una volta respinto l'ordine del giorno Calderoli, che esprimeva apprezzamento per la Guardia di finanza, è assolutamente preclusa la seconda parte dell'ordine del giorno, presentato dalla maggioranza, che riesprime apprezzamento per la Guardia di finanza. se un problema politico esisteva, doveva andare un po' al di sopra del clima da stadio che c'è stato questa sera e doveva indurre i colleghi della

io capisco le ragioni politiche, le ragioni di opportunità, le dichiarazioni che si fanno. Il voto formale, però, non lo cambio perché non c'è da avere dubbi su ciò che è stato votato. Deve essere chiaro.

Presidente, proprio per stigmatizzare la vicenda, se una persona legge sul giornale che qualcuno utilizza un termine e lo riprende in quattro ordini del giorno, e quella persona poi presenta un ordine del giorno di maggioranza, riutilizzando quel termine, mi si scusi, ma fa proprio la figura del pollo, perché se l'è cercata. Ad ogni modo,

Do lettura dell'ordine del giorno G13: «Il Senato, udito il dibattito odierno, esprime fiducia sull'operato del vice ministro Visco e impegna il Governo ad intraprendere iniziative amministrative contro gli ufficiali della Guardia di finanza che, nell'ambito dell'autonomia loro garantita, non si dimostrino asserviti alle direttive dell'Esecutivo». *(Applausi

Il Regolamento prevede che le decisioni del Presidente del Senato siano inappellabili e io non intendo tornarci sopra. Voglio però aggiungere due concetti. Il primo è che noi (giustamente, a mio avviso) abbiamo votato contro l'ordine del giorno G9,

esprimiamo piena solidarietà alla Guardia di finanza nella sua lotta contro l'evasione fiscale e contro coloro che parlano di sciopero fiscale e che invitano i cittadini a non pagare le tasse.

Mi consenta di intervenire: non mi intimidisca, per così dire. Ho molta ammirazione per il senatore Salvi però, esattamente come il senatore Massimo Brutti, credo di avere anch'io il diritto di parlamentare.

Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, visto il modo con il quale sono stato trattato. Ho chiesto prima la parola e mi dispiace, presidente Marini, perché mi considero un suo vecchio e caro amico, ma non si è comportato con la stessa reciprocità; mi dispiace doverlo riconoscere.